È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà. Governo, senatori, è l'ora di cambiare le regole di finanza pubblica soprattutto se prevale una finanziaria di stampo elettorale di ben 1.365 commi e senza riforme strutturali. Tanto valeva forse fare una lotteria con l'estrazione a sorte degli emendamenti di presentazioni parlamentari. Essa giunge in Aula senza relatore e senza un testo della Commissione, fatto questo già di per sé eccezionale. Purtroppo, senatore Morando, non siamo alla Camera dei comuni. Non c'è un cancelliere dello scacchiere capace di affrontare il confronto parlamentare. Qui di Ministri dell'Economia non abbiamo visto neppure l'ombra.

Questo vostro fallimento è anche il frutto della incapacità di valutare appieno il significato politico del risultato elettorale di aprile del Senato. Avete sovraccaricato il convoglio che è affondato. Non volete prendere atto di un equilibrio politico precario e della composizione eterogenea che vi impedisce di affrontare i problemi reali del Paese. Una legge finanziaria sbagliata ed inutile perché poggiava sulle errate valutazioni della *due* *diligence* che ha portato ad una catena sequenziale di errori; una finanziaria che contraddiceva il DPEF di luglio, da parziale compressione della spesa si è passati ad una tutta tasse; le indicazioni di una finanziaria che alteravano il rapporto entrata-spesa squilibrandosi fortemente nel prelievo, senza considerare di alcun rilievo il maggiore gettito, senza correggere la sua impostazione di fondo. Rivendichiamo il merito come UDC di avere privilegiato il confronto parlamentare serio e costruttivo che ha portato ad ottenere un grande risultato: quello della trasparenza dei conti pubblici facendo una operazione di verità sulla dinamica delle entrate fiscali. Solo la nostra azione ha permesso di evidenziare maggiori entrate per 34 miliardi di euro fino al 30 novembre che devono essere incorporate nel bilancio senza trucchi contabili. Abbiate il coraggio di riconoscere con serietà ed obiettività di giudizio che non di buco di bilancio si tratta ma di autentico *boom* delle entrate e che Tremonti vi ha lasciato un tesoro, che state per usare in malo modo, in mille rivoli assistenzialistici.

Queste maggiori entrate sono state pagate dai cittadini italiani, da contribuenti onesti, da quei contribuenti che con la vostra manovra volete ulteriormente torchiare. È questa la prospettiva che si apre e che si unisce al rischio di soffocare la ripresa. Come potete non sorprendervi delle contestazioni vaste e diffuse nel Paese che vanno da Mirafiori ai ricercatori di Bologna e a quelli di Carini, dai piccoli imprenditori e dagli artigiani di Vicenza fino ai giovani del Motor che hanno visto, in una ingiustificata presenza del Presidente del Consiglio, un'invasione di campo mediatica e provocatoria? Non vi sfiora neppure il dubbio della vostra inadeguatezza a comprendere un così imponente disagio che si manifesta in tutto il Paese e che muove dalla classe lavoratrice a Mirafiori, nel cuore pulsante del movimento operaio, e che si sente tradita dalle vostre scelte improntate a logiche scambiste? Avevamo anticipato noi già in Commissione, ben prima della presa d'atto del *leader* della CGIL Epifani, che la ondeggiante e contraddittoria decisione sulla rottamazione penalizza i più poveri e i più deboli, spingendo verso mezzi pubblici che sono totalmente inquinanti. Alla pubblica amministrazione non date soluzioni in termini di efficienza di competitività e di neutralità, ma date una risposta tardosessantottina come è, appunto, il tentativo di stabilizzare il precariato usando demagogicamente i depositi dormienti che in quanto risparmio dovrebbe andare semmai alla comunità locale e non ad operazioni di questo tipo. Manca la copertura del contratto degli statali per il 2007, cifrata in 2 miliardi di euro. Non serve unificare gli Uffici del bilancio di Camera e Senato se le eccellenti analisi non vengono tenute nella debita considerazione. II problema, allora, è dei poteri, di quali poteri attribuire alla Commissione bilancio rispetto a «coperture *cabriolet*» sempre all'interno dei fondi di dotazione del Parlamento, naturalmente. Proponete una riforma dell'IRPEF con limiti e contraddizioni. Non si affronta il problema del quoziente familiare. Non si dà quindi una risposta alla denatalità in un orizzonte di lungo periodo. La funzione redistributiva è veramente esigua. Non tocca infatti né le fasce povere della popolazione, né la platea degli incapienti. Non incidete sulla linea della povertà che passa da 11,89 a 11,79 per cento, perché trascurate le famiglie povere e i pensionati. La manovra dei redditi appare demagogica perché la redistribuzione in realtà è molto modesta, la esiguità redistributiva, come ho dimostrato in Commissione, sul reddito familiare disponibile equivalente passa da 0,343 a 0,3402. Avete dato risposte classiste e risarcitorie a una società articolata e complessa, accrescendo le ingiustizie e le disuguaglianze anziché diminuirle perché poggiavano su impostazioni monche e fuorvianti, come ricordava Sylos Labini. Avete fatto retorica giustizialista, colpendo il ceto medio produttivo e privilegiando scelte antagoniste. Per dare soluzione ai vostri errori sul regime fiscale delle successioni e donazioni e per salvaguardare la posizione dei fratelli, che fate in minima parte con una franchigia di euro 100.000 assolutamente risibile, e i passaggi generazionali delle imprese nella loro continuità, come noi sostenevamo, avete tentato di operare un riconoscimento surrettizio delle coppie di fatto e dei PACS attraverso un tarlo fiscale, attribuendo un privilegio fiscale e creando uno *status* parafamiliare che non esiste nell'ordinamento e che minava il principio costituzionale dell'articolo 29 della società naturale fondata sul matrimonio, non di quella innaturale. È una realtà che non si può né menomare né mutare. E' una chiara delimitazione di limiti, disse Aldo Moro, ma abbiamo sentito il silenzio in Commissione dei colleghi della Margherita. Abbiamo dunque bloccato le vostre scelte. Chiediamo il rispetto di quel modello di famiglia e di quel vincolo. I diritti di libertà sono garantiti. Non c'è alcuna discriminazione. Non possono però essere tutelate figure giuridiche in contrasto con le scelte dei Costituenti. Nessuno vieta ai conviventi di stipulare accordi di tipo privatistico. Vi preoccupate delle unioni di fatto e dei PACS, ma non dei loro figli, dei deboli, degli indifesi, non tutelati da scelte individualistiche ed egoistiche. Volete una famiglia volatile, precaria, con soli diritti e nessun dovere. Chi pensa ai figli? Avete espropriato il TFR dei lavoratori, i quali dovranno decidere la scelta strategica del loro futuro pensionistico in un quadro fiscale non definitivo e senza la riforma degli ammortizzatori sociali. Ciò consente solo al Governo di fare cassa. Incidete sulla struttura patrimoniale delle imprese con maggiori costi finanziari penalizzandole nella loro crescita dimensionale. La stessa operazione cuneo fiscale, che rappresentava un punto di forza della politica economica, opera in modo poco incisivo perché si è scelta la strada di ridurre il cuneo attraverso il fisco e non passando per le componenti di assicurazione e previdenza. Sembra più assimilabile ad una svalutazione competitiva che a una misura strutturale capace di liberare risorse per renderle competitive, liberandole da una zavorra. L'aumento dei contributi previdenziali è poi in palese contraddizione con la riduzione del cuneo, essendo una componente del cuneo stesso. Anziché ridurre il *deficit* infrastrutturale lo aggravate con la vostra incapacità di dare soluzioni alle grandi opere, come le direttrici europee Torino-Lione e Palermo-Berlino, vanificando i cofinanziamenti europei. Sulla Torino-Lione si gioca lo sviluppo e quindi il destino di tutte le Regioni settentrionali e del loro apparato produttivo. Per il ponte di Messina si tratta invece di una sfida tecnologica imponente, capace di attrarre investimenti e promuovere sviluppo e occupazione. Avete preferito la strada di nuovi balzelli di ogni tipo, imposte dirette, indirette e contributive, un'autentica grandinata che farà innalzare la pressione fiscale. Con le vostre imposte di scopo colpite pesantemente il bene casa: il risparmio degli italiani. Il settore immobiliare viene colpito sulla base del valore dei beni

Colpite il risparmio degli italiani con il riordino della tassazione che spingerà verso la liquidità. Le vostre decisioni non sono funzionali al Paese ma alla composita ed eterogenea coalizione con illusioni finanziarie che dilatano la spesa pubblica e soffocano la ripresa. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'assalto alla diligenza ha portato a microinterventi privi di qualsiasi razionalità, senza privilegiare obiettivi seri di sviluppo. Le vostre divisioni impediscono qualsiasi riforma sulla previdenza, sul pubblico impiego e sui problemi reali del Paese. Solo il settore agricolo possiamo dire che ha avuto attenzione adeguata. È assente qualsiasi progetto qualsiasi liberalizzazione. Sostenete i settori maturi e gli amici degli amici, piuttosto che puntare su politiche di innovazione e di competitività. È dunque una finanziaria senza obiettivi, l'esaltazione non dello Stato regolatore, ma dello Stato intermediario del consenso politico e invadente nella sfera delle libertà economiche e sociali. Quella che proponete è una navigazione senza rotta, perché avete fatto troppe promesse elettorali e non siete in grado di soddisfarle tutte: l'opinione pubblica lo ha avvertito con grande consapevolezza; ciò che la maggioranza e il Governo non riescono invece ancora a comprendere. Quindi, non c'è né equità né sviluppo, ci sono solo tante tasse. Quando lo comprenderete sarà troppo tardi. Quello che è indiscutibile è che non avete più la fiducia del Paese:

sulla finanziaria e sulle possibili soluzioni atte a renderla più attinente alle esigenze e ai bisogni del Paese, ci siamo trovati, con l'ennesima mortificazione dei principi parlamentari, chiamati a votare e ad esprimere il nostro giudizio sul preannunciato maxiemendamento, onnicomprensivo di oltre 1.300 commi, un vero record, il cui voto, di fatto, cancella ogni possibilità di dialogo tra le diverse espressioni presenti in Parlamento. Esiste - io credo - un consenso largo tra tutti noi sul fatto che il risanamento finanziario sia necessario per il nostro Paese, non solo perché ce lo impone l'Unione Europea, ma anche e soprattutto per la necessità di creare le basi per una crescita più solida del nostro Paese. Ma il problema che esisteva ed esiste è quello di conciliare il risanamento con la crescita e lo sviluppo. Tuttavia, se dovessimo giungere ad attuare questo risanamento, attraverso misure che, colpendo i settori produttivi e vitali della nostra economia, di fatto ne bloccassero la crescita e ne minassero le fondamenta, allora, il risultato ottenuto non solo sarebbe garantito, ma anche gli effetti positivi che apparentemente potrebbero presentarsi non sarebbero che degli effimeri palliativi se proiettati nel lungo periodo, come a dire che la cura adottato, ha guarito la malattia uccidendo il malato. Cari colleghi della maggioranza, il Governo Berlusconi in questi anni si è posto questo problema e la cautela adottata nel far ricorso a politiche fortemente caratterizzate da artifizi e misure fiscali spinte, in un contesto economico generalizzato di forte flessione, scaturiva dalla considerazione che un uso così eccessivo della leva fiscale avrebbe generato più danni che altro. Ed è proprio questo il punto di debolezza di questa finanziaria, tutta incentrata su manovre fiscali e aumenti della pressione tributaria, diretta e indiretta; considerazione che credo possa essere condivisa anche dagli esponenti della maggioranza, che non possono tuttavia che «turarsi il naso» e votare questa legge finanziaria, che non trova alcun riscontro nel Paese ed è fortemente criticata anche dalla Banca d'Italia. Quest'ultima ha fatto notare come sia effettivamente eccessivo il ricorso alla spesa corrente e alla leva tributaria, utilizzata più come clava che non come strumento di crescita sana e sviluppo equilibrato. In sostanza, possono riassumersi in tre gli obiettivi che si sarebbero voluti raggiungere con questa finanziaria: risanamento del bilancio, equità sociale e sviluppo economico. Di questi credo nessun possa dirsi centrato. Per quanto riguarda i conti pubblici - come detto dal Ministro dell'economia delle finanze - la crescita della spesa pubblica è iniziata nel 2000 con il Governo di centro-sinistra. Come risulta anche dallo scritto della Commissione europea, presieduta dal professor Prodi, l'Italia è stato il primo grande Paese europeo con un *deficit* eccessivo, certificato al 3,2 per cento nel 2001. Questa è l'eredità lasciata dal Governo di centro-sinistra al Governo Berlusconi. Nel 2002 è arrivata la grande crisi economica europea e mondiale che ha colpito anche i bilanci pubblici e il rapporto spesa pubblica-PIL non è salito perché aumentava la spesa pubblica quando scendeva il PIL. Nonostante questo, il 2006 si è chiuso più che in linea con i parametri fissati dall'Unione Europea, non certo per merito del vostro intervento di luglio che ha inciso solo per lo 0,1 per cento, bensì per il certificato effetto positivo delle maggiori entrate fiscali fatte registrare proprio grazie alla politica strutturale messa in campo dal precedente Governo, i cui effetti positivi cominciano a dispiegarsi in tutta la loro consistenza: maggiori entrate fiscali di quest'anno pari a 34 miliardi di euro fino al mese di novembre. Questa è la dote sulla quale voi oggi potete contare! La verità di fondo è che questa vostra finanziaria non introduce nuove misure strutturali, mentre, di contro, si affanna a smontare quelle introdotte dal Governo Berlusconi. Circa la presunta ricerca dell'equità sociale, le misure che sono state adottate e delle quali vi assumete la responsabilità politica sono di fatto poco incidenti sui redditi alti, pesanti sui redditi medi e massacranti per i redditi più deboli, che vengono tartassati da più di 60 nuove forme di tributi, tasse e balzelli. Maggiorazioni dei bolli auto sulle utilitarie, più *tickets* sulle ricette, più IVA sui riscaldamenti, poi arriverà la tassazione delle rendite catastali, BOT, aumento dell'ICI. Questa la vostra finanziaria, questa la vostra equità, tesa a rendere sempre più poveri e deboli i più sfortunati e a garantire sacche di privilegio ad alcune categorie. Togliete i soldi ai cittadini italiani per utilizzarli per i vostri fini, per aumentare il vostro potere politico di intermediazione. Basti pensare che solo un terzo dell'entità della manovra serve per sanare i conti pubblici. Certo questa finanziaria un merito indubbio lo ha: ha fatto scendere in piazza, tutte le categorie di lavoratori, ed anche la stessa maggioranza è scesa in piazza per manifestare contro sé stessa. Gli unici che brillano per la loro assenza sono i sindacati, che dovrebbero tutelare gli interessi dei lavoratori ed invece si confermano cinghia di trasmissione della sinistra e portatori dei suoi interessi. Mi chiedo come si sarebbero comportati gli stessi sindacati se oggi questa manovra fosse

una operazione di sollievo a vantaggio delle classi più povere sarebbe stato sufficiente aumentare il minimo imponibile e diminuire l'aliquota sui redditi più bassi, una operazione chiara e semplice che magari avrebbe evitato ai vostri *leader* qualche contestazione nelle fabbriche e nelle piazze. Cari colleghi, in conclusione, permettetemi di ricordare che uno dei principi fondamentali del bilancio è la veridicità. In questa manovra abbiamo assistito a tutto e al contrario di tutto. Questo Governo ha agito con recitazioni, enunciazioni, presentazioni e smentite, errori, mistificazioni, tabelle presentate e poi ritirate sotto la pressione di questo o quel gruppo di potere o portatore di interessi particolari. PRESIDENTE. Senatore, bisogna che concluda, perché i tempi sono tempi per tutti, mi spiace. FAZZONE *(FI)*. Questa Questa che vi accingete a votare è una manovra di 35 miliardi di euro, che smentisce nei fatti quanto programmato nel vostro DPEF. E', in sostanza, una manovra contraddittoria che non fa il bene del Paese e della quale vi assumete tutta la responsabilità dinnanzi ai cittadini italiani. *(Applausi

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, signori rappresentanti del Governo, esprimo un giudizio critico sulla finanziaria, un giudizio che non ha nulla a che vedere con quanto abbiamo sentito avanzare in questa sede e nel Paese dai rappresentanti della destra; una critica da sinistra che prova invece a interpretare le preoccupazioni di una parte della società, compresi i lavoratori e le lavoratrici di Mirafiori. Quella parte della società che ha sostenuto lo schieramento dell'Unione e che vuole un profondo cambio di indirizzo rispetto al precedente Governo, una rottura decisa con le politiche economiche liberiste che hanno determinato un disagio sociale sempre più ampio e lo stesso declino economico del Paese. Il mio assenso alla fiducia richiesta dal Governo è quindi correlata alle decisioni del mio Gruppo e del partito Se dovessi dare un titolo alle speranze e alle attese del mondo del lavoro, userei la parola risarcimento, parola che è risuonata fortemente in tutta la campagna elettorale e che viene ripresa quotidianamente sui luoghi di lavoro. Risarcimento sul terreno del salario, del lavoro, dei diritti; misure che permettano consistenti recuperi del reddito disponibile, radicali interventi sul terreno della precarietà, rinnovate e recuperate garanzie previdenziali, nuovi diritti sui luoghi di lavoro. Purtroppo, la finanziaria risponde solo in minima parte a queste attese. La manovra contiene infatti al suo interno alcuni parziali elementi positivi - guarda caso proprio quelli contestati dagli esponenti della destra - cioè una nuova curva delle aliquote e un più forte contrasto all'evasione fiscale, ma ogni lavoratore e ogni lavoratrice si interroga se i vantaggi che otterrà dall'intervento sull'IRPEF non saranno poi vanificati dai cospicui tagli operati sul terreno degli enti locali, dall'aumento dei contributi e dall'imposizione indiretta. Così come di fronte alle misure positive parziali sul terreno della regolarizzazione dell'enorme esercito dei precari, *in primis* quelli degli enti pubblici, ci si interroga sui ritardi del Governo a predisporre un organico intervento su tutta la legislazione che ha reso precarie milioni di persone, un enorme esercito di lavoratrici e lavoratori, pubblici e privati, sottopagati e sfruttati, impossibilitati dalla loro condizione a programmare il futuro. Registro poi che una delle proposte fiscali più importanti, quella dell'aliquota del 20 per cento sulle rendite finanziarie, si è persa per strada nella finanziaria; vedremo se sarà recuperata, come spero, con un disegno di legge ordinaria. E ancora: i lavoratori, molti lavoratori, si interrogano sul trasferimento del TFR (vale quasi un sesto delle risorse della finanziaria), sul suo utilizzo, sull'anticipo della legge Maroni e sul mantenimento dell'inaccettabile norma del silenzio assenso, sul fatto che viene loro negata la possibilità di utilizzare il TFR per migliorare la loro pensione pubblica. pubblica. Mi chiedo per parte mia quale sarà il saldo finale tra i 2,2 miliardi posti per l'intervento sociale e i contemporanei tagli per 4,4 miliardi operati sugli enti locali che sono quasi sempre i gestori dei servizi sociali stessi. Prendo atto

constatare con dispiacere e rammarico che non si è voluto costituire, come pure suggerito dalla Commissione lavoro, un fondo iniziale, pur contenuto, per le vittime dell'amianto, come impegno per un intervento legislativo più ampio e complesso per affrontare una calamità che coinvolgerà il Paese per molti anni. In realtà, la finanziaria interviene soprattutto a favore di quei soggetti sociali rappresentati da Montezemolo, cioè gli imprenditori, la borghesia, quelli che, senza dare l'impressione di alzare la voce, facendo quasi la parte delle vittime, hanno imposto con estrema determinazione e lucidità di classe i loro interessi. Quanto avranno infatti le imprese dalla riduzione del cuneo fiscale, dalle compensazioni per il trasferimento del TFR e da molti altri provvedimenti presenti euro, o forse più, a regime; una cifra enorme, che modifica ancora in senso negativo la distribuzione del valore aggiunto prodotto nelle aziende a vantaggio degli imprenditori: quella distribuzione era al 35 per cento nel 1990, poi ha continuato a crescere e oggi si attesta intorno al 46 per cento, quale trasferimento di ricchezza. Secondo quanto ci viene detto, queste risorse saranno a disposizione delle aziende per lo sviluppo del Paese. C'è per lo meno da essere prudenti su questa affermazione: quante sono le risorse date negli ultimi vent'anni alle aziende a fini di sviluppo e occupazione che invece sono diventate ristrutturazioni, speculazioni, precarietà e scarsa innovazione? Allo stesso modo è ingiustificabile che mentre si taglia la spesa pubblica di 12 o più miliardi, le spese militari aumentino di 2 miliardi, superando la soglia dei 20 miliardi complessivi. Qualcuno, se ha il coraggio, provi a spiegarlo nei luoghi di lavoro e nei mercati, nelle scuole, nei paesi grandi e piccoli. La finanziaria resta così prigioniera della logica liberista che ha, come nuove tavole della legge, il Trattato di Maastricht e il Patto di stabilità, che già hanno combinato troppi guai. Per concludere, signor Presidente, voglio aggiungere ancora un elemento: le lavoratrici e i lavoratori sono soprattutto preoccupati per la «fase 2»: nuovi tagli, innalzamento dell'età pensionabile, ennesima controriforma delle pensioni. pensioni. Se il Governo vuole rispondere alle attese del Paese, non volti lo sguardo verso la Confindustria, che ha già avuto troppo; dia un segno diverso alla cosiddetta fase 2, ne rovesci la logica e i contenuti liberisti avanzati in queste settimane.

ci sono alcuni argomenti, legati all'ambito sanitario e della ricerca scientifica, che sono stati inseriti nel maxiemendamento della legge finanziaria per il prossimo anno e che hanno recepito le esigenze di innovazione e di cambiamento che il Paese sollecita da anni: ultimamente con richieste sempre più insistenti e, a mio avviso, davvero legittime. Faccio riferimento in particolare al settore della ricerca in campo medico ed ai criteri di assegnazione dei finanziamenti ai nostri ricercatori più giovani L'obiettivo a cui puntare è quello di rinnovare il settore della ricerca partendo dal metodo di selezione dei ricercatori e dell'attribuzione dei fondi basandolo su criteri esclusivamente meritocratici, sulla trasparenza e sulla reale originalità e potenzialità dei progetti. Non solo: dobbiamo favorire i progetti dei ricercatori più giovani che devono essere giudicati in maniera rigorosa attraverso il sistema della valutazione tra pari. Per questo il Governo si è dimostrato sensibile nel sostenere una proposta avanzata qui al Senato per far sì che almeno il 5 per cento - ripeto il 5 per cento - dei finanziamenti per la ricerca in medicina siano riservati ai ricercatori al di sotto dei quarant'anni. E' infatti proprio prima di quell'età che le persone che si occupano di scienza esprimono le loro migliori idee e la maggiore capacità di produzione scientifica. Del resto, non è un segreto che anche Albert Einstein abbia condotto le sue ricerche più innovative prima dei trentacinque anni e quindi, se vogliamo puntare sull'innovazione, è inevitabile indirizzarsi verso i più giovani. La norma che è stata accolta dal Governo prevede, inoltre, che la valutazione dei progetti di ricerca sia affidata ad una commissione composta da ricercatori anch'essi sotto i quarant'anni, di cui almeno la metà operanti in enti di ricerca non italiani. Questi sono criteri riconosciuti e adottati a livello internazionale e per la prima volta vengono introdotti anche nel sistema pubblico italiano. Peraltro sono i criteri invocati anche dagli stessi ricercatori italiani, che noi politici abbiamo il dovere di ascoltare e sostenere, anche per cercare di invertire la tendenza all'esodo che da troppi anni svuota il nostro Paese di risorse preziosissime. Un secondo punto a mio avviso molto importante che è stato recepito dal Governo, e che va sottolineato, riguarda l'esclusività del rapporto di lavoro per i vertici amministrativi e scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e la conseguente incompatibilità con altre attività professionali svolte sia in ambito pubblico che privato. Personalmente sono convinto, e mi fa piacere che anche il Governo la pensi allo stesso modo, che un direttore di un istituto che si occupa sia di assistenza ai malati ma anche di portare avanti innovativi progetti di ricerca, di attrarre fondi pubblici e privati, di produrre brevetti che siano vantaggiosi anche economicamente, non possa avere il tempo e la concentrazione per dedicare una parte della sua giornata ad attività diverse. Del resto, la regola dell'esclusività è scontata e prevista per qualunque carica dirigenziale di ogni azienda, per non incorrere in un inevitabile conflitto di interessi e per assicurare che l'impegno richiesto ad un professionista non vada vanificato a causa delle troppe attività che svolge, non solo all'interno della struttura che dirige ma anche al di fuori di essa. Mi preme però sottolineare come alcuni degli aspetti sociali legati all'ambito sanitario che avevamo posto all'attenzione del Governo non abbiano invece trovato risposta e mi rammarico perché non siamo riusciti in questa sede a trasmettere ai cittadini un messaggio importante di attenzione verso i più deboli. Mi riferisco in particolare ad un problema che si trascina da molti anni senza trovare una soluzione adeguata, quello relativo alle persone, tra cui i talassemici, che hanno contratto virus molto gravi, come quello dell'AIDS o dell'epatite B o C, in seguito ad una trasfusione con sangue non controllato. Questo gruppo di persone deve essere risarcito, come è già stato fatto per esempio per altri gruppi di pazienti, al fine di rispettare in tal modo l'equità e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Occorre, a mio modo di vedere, riconoscere il dovere dello Stato verso quei cittadini che, indipendentemente dalla loro volontà, sono vittime di una grave menomazione. Si tratta, al tempo stesso, di non comprimere un diritto che deve sempre e comunque essere garantito a chi ha subito proprio da parte dello Stato un danno irrimediabile per la propria salute. C'è anche da considerare che molte di queste persone moriranno per tali malattie. Infine, vorrei sottoporre alla vostra attenzione la situazione dei nostri medici specializzandi, il cui lavoro rappresenta spesso una fonte di manodopera a basso costo per il Servizio sanitario nazionale e non solo un'occasione di apprendimento e di professionalizzazione, come dovrebbe essere. Il loro inquadramento contrattuale è di tipo precario, nonostante nessuno possa ignorare il prezioso ed insostituibile apporto di questi giovani professionisti nella gestione dei reparti dei nostri ospedali e il supporto costante ai medici strutturati in tutte le funzioni di assistenza ai pazienti, talvolta coprendo anche le carenze di organico e svolgendo turni di guardia notturni e festivi, ben oltre quanto previsto dal loro contratto e dai compiti di un medico in formazione. Proprio in virtù di queste peculiarità, dell'impegno e anche delle responsabilità che gli specializzandi assumono, chiedevamo di andare incontro alle giuste rivendicazioni di questi giovani medici attraverso un adeguato trattamento previdenziale che, attualmente, risulta inadeguato rispetto a quanto dovuto. Purtroppo, la nostra richiesta non è stata accettata. Confido, tuttavia, che il problema non venga messo in disparte e che si senta l'esigenza di trovare, al più presto, l'occasione per affrontare in maniera complessiva il nodo della situazione contrattuale dei nostri specialisti di domani. Dopotutto, essi sono i professionisti che dovranno garantire la continuità e l'eccellenza del nostro Servizio sanitario nazionale. Per queste ragioni, ribadendo il mio sostegno all'azione di Governo ritengo necessario non accantonare questi temi ma imprimere, piuttosto, una significativa accelerazione, con una più determinata attenzione, alle tematiche degli investimenti nel campo della ricerca e della solidarietà sociale. Proprio in merito a questi specifici obiettivi, mi auguro che in futuro sia confermata una necessaria e più adeguata riflessione nella nostra attività parlamentare e in quella di Governo.

otto minuti. Interverrò per fare tre osservazioni. La prima recupera in pieno l'intelligente provocazione del senatore Morando, al quale va tutta la mia stima e il mio rispetto nel riconoscimento dell'attività svolta con grande correttezza e con grande

approvando il 30 settembre di quest'anno un testo di finanziaria poi modificato tante, troppe volte. Signor Presidente, all'avvio dei lavori della Commissione bilancio del Senato

preferendolo al confronto serrato, costruttivo e concreto sui singoli temi che avrebbero potuto vederci ancora più protagonisti di quanto finora siamo stati. Prendiamo atto di ciò e sforziamoci di immaginare al più presto rimedi a questa patologia che va assolutamente superata. Da dove cominciare? Il senatore Morando ha fatto proposte convincenti. Partiamo da qui: se l'Italia è ancora una Repubblica parlamentare, e il Parlamento è il centro dell'organizzazione politica e istituzionale del nostro Paese, occorre potenziare i suoi poteri, specie quelli che riguardano le strumentazioni a disposizione di Commissioni strategiche quale è la Commissione la Commissione bilancio. In questa direzione, la proposta di unificare i Servizi bilancio di Camera e Senato va nella direzione giusta. Cito un fatto per recuperare un dato storico, signor Presidente: nel 1997, il senatore Lorenzo Forcieri, presidente del Collegio dei Questori, con il sottoscritto e con la senatrice Manieri, all'interno del progetto di riforma dell'organizzazione del Senato, fece questa proposta

soprattutto, e le organizzazioni sindacali della Camera impedirono di fatto che si accedesse a questo risultato che oggi avrebbe potuto mettere in condizione le Commissioni bilancio di Camera e Senato di avere un'organizzazione più pronta allo scopo di cui stiamo parlando.

Nel Congresso americano c'è un unico Ufficio studi che è a disposizione di maggioranza e opposizione, di Camera e di Senato. C'è però un piccolo particolare: nel 1998 nell'Ufficio studi del Senato americano lavoravano 280 economisti; noi al Senato abbiamo sette funzionari economisti (perché di recente ne abbiamo recuperato uno). In Banca d'Italia - il professor Sartor, di cui abbiamo apprezzato la professionalità

Presidente, perché siamo contro questa finanziaria? Il motivo è molto semplice: questa finanziaria propone una ricetta strutturalmente sbagliata. Chi conosce il mio Paese, gli economisti che studiano la storia di questo Paese sanno che l'economia dell'Italia in questo momento è assimilabile all'economia che avevamo all'indomani della Seconda guerra mondiale. Il congiunto operare del rapido progresso tecnologico e la globalizzazione hanno creato, come dice Schumpeter, un processo di distruzione creatrice: non siamo più competitivi. Non siamo più competitivi perché il costo per unità di prodotto non tiene il passo con i Paesi più evoluti, soffriamo la competitività dei Paesi avanzati che hanno il dominio delle tecnologie e dei Paesi poveri il cui costo del lavoro è assolutamente più competitivo del nostro. Negli anni Negli anni Novanta abbiamo realizzato l'equilibrio dei conti economici praticando una ricetta sbagliata: aumentando la pressione fiscale. Questa situazione ha formalmente soddisfatto le esigenze dei sacerdoti di Bruxelles che ci hanno in qualche modo convinto dell'ideologia dei parametri di Maastricht, però non è servita ai bisogni del nostro Paese. Non è servita ai bisogni dell'Italia perché l'Italia, oltre al riequilibrio monetario e formale, ha a che fare con due situazioni che sono tipiche del nostro Paese e non di altri: la frammentazione dell'apparato produttivo e il fatto che il tessuto connettivo non è formato dai grandi imprenditori; quelli sono grandi prenditori, non imprenditori.

La pressione fiscale grava ovviamente in gran parte sull'economia regolare e non su quella sommersa. In questo contesto, immaginare una finanziaria che aumenta la pressione fiscale e la spesa pubblica è esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un Governo che ha a cuore le sorti del Paese. Non entro nelle tecnicalità, non mi interessano i 1.400 commi di cui è composto il maxiemendamento proposto ieri dal Governo, ma far passare il messaggio che nel 2006, in un Paese come l'Italia, la cui realtà storico-produttiva è quella a cui ho fatto riferimento, la ricetta sbagliata è aumentare la pressione fiscale e avere più risorse perché si aumenta la spesa pubblica. Noi dovevamo contenere la spesa pubblica e la pressione fiscale, esercizio assai difficile al quale tanti hanno provato ad esercitarsi senza molto successo. Ancora trenta secondi, signor Presidente, devo fornire alcune risposte

Presidente, intervengo nel dibattito per esprimere il mio disagio di neosenatore nel prendere atto della quasi inutilità del mio ruolo di parlamentare

In questo contesto credo di non essere solo, anche altri parlamentari provano un forte disagio. Questa pessima finanziaria è parte essenziale del mio disagio. Pensata male e scritta peggio, è stata fin dalla sua prima stesura incomprensibile e particolarmente punitiva per il lavoro autonomo, per le imprese, per gli stessi lavoratori che hanno protestato e contestato i loro *leader* sindacali. Finanziaria complessa, invasiva, impossibile da attuare. Dal giorno di presentazione alla Camera dei deputati è iniziato il saliscendi continuo dei nuovi e vecchi balzelli fiscali. Componenti del Governo e rappresentanti dei partiti di questa attuale maggioranza hanno anticipato tantissimi emendamenti inerenti sostanziali modifiche di leggi esistenti che poco hanno a che vedere con la finanziaria. La pantomima è stata sotto gli occhi di tutti e ha provocato tantissime proteste e manifestazioni di cui quella di piazza San Giovanni ha presentato solo una parziale sintesi. Rimarco il mio disagio: il Senato non è messo in condizione di svolgere il proprio compito, di discutere seriamente tale importante provvedimento. Ho apprezzato ieri in Aula gli interventi dei colleghi Salvi, Manzione e Boccia quando hanno stigmatizzato il comportamento del Governo che, prima di fornire copia del testo del maxiemendamento fiduciario, lo ha di certo trasmesso via *e-mail* al «Corriere della Sera», vista la sua quasi istantanea pubblicazione sul sito di questo giornale. Tutto ciò è gravissimo, ma lo accettiamo passivamente, poiché viviamo nel nostro bel Paese, ove tutti i giorni leggiamo sui quotidiani le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed il contenuto di delicate e riservate indagini della magistratura

pur apprezzando competenza e capacità dei componenti la Commissione bilancio - *in primis* del presidente Morando - giudico poco serio l'esame avvenuto oggi (anzi, stamattina), in meno di due ore, di un provvedimento composto da 1.365 commi, stampato in 358 pagine (senza considerare la relazione tecnica). riconosciamo - rinunciamo a frenare una deriva che diventa inarrestabile e ci squalifica, non solo nel panorama europeo. Il Governo Prodi ha esautorato il Senato dei propri diritti-doveri ed ha annullato il ruolo dei senatori. Mi domando se accettare tale tempistica ed accogliere - com'è avvenuto stamattina - errori (materiali e non) un atto di responsabilità da parte nostra, da parte dell'opposizione. Verrà capito dal Paese, questo atteggiamento? Esprimo qualche dubbio, anche perché non ho mai considerato l'esercizio provvisorio

Parlamento). Prodi è allo sbando: nella sua ultima comparsa al Senato gli donai una bussola, solo per ritrovare l'orientamento; non l'ha utilizzata. Colleghi, vi partecipo un dubbio: per consentirci ferie anticipate, nel rispetto dei cenoni dei colleghi deputati, non stiamo perdendo - anche noi - l'orientamento? *(Applausi Signor Presidente, colleghi, voglio svolgere il mio breve intervento sul tema della sanità, che abbiamo ampiamente

L'altra grande bugia riguarda l'iniziativa di questo provvedimento, volto a reinserire il *ticket* nel pronto soccorso.

perché 96 miliardi di euro sono una cifra che oggettivamente non si può dire non sia superiore a quelle stanziate negli anni precedenti: lo è, anche in maniera consistente, anche perché lo avete fatto pure per gli anni 2008 e 2009, dando alle Regioni una

di frenare la crescita del costo della sanità che, negli ultimi anni, è stata del 7 per cento all'anno, come sarà ancora quest'anno, nonostante siano cambiate molte giunte da centro-destra e centro-sinistra, e nonostante ci sia un Governo di centro-sinistra. Mi sembra, dai dati che ho e che verifico, che la spesa sanitaria sia comunque in incremento costante. Per questo avete preso un provvedimento che avevamo fatto noi, il 3 marzo del 2005, e cioè la delibera che riprendeva il concetto,

Questi soldi sono un debito e, se sono un debito, chi lo pagherà? Su quali conti lo metterà l'attuale Governo? Soprattutto non dimentichiamo che ai cittadini che pagano 10 euro in più sui *tickets* della diagnostica, che pagano 25 euro se che pagano 25 euro se vanno al pronto soccorso, dovremo aggiungere le aliquote IRPEF e IRAP che alcune Regioni dovranno inserire per coprire il disavanzo sanitario.

naturalmente ci sono dei soldi in più, e questo è un bene; un Governo come il vostro, che ha sempre dichiarato, in ogni occasione, di essere chiaramente molto più bravo, molto più capace - sto pensando alla fase due che avete annunciato

fatele e vedrete che anche l'opposizione vi asseconderà.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci siamo occupati più volte di questa infausta, fallimentare finanziaria, in più occasioni e in vari interventi abbiamo sempre sottolineato la sua iniquità fiscale e la sua quasi inutilità rispetto al rilancio economico del Paese che addirittura ha fatto, invece, un notevole passo indietro. non lo diciamo solo noi, come attesta proprio oggi la più accreditata agenzia di *rating*, la Standard & Poor's, che ha confermato ancora una volta la veridicità delle nostre osservazioni. Questa finanziaria, ripeto, non solo ci ha fatto fare un passo indietro, ma ha vanificato e reso ancora più inutili tutti gli sforzi fatti dal Governo Berlusconi nella passata legislatura. Come riportato anche da autorevoli organi di stampa, proprio di oggi, ci troviamo di fronte alla finanziaria dei fischi e alla finanziaria che non piace neppure allo stesso *Premier*, il quale è stato ostaggio nella sua coalizione di più parti politiche contrapposte tra loro. Dicevo che la stessa agenzia Standard & Poor's boccia tutta la manovra perché non contiene nessuna riforma efficace. Non solo, per l'agenzia di *rating* la politica dell'Esecutivo in tema di riforme strutturali è assolutamente inadeguata, mentre le misure previste non produrranno una robusta e coerente riduzione del debito, il che significa, signor Presidente, che gli italiani sono chiamati a sostenere pesanti, pesantissimi sacrifici, ma assolutamente inutilmente. Mi piace precisare altresì che già ad ottobre l'Italia aveva subito il declassamento da AA ad A+ e il Governo, invece di correre ai ripari, ha continuato pervicacemente nella sua marcia infausta contro i cittadini e contro l'economia del Paese. Il risultato? Anche nel 2007 resteremo ultimi nella crescita dei grandi Paesi europei. Il ritardo rispetto alla Spagna

Ma la bocciatura della Standard & Poor's è solo l'inizio; tra poco seguirà la bocciatura di tutti gli altri italiani quando si renderanno veramente conto che, nelle loro tasche, dei loro guadagni non rimarrà più niente.

credevamo che su questa manovra di bilancio fosse stato detto tutto il peggio possibile e, invece, di giorno in giorno, se non di ora in ora, si aggiunge sempre qualcosa di più. Già alla Camera abbiamo assistito alla completa esautorazione della Commissione bilancio, prima, e dell'Assemblea, poi, rispetto all'esame dei testi del bilancio e della finanziaria, con la presentazione di una valanga di emendamenti, non dell'opposizione, ma del Governo stesso, lacerato al suo interno da mille contraddizioni e dalla presenza di posizioni ormai inconciliabili. Lo stesso spettacolo vergognoso si è ripetuto qui al Senato e, anche questa volta, per superare l'*impasse* all'interno della stessa maggioranza siete stati costretti a ricorrere al voto di fiducia. Tutto ciò è di estrema gravità perché per risolvere i conflitti interni questo Governo ha impedito il normale svolgimento dei lavori parlamentari su un provvedimento fondamentale per la vita del Paese, quale è la legge finanziaria. Non c'è stato, quindi, alcuno spazio per il dialogo con l'opposizione, di cui nessuno potrà negare il comportamento più che responsabile e tutt'altro che ostruzionistico, soprattutto in quest'Aula. Le nostre proposte migliorative, relative al sostegno alle famiglie, soprattutto quelle più numerose, all'apprendistato, ad una maggiore attenzione allo sviluppo e all'innovazione, alla piccola e media impresa, per quanto ragionevoli, non sono state prese in considerazione. Ma, al di là delle possibili misure correttive, questa manovra rimane sbagliata nel suo impianto generale. E' innanzitutto smisurata rispetto agli obiettivi di rientro del *deficit*, soprattutto alla luce del notevole incremento delle entrate fiscali. I segnali di ripresa economica, dopo anni di congiuntura negativa, andavano sostenuti con misure adeguate a favore del sistema industriale, visto anche il notevole sforzo che il Paese sta affrontando per recuperare competitività sui mercati internazionali. Al contrario, il forte incremento della pressione fiscale rischia di strangolare la fragile ripresa in corso. I piccoli e medi imprenditori vengono visti più come soggetti da vessare che come motore dell'economia. Vi è una vera e propria caccia alle streghe con una notevole complicazione degli adempimenti burocratici e un aumento abnorme delle sanzioni che rischiano di causare forti difficoltà, oltre che criminalizzare le aziende. Altro che equità di cui parla tanto questa maggioranza: la verità che questo Governo cerca di nascondere è che ci sarà un aumento indiscriminato della pressione fiscale dovuto ad una miriade di nuove imposte, molte delle quali occulte e indirette. Tutto questo graverà sulle famiglie italiane, anche su quelle meno abbienti, che andrebbero invece tutelate e aiutate con sgravi fiscali e con incentivi. Ma a quanto pare agli occhi di questo Governo ogni cittadino è guardato con sospetto e la sua unica funzione diventa quella di contribuente da cui spremere fino all'estremo senza dare niente in cambio. E gli italiani si sono resi conto di questa situazione, viste le proteste che provengono da ogni parte e da ogni categoria. Se questa finanziaria ha raggiunto un *record* è sicuramente quello di aver scontentato tutti. E mi pare che alcuni interventi della maggioranza stessa lo stiano confermando Non vi è traccia di tagli alla spesa che pure doveva essere uno dei principali obiettivi enunciati nel DPEF; infatti non si interviene neanche marginalmente sulla razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione, sul sistema pensionistico, sul sistema sanitario né sulla finanza locale. Anzi, i tagli previsti su sanità ed enti locali vengono trasferiti anche con un aumento della tassazione locale. Quindi, la manovra è basata unicamente sulle tasse. E come una manovra del genere possa essere definita equa il Governo ce lo deve proprio spiegare: più che di equità, parlerei di falso egualitarismo che in sostanza non aiuta nessuno. Non aiuta i più poveri che tali rimangono, mentre penalizza tutti gli altri indistintamente. Non è con il pregiudizio nei confronti del mondo dell'impresa e del lavoro autonomo che si risolvono i problemi del Paese, ma con politiche serie di incentivo allo sviluppo e all'innovazione. Ma anche su questo versante le scelte sono del tutto sbagliate, visto che allo sviluppo si destinano le risorse, del tutto aleatorie, drenate attraverso la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Ci chiediamo quale possa essere la ricaduta positiva in termini di crescita e sviluppo di fronte ad una situazione così indeterminata. Ma anche per le infrastrutture non c'è traccia di misure organiche e strutturali, poiché per esse si utilizzerà il fondo INPS presso cui confluirà il TFR delle imprese: ma anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione di incertezza assoluta, visto che non è prevedibile quanto del TFR alla fine arriverà all'INPS. Noi eravamo fortemente contrari a questa operazione di natura puramente contabile, che non fa altro che sottrarre risorse alle imprese senza avere effetti migliorativi sui conti pubblici, il cui unico effetto sarà ostacolare il decollo della previdenza integrativa. Non solo; non si danno incentivi dunque, ma si sottraggono risorse preziose alle imprese costringendole a ricorrere al sistema creditizio a condizioni sicuramente più onerose. Non sfuggono alla manovra punitiva neanche i lavoratori autonomi a cui vengono innalzate le aliquote contributive e vengono introdotte quelle per l'apprendistato nel settore dell'artigianato e ancora le previsioni in materia di studi di settore, che vengono inaspriti senza tener conto delle particolarità dei singoli settori: non tutti i settori produttivi godono della stessa situazione produttiva nel Paese. E si potrebbe continuare sullo stesso tenore a proposito di politica energetica, di ricerca, di scuola, di sanità. In ogni aspetto questa finanziaria non è altro che un coacervo di misure disomogenee senza un filo conduttore, laddove invece sarebbero necessarie riforme organiche da realizzare attraverso il normale *iter* parlamentare. Ma a questo Governo evidentemente non interessa il bene del Paese e questa finanziaria ne è la chiara dimostrazione: se la sua politica economica si risolve nell'introduzione di nuove tasse ci chiediamo in cosa consista il riformismo di questa maggioranza. O forse esso si risolve nel riconoscimento delle coppie di fatto, comprese quelle omosessuali? Se le cose stanno così, siamo certi che la maggioranza degli italiani non sia d'accordo con questa linea e l'UDC si è fatta portavoce di questo dissenso in Parlamento, con un'opposizione seria e determinata, fatta di argomenti concreti e di proposte alternative, e continuerà a farlo nei prossimi mesi su problemi specifici e qualificanti quali la difesa della famiglia, la flessibilità del mercato del lavoro, la riforma pensionistica, la bioetica. *(Applausi

ho sentito invece in maniera molto puntuale fatta dai miei colleghi in precedenza; cifre che ritengo siano significative del male di questa finanziaria, ma non ne siano necessariamente la causa, e sono assolutamente l'effetto di una politica economica, o meglio di una non politica economica! I tre pilastri citati nel Documento di programmazione economica e finanziaria, che poggiavano sul rigore del risanamento, su equità e sviluppo, sono stati tutti e tre obiettivi assolutamente non centrati e falliti. È fallito, per effetto dell'aumento della spesa, il primo pilastro, ce lo diceva anche l'OCSE, che ci riportava alla realtà ricordandoci che nel 2008 il rapporto*deficit-*PIL supererà il 3 Avete fallito il secondo pilastro perché, a fronte di uno sconticino di 700-800 euro nelle aliquote IRPEF sotto i 20.000 euro lordi l'anno, avete comunque costretto

Quindi, una finanziaria di più tasse e più spese. Più spese concesse ai Ministeri e più spese per i Ministri, che potranno elargire prebende agli amici degli amici, come sempre. Abbiamo dato di questo Paese un'immagine assolutamente negativa. assolutamente negativa. Siete intervenuti per 600 volte con modifiche del Governo sul testo originario della finanziaria per approdare in Aula, roba di qualche ora fa, con un maxiemendamento di circa 1.400 commi, che nemmeno 1.800 tecnici avrebbero potuto studiare attentamente in queste poche ore, figuriamoci noi poveri senatori, costretti ad arrangiarci in qualche minuto per poter dire la nostra su questo faldone.

come è stato possibile - già qualche collega lo ha sottolineato - contrarre un debito verso i lavoratori, trasferendo il TFR, e facendolo passare in questa finanziaria come nuove entrate? Ancora non sono riuscito a sentire una sola volta una risposta a tale quesito. Poi, qualcuno si è posto il problema dell'incostituzionalità, del fatto che questo elemento di bilancio nelle aziende non è un debito; è ascritto nelle poste di bilancio come fondo e non come debito contratto, quindi un debito a maturare, il quale probabilmente non può essere prelevato dalle aziende? Credo che in questo caso occorra fare qualche riflessione in più. Dico poi che non riesco a capire perché nelle tabelle che vengono date dai Ministeri si acclara che dei 33-34 miliardi di nuove entrate di quest'anno forse sono poi effetto della buona politica economica del Governo Berlusconi, piuttosto che di questo Governo), di questa somma, di cui 25 miliardi sono assolutamente strutturali perché non provengono da *una tantum*, perché nelle tabelle di quest'anno, facendo un falso in bilancio, se ne appostano solo 5? Abbiamo detto che avete fatto un sconticino di 700-800 euro a quel ceto medio - io dico ceto povero - che guadagna al di sotto dei 20.000 euro lordi l'anno, togliendo 700-800 euro; gli avete aumentato il bollo, avete indotto tasse in aumento sui rifiuti, ICI ed acqua, avete raddoppiato l'IVA sul riscaldamento, avete messo il *ticket* sul pronto soccorso e sui farmaci: che sconto gli avete fatto? Avete tolto da una parte e avete rimesso dall'altra in quantità superiori. Visco con il suo fisco ideologico si è accanito prepotentemente contro imprese e lavoratori autonomi, con un sistema di deducibilità e di retroattività da far rabbrividire. concludere, Presidente, il più rapidamente possibile. L'esercizio della retroattività è piaciuto così tanto a Visco che addirittura in questo maxiemendamento lo ha esercitato per la tassa sulle successioni; come a dire che chi è morto prima del 31 dicembre - perché il provvedimento è del 6 ottobre, se non sbaglio - lo ha fatto per sfuggire alle tasse: mi sembra che siamo al grottesco e al ridicolo. Io credo che tutti i monitoraggi, i vincoli messi alle imprese, tutto quello che è oggi, rappresenta un appesantimento per la possibilità di sviluppo. I veri pilastri di questa finanziaria sono il dilettantismo, la visione ideologica del fisco e l'ala sinistra di questa maggioranza, di cui è prigioniera la maggioranza stessa, che ha fatto di tutto per arrivare a una finanziaria che crea recessione e non sviluppo, che non tassa ma tartassa e che sarà la tomba politica di questo centro-sinistra. avevamo auspicato una discussione sulla finanziaria capace di intervenire sui punti critici e di modificarli nel segno della giustizia sociale. Per quel che riguarda la sanità e l'introduzione di nuovi *tickets*, registriamo punti di avanzamento in una discussione che ha dato un primo ascolto alle preoccupazioni di soggetti sociali e ai segnali di disagio espressi dai territori. La contrarietà all'introduzione di nuovi *tickets*, pur avanzata da subito dalle organizzazioni sindacali e ribadita nel parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria della Commissione igiene e sanità del Senato, aveva visto all'inizio della discussione la solitudine di Rifondazione Comunista tra le forze politiche dell'Unione. Senza enfatizzare i risultati raggiunti, nella consapevolezza delle criticità rimaste come delle questioni di fondo che il passaggio della finanziaria consegna all'agenda politica in tema di diritto alla salute e di precarietà del lavoro nel Servizio sanitario nazionale, tuttavia, nel dibattito pubblico è apparso chiaro come la contrarietà ai *tickets* fosse ampia a livello di massa. Non è in grado di produrre mobilitazioni, forse, presa di parola di soggetti collettivi organizzati (anche in ragione del fatto che le associazioni di promozione sociale per le malattie croniche e per le condizioni di invalidità hanno già ottenuto esenzioni per i loro assistiti e che queste sono state estese nella stessa finanziaria), ma certamente una percezione di iniquità, un disagio diffuso. Le modifiche introdotte mandano un primo segnale positivo, rompono l'effetto distorsivo prodotto dall'introduzione dei *tickets*, per cui una finanziaria che complessivamente aumenta le risorse alla sanità di 11 miliardi di euro tra spesa corrente e investimenti, in particolare a favore del Sud, veniva vissuta come una finanziaria di tagli sulla sanità. Non lo è, in netta discontinuità con le politiche del Governo precedente. Due sono i punti significativi: il primo riguarda l'eliminazione dell'obbligo per le Regioni di mettere i *tickets* sui farmaci, nel caso in cui abbiano superato il tetto del 13 di spesa farmaceutica convenzionata, pur essendo in condizioni di equilibrio di bilancio: una misura che avrebbe colpito lavoratrici, lavoratori, pensionati e pensionate e che è stata eliminata. Il secondo riguarda l'eliminazione dei *tickets* sul pronto soccorso per i cosiddetti codici verdi, che avrebbero rappresentato un elemento di iniquità privo di ogni giustificazione. Resta aperta la questione dei «codici bianchi» presenti in dodici Regioni (ma non sempre riscossi): continuiamo a ritenere che vadano tolti, almeno fino a quando l'organizzazione della sanità territoriale non abbia messo a disposizione strutture alternative a cui rivolgersi. Questa è l'unica misura che può ridurre gli accessi al pronto soccorso. È pur vero - ne prendiamo atto - che si tratta di un misura temporanea. Così come resta aperto l'aumento dei *tickets* sulle prestazioni diagnostiche, che andrà monitorato sul piano dell'equità sociale e degli effetti indotti nel rapporto tra pubblico e privato in sanità. Vorrei ricordare al collega Ghigo che i *tickets* per le prestazioni diagnostiche si attestano sui valori che la Regione Lombardia pratica da anni: lo dico perché un uso strumentale delle posizioni politiche non può essere fatto in un'Aula come questa e in una discussione sulla legge finanziaria. altro elemento positivo è il riconoscimento dell'autonomia regionale per praticare esenzioni di categorie di soggetti o di attività economiche sulle addizionali IRAP e IRPEF. È vero che restano escluse le Regioni con *deficit* nella sanità vero che questo tema andrà affrontato nella necessaria riforma dell'imposizione locale e regionale. Certo è che se ragioniamo sul *deficit* della Regione Lazio dobbiamo anche sapere che si tratta di un'eredità pesante che l'attuale Giunta Marrazzo ha ricevuto dalla precedente Giunta Storace. Così come andranno affrontate le questioni che sono state sottolineate dal senatore Marino, cui rinvio per ragioni di tempo; questioni tutte che il Governo Berlusconi ci ha consegnato irrisolte. Resta aperto il tema, che pur viene affrontato, della qualificazione e della ricerca pubblica in sanità. Siamo all'ultimo atto della discussione; certo la politica sanitaria non può essere ridotta alla finanziaria; per questo dovremo assumere subito un'iniziativa politica che valorizzi le cose positive presenti nel Patto per la salute, che affronti anche i nodi irrisolti e che forse la finanziaria non poteva risolvere. Che valorizzi le risorse in più stanziate per la sanità che sono molte - con la consapevolezza, certo, che esse non coprono la crescita della spesa tendenziale e che la spesa pubblica italiana per la sanità resta inferiore, ancora oggi, alla media dell'Unione Europea. Che costruisca criteri oggettivi per stimare la crescita nel fabbisogno di risorse in sanità e del fabbisogno pubblico di risorse in sanità e, al tempo stesso, metta a tema interventi strutturali di riduzione degli sprechi che, tuttavia, che, tuttavia, non riducano il servizio e non aumentino la partecipazione diretta alla spesa sanitaria. Che rimettano in discussione l'aziendalizzazione, le remunerazioni a prestazione e l'esternalizzazione a ribasso del costo del lavoro, la carenza di personale infermieristico. Che diano seguito agli interventi di controllo dell'accreditamento delle strutture private, affrontando altri capitoli, come la spesa farmaceutica e la riduzione delle posizioni di privilegio di cui gode in Italia questo settore, senza che ad essa corrisponda più ricerca e più lavoro. Che rilanci il carattere universalistico del sistema sanitario nazionale e del suo finanziamento per andare, oltre alla finanziaria, a realizzare quell'alternativa nella politica economica sociale che è nella attese delle donne e degli uomini che hanno votato per l'Unione garantendo il passaggio dal Governo Berlusconi a questo Governo e soprattutto Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, interverrò su un tema specifico, ma molto rilevante che riguarda il disegno di legge finanziaria per il 2007, e cioè quello relativo al sistema delle Regioni e delle autonomie locali. Dico subito che per quanto riguarda le Regioni la novità più importante e più rilevante è il Patto per la salute. per la salute. Finalmente vengono stabilite su un piano poliennale certezze per la spesa sanitaria delle Regioni, che sarà trattato più ampiamente dagli interventi degli altri miei colleghi che si soffermeranno particolarmente su questo aspetto. Per quanto riguarda il tema degli Enti locali ricorderete come la proposta di finanziaria, approvata dal Consiglio dei ministri il 30 settembre, fu criticata da parte delle rappresentanze delle autonomie e poi si pervenne il 10 ottobre ad un'intesa. ad un'intesa. Grazie a quello che è stato fatto alla Camera, ma soprattutto a quello che abbiamo fatto al Senato, si è riusciti finalmente a dare pienezza di attuazione a quella intesa, almeno per quanto riguarda il comparto dei Comuni, e questo lo ritengo molto importante.

L'intesa e la collaborazione istituzionale deve dunque essere un principio fondamentale della nostra azione. Ed è importante anche perché in questo modo, cioè attuando quello che era stato concordato, si riesce anche a rispondere a uno degli obiettivi che lo stesso Governo si è dato con questa legge finanziaria, cioè quello di contenere il più possibile il ricorso alla leva fiscale. Poiché

occorre alleggerire la manovra per impedire che gli enti locali siano costretti a utilizzare in modo eccessivamente diffuso questo strumento, solo e semplicemente per assicurare la gestione dei servizi esistenti.

La prima riguarda il patto di stabilità: viene superato il criterio ibrido per il suo calcolo e viene consentito ai Comuni che non hanno rispettato il patto per il 2006 di vedere abolite le sanzioni, prevedendo un segnale di attenzione

dell'articolo 1 prevede esplicitamente l'abolizione di tutte le sanzioni, mentre il comma 562 mantiene in vigore la sanzione relativa all'assunzione del personale. Penso fosse chiara la volontà non solo della maggioranza, ma di tutta la Commissione quando ha affrontato questo tema: il sottosegretario Sartor sicuramente prenderà atto in modo tale che si possa, con un prossimo provvedimento legislativo, porre rimedio ad un'incongruenza che purtroppo è contenuta nel maxi emendamento e che deve essere senz'altro corretta.

e il provvedimento organico di attuazione della norma costituzionale sul federalismo fiscale. Il terzo punto è costituito dall' abrogazione di una norma introdotta alla Camera sull'imposta di pubblicità che riduceva il gettito per i Comuni senza compensarli adeguatamente. Il quarto è rappresentato dalla maggiore possibilità di utilizzare in modo flessibile gli oneri di urbanizzazione, fino al 50 per spesa corrente, dal 50 al 75 per cento per la manutenzione ordinaria. Infine il quinto punto riguarda le norme ordinamentali, in modo particolare quelle riferite agli amministratori locali

positivo e ci deve aiutare a creare un clima nuovo anche nel rapporto tra Governo, Parlamento e autonomie locali e regionali. Il 2007, ed è l'ultima cosa che voglio dire, dovrà essere davvero l'anno dell'attuazione

legge finanziaria per il 2008, per quanto riguarda il rapporto con gli enti locali e le Regioni, sarà certamente più semplice e meno travagliata anche per il Governo e per il sottosegretario Sartor.

Signor Presidente, colleghi senatori, la ringrazio, anche di avermi dato la parola, perché così almeno riesco a vedere i rappresentanti del Governo in faccia, dal momento che per tutto l'intervento precedente hanno voltato la schiena all'opposizione, ma credo che in questa finanziaria sia diventato un fatto normale: questo Governo non solo ha voltato la schiena all'opposizione, ma l'ha voltata, credo, all'intero Paese, se è vero, com'è vero, che anche oggi ci sono state, anche davanti al Senato, manifestazioni di protesta, scioperi contro questa finanziaria. Ricordo quando, nella scorsa legislatura, ogni qual finanziaria puntualmente presentasse il Governo di centro-destra, da parte del centro-sinistra sembrava di assistere alla replica del venditore di almanacchi di Giacomo Leopardi, quando dicevano: «Questa è una finanziaria brutta, ma quando ci saremo noi, allora sì che faremo una finanziaria condivisa, discussa con tutti, discussa con i sindacati». Ebbene, mi risulta che ieri il Presidente del Consiglio abbia detto: «Abbiamo dato troppo spazio ai sindacati », con tanti saluti alla concertazione.

Ho sostenuto molto spesso, nelle riunioni del mio Gruppo, che era inutile presentare emendamenti a questa finanziaria, perché si poteva ottenere qualche piccolo spostamento, ma questa era ed è una finanziaria inemendabile, è una finanziaria che andrebbe presa e buttata, così com'è, nel cestino e andrebbe comunque riscritta. Aveva ragione il senatore Andreotti, quando stamattina, dall'alto della sua saggezza e della sua lunga carriera parlamentare, diceva che se si andasse ad un esercizio provvisorio non sarebbe certo un dramma e non sarebbe certo l'assedio della Capitale. Ha perfettamente ragione: questa è una finanziaria che voi avete cambiato esattamente 348 esattamente 348 volte dalla sua presentazione: da settembre ad oggi questa finanziaria, tra annunci veri, annunci falsi, lavori parlamentari, è cambiata 348 volte.

e com'è capitato con questo maxiemendamento, che la maggior parte delle modifiche siano state apportate, guarda caso, all'articolo 18, che è uno degli articoli che la Commissione bilancio non è riuscita ad affrontare, con tanti saluti a quella che si diceva da parte vostra e da parte di qualche santone che siede sui banchi dei senatori a vita (e per non far nomi faccio dei cognomi: mi riferisco al sagrestano del regime, il senatore Oscar Luigi Scalfaro),

io sono un cattolico e riconosco una funzione ai sagrestani nel far funzionare la Chiesa cattolica. Quello che volevo dire - purtroppo sei minuti sono pochi, ma i tempi sono europei che il premier Prodi, in campagna elettorale, aveva detto: «Riporterò serenità agli italiani», ma credo che gli italiani in questo momento tutto abbiano meno che serenità. Basta andare in giro nelle nostre città, basta assistere a cosa sta accadendo nelle nostre città in questi che dovrebbero essere giorni di gente felice, di gente che va a comprare, di luminarie: sembra di essere a Budapest negli anni del regime comunista; tutto c'è, meno che la serenità degli italiani nei confronti di questo Governo. Questa è una finanziaria da buttare: altro che «anche i ricchi piangano»! Mi riferisco ad alcune tasse molto banali. Mi spiace non sia più presente in Aula il sottosegretario Cento, ma siamo davvero di fronte ad un esercizio di ambientalisti della domenica o di ambientalisti alla Khomeini.

Signor Presidente, cari colleghi, membri del Governo, dico subito di condividere pienamente il parere già espresso in Aula da parte di molti colleghi: disegno di legge finanziaria 2007 rappresenta, per le modalità della sua definizione e per le sue proprie caratteristiche, un vero e proprio *monstrum* legislativo. Ad esso hanno contribuito una serie di circostanze, quali il fatto che si tratta della prima legge finanziaria di questa legislatura, proposta inoltre da un Governo di sinistra-centro che si è insediato al potere dopo cinque anni di centro-destra, il fatto che le prime importanti elezioni si tengano solo fra due anni e mezzo, il fatto che la composita coalizione di Governo abbia su non poche questioni profonde divergenze di vedute, il fatto che la maggioranza esistente al Senato sia assai risicata. I seguenti sintetici elementi possono dare un'idea di questa patologica connotazione: il testo del disegno di legge, già inizialmente molto pesante (dotato di ben 202 articoli al 30 settembre), si presenta, alla conclusione della sessione di bilancio, costituito da oltre 1.350 commi, ciascuno contenente in media varie disposizioni. Molte decine di norme sono ordinamentali o riguardanti argomenti di modesto rilievo, disposizioni entrambe esplicitamente vietate dalla legge che stabilisce le modalità di realizzazione delle legge finanziaria. Nel disegno di legge vengono considerati i più svariati argomenti: non solo quelli propri della legge finanziaria, ma tanti altri relativi alle politiche del lavoro e della previdenza sociale, della sicurezza, della difesa, della salute, dello sviluppo economico, dell'energia, dell'ambiente, dell'agricoltura, della scuola, dell'università, della ricerca, dei trasporti, delle infrastrutture, dei lavori pubblici, del demanio, della giustizia, del rapporto tra Stato, Regioni e Comuni, dello sport, della cultura, del turismo, dell'immigrazione. Di fatto siamo in presenza di un contenitore legislativo *omnibus*, buono cioè per qualunque norma. In nessun altro Paese europeo la legge finanziaria annuale presenta questa caratteristica con tale estrema estensione. In particolare, nel disegno di legge risultano evidenti gli sforzi fatti dai vari Ministri per inserirvi gli elementi principali dei futuri disegni di legge di propria specifica competenza. Queste anticipazioni legislative, private come sono del necessario contesto informativo e giuridico, risultano spesso poco comprensibili e poco motivate, manifestando anche in questo il loro carattere sostanzialmente anticostituzionale. La continua e profonda azione emendativa del testo del disegno di legge finanziaria presentato alla Camera il 30 settembre, posta in essere lungo tutto l'arco della sessione di bilancio da parte del Governo, del relatore e di esponenti della maggioranza, ne ha determinato un cospicuo stravolgimento; quanto sia stata disordinata, farraginosa ed esagerata tale azione possono essere indicativi i seguenti tre esempi: relativamente alle aliquote dell'imposta IRPEF, Governo e relatore hanno presentato e fatto approvare in successione con appositi emendamenti ben undici diverse versioni, ciascuna smentente la precedente. Al Senato, in seconda lettura, gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore sono stati oltre 160; in alcuni casi le disposizioni modificano pesantemente norme di leggi dello Stato approvate solo poche settimane o pochi mesi fa. La grande varietà delle disposizioni presenti nel disegno di legge in esame, la continua loro variazione a seguito dell'azione emendativa del Governo, nonché l'enorme numero di tali disposizioni, hanno reso sempre difficile, e in alcuni casi impossibile, un esame accurato delle disposizioni del testo del disegno di legge. In particolare, a entrare in pesante sofferenza è stato il lavoro delle Commissioni bilancio di entrambe le Camere, che ovviamente non possono essere onniscienti. In sostanza, non infrequentemente il Parlamento è stato posto nella condizione di impossibilità ad assolvere con la necessaria qualità al proprio mandato costituzionale di legislatore. Alla fine, il vero legislatore risulta essere il Governo, con scarso controllo da parte del Parlamento. Un bel risultato per la coalizione di sinistra-centro, che per pagine e pagine del suo programma elettorale si è riempita la bocca di centralità del Parlamento. In termini di contenuto, il disegno di legge finanziaria in esame si caratterizza come ispirato principalmente alla ben nota politica radicale di sinistra del *tax and spending*, che non mancherà di produrre i suoi perniciosi effetti: da un lato minore sviluppo economico rispetto a quello che si sarebbe verificato a legislazione vigente, dall'altro proliferazione incontrollabile delle clientele. Gli aumenti delle imposizioni fiscali e contributive sono numerosi e importanti e determineranno, a partire dal 1° gennaio 2007, un imponente incremento delle entrate, che si aggiungerà al notevole incremento che già si registra nel 2006 a legislazione vigente. Assai blanda è invece l'azione di contenimento della spesa pubblica, anzi, nel disegno di legge sono presenti numerose disposizioni che aprono nuove modalità di spesa. Ad esempio, vengono istituiti decine e decine di fondi di spesa completamente nuovi;

senatori, la finanziaria e la legge di bilancio che stiamo esaminando rappresentano l'atto politico più rilevante di questo primo anno di legislatura. Non mi soffermerò sulle riflessioni che già altri colleghi hanno sviluppato sull'opportunità e la possibilità di rendere più leggera e flessibile la sessione di bilancio. Allo stato delle cose, sebbene questo debba e possa essere oggetto di riflessione, non possiamo non prendere atto che i provvedimenti in esame danno il segno chiaro di una tendenza, di una linea di lavoro e di Governo. Risanamento, equità e sviluppo non sono state solo le linee guida definite nel DPEF ma anche un patrimonio concreto che ha innervato questo percorso e questi provvedimenti. Penso alla centralità e al peso che nella discussione hanno avuto i comparti del sapere, le opzioni strategiche volte a costruire una vera e propria società della conoscenza. Come è noto, nel programma dell'Unione, in quel patto fondamentale con i cittadini che hanno consegnato alla nostra coalizione l'onere e l'onore del governo del Paese, del Paese, i temi della conoscenza, dell'università, della scuola e della ricerca erano centrali; erano il motore e la leva attraverso i quali rilanciare uno sviluppo solido e duraturo. Questo è un aspetto che vorremmo sottolineare: la questione della conoscenza è investimento che ha bisogno di anni per dispiegare tutte le proprie potenzialità, ma fondamentali. E ci sembra che questa consapevolezza sia evidente in questa sessione di bilancio; basti pensare alla grande questione dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione, una battaglia e un obiettivo di prima grandezza per innalzare il livello culturale e la competitività del nostro Paese. Può sembrare inusuale che un impegno riformatore di questa portata venga inserito nella legge di bilancio. Ed in effetti la sua realizzazione dovrà essere accompagnata da un esame attento e dal coinvolgimento del mondo della scuola, della cultura e di tutta la società. Tuttavia, ritengo che nel contesto in cui operiamo la scelta sia corretta ed opportuna. Questo obiettivo è infatti caratterizzante il programma dell'Unione, è atteso anche per superare la distanza che divide il nostro Paese da altri Paesi dell'Unione Europea. Con questa decisione si applica la Costituzione, si torna ad usare la definizione di obbligo scolastico anziché quella, ambigua, di diritto-dovere all'istruzione. Alla scuola viene assegnato il compito che le compete di istituzione della democrazia. Come l'istituzione della scuola media unica nel 1962 che accompagnò e fu una leva dello sviluppo economico e culturale dell'Italia, così l'innalzamento dell'obbligo scolastico è destinato ad incidere positivamente sulle generazioni future. Non riguarda solamente quel 2 per cento di quattordicenni che oggi non frequenta la scuola. Concerne tutti i ragazzi italiani che, dopo l'approvazione della finanziaria, frequenteranno la scuola fino a sedici anni e non potranno accedere al lavoro a contratto. Riguarda le famiglie, la società intera, che potrà trarre giovamento da una nuova generazione più istruita, culturalmente preparata, capace di esercitare in modo attivo il diritto di cittadinanza. L'obiettivo è dunque ambizioso; la sua applicazione richiede il coinvolgimento pieno delle forze politiche e culturali, la sua importanza deve essere avvertita dal mondo della scuola che è chiamata a rinnovarsi, ma non solo da esso. Si tratta di una opportunità concreta per cambiare il nostro sistema e colmare le lacune nell'acquisizione delle competenze di base, soprattutto quelle scientifiche, che le più recenti indagini evidenziano come carenti, ma anche per superare la staticità sociale che caratterizza il sistema scolastico italiano. Un'altra discussione che ha profondamente attraversato il nostro dibattito è quella sulla condizione di drammatica precarietà in cui sono costretti migliaia di giovani e meno giovani nel nostro Paese. Crediamo di aver dato una prima risposta proprio nei comparti strategici della conoscenza: con un piano triennale di assunzione di 150.000 insegnanti e con una soluzione certa in grado di superare l'eliminazione delle graduatorie, si dichiara, con grande nettezza, come il destino e il futuro della formazione dei nostri studenti non possa essere affidato a persone che, giorno dopo giorno, siano costrette a cercare una cattedra, senza sicurezze, senza continuità didattica. La soluzione collocata nel maxiemendamento per le graduatorie degli insegnanti è una soluzione equilibrata che saprà coniugare le necessarie certezze dei precari della scuola con la necessità di rendere più chiari e trasparenti i criteri della loro composizione. E ancora: le classi primavera, le novità sul comodato d'uso dei libri e sul noleggio, l'apertura delle scuole al pomeriggio sono passi importanti per una scuola più moderna ed efficace. Sono questi risultati che ci consentono di sostenere con convinzione questa finanziaria, nonostante essa contenga anche interventi sbagliati e criticabili, soprattutto in una fase di risanamento, come l'ennesima mancia alle scuole private o come la mobilità obbligata in altre amministrazioni per gli insegnanti inidonei. Dall'altro lato, i segnali dati per la stabilizzazione dei precari nelle università e negli enti di ricerca sono, anche in questo caso, un primo, fondamentale segnale. Rileviamo con soddisfazione come, negli enti di ricerca, grazie anche alla nostra iniziativa, si siano allargate le maglie che consentono di stabilizzare i precari della ricerca a fronte dell'uscita in pensione di operatori che lavorassero a tempo indeterminato. Bisogna essere consapevoli della drammaticità della situazione prima di parlare di assunzioni senza contratto o sanatoria: più della metà dei professori universitari nei corsi di nuova istituzione, circa 3.000 sui 5.000 esistenti, sono professori a contratto, cioè persone che dedicano cinquanta ore di lezione all'anno a fronte di meno di 2.000 euro all'anno: persone che sono costrette a fare i professori universitari per *hobby*. A questi volontari del sapere affidiamo la formazione d'eccellenza, le lauree specialistiche, i *master*. Questa è la situazione: una situazione che depaupera profondamente il nostro patrimonio intellettuale. Per quanto riguarda i ricercatori, è ancora peggio: gli investimenti presenti in questa finanziaria e lo sblocco del *turnover* dei ricercatori sono un primo passaggio, particolarmente importante e delicato. In una fase di risanamento, anche la scuola soffre di alcuni interventi di riduzione degli stanziamenti, come avviene attraverso l'aumento del numero degli studenti per classe. Speriamo che la riforma dell'Agenzia di valutazione (quell'inefficiente INVALSI che tanto abbiamo criticato), riforma contenuta anch'essa nella finanziaria, consenta nel futuro interventi maggiormente selettivi ed efficaci non possiamo che augurarci, allora, nel prosieguo della legislatura - dato che la Commissione bilancio non ha potuto valutare tutta la finanziaria ed il bilancio - che la riforma della legge n. 468 del 1978 e la revisione delle regole della sessione di bilancio divengano una priorità, priorità, che deve essere iscritta in una riforma più complessiva del lavoro parlamentare, al fine di rendere più celeri e puntuali i nostri lavori, anche rafforzando il ruolo delle Commissioni. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranieri. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dedicare il mio intervento ad una valutazione di come esce il mondo dell'università e della ricerca da questa finanziaria, da questa finanziaria, seria ed impegnativa, che aveva ed ha, come obiettivo fondamentale, il risanamento del debito,

se ne esce con qualche pesante criticità, su cui sarà necessario intervenire (se, finalmente, la politica ed il Governo italiani decideranno di fare dell'università e della ricerca il problema fondamentale che il Paese dovrà affrontare per volgersi davvero

lì vi sono risorse importanti per la ricerca, in relazione ad un progetto di innovazione, di rinnovamento e di salto in avanti qualitativo del sistema produttivo del nostro Paese. Il Il sapere nel nostro Paese soffre di due problemi: in primo luogo, se ne fa poco (abbiamo una percentuale di laureati inferiore a quella di altre Nazioni europee e un investimento pubblico in università e ricerca inferiore alla media dell'OCSE); in secondo luogo, vi è un sistema produttivo e sociale che non riesce ad utilizzare pienamente nemmeno quel sapere, del tutto insufficiente, che il nostro sistema dell'università e della ricerca produce. produce. Un intervento per innovare e innalzare la qualità del nostro sistema produttivo dei servizi, allora, è premessa e condizione fondamentale

Parlo di beni culturali, di trasporti, di nuove tecnologie dell'informatica e della comunicazione, di risparmio energetico: di settori nodali, insomma, su cui è necessario concentrare non solo attività produttiva, ma anche molta attività di ricerca;

possano aprire un'utilizzazione intelligente e sinergica delle risorse che, in questi settori, l'Europa ci mette a disposizione. Credo che non possiamo tralasciare nemmeno il fatto che il FIRST, il nuovo fondo che unifica i centri preesistenti a sostegno della ricerca, gode di 300 milioni in più per anno per tutte e tre le annualità. Quindi abbiamo un arco di progetti e di potenzialità, a disposizione del mondo dell'università e della ricerca, più ampio che nel passato e che costruiscono un collegamento più stretto che nel passato tra l'attività di ricerca, di didattica e la produzione di nuove e la produzione di nuove opportunità per lo sviluppo del Paese. Ma attenzione: credo che l'indebolimento del finanziamento ordinario all'università, che avviene con questa finanziaria, rischia di rendere problematica e difficile la stessa possibilità, per l'università, di interfacciare con i nuovi progetti che pure il decreto Bersani e il FIRST gli mettono a disposizione. Credo che esista un rischio, e cioè che si crei uno scompenso tra le risorse disponibili per la ricerca applicata allo sviluppo e la ricerca di base, quella che normalmente l'università finanzia con risorse e con progetti propri. Questo sarebbe un brutto segnale, perché l'Italia non ha bisogno semplicemente di una ricerca tesa a innovazioni incrementali, rispetto a quello che attualmente produce, ha bisogno di cambiare il proprio assetto produttivo e le proprie priorità, e, per cambiare il proprio assetto, per le innovazioni radicali, c'è bisogno di tanta ricerca di base. È quello che stanno facendo la maggior parte dei Paesi del mondo, anche quelli che in passato hanno investito di più sulla ricerca applicata, che oggi si rendono conto dell'improduttività degli investimenti in ricerca applicata se non accompagnati da analoghi investimenti sulla ricerca di base.

in maniera stringente una parte delle risorse del FIRST proprio ai progetti autonomamente presentati dalle università, a sostegno della ricerca libera «tirata» dalla curiosità e dalla voglia di innovazione dei ricercatori e delle università stesse. Comunque è indubbio che l'università e la ricerca rischiano di uscire da questa finanziaria indebolite nella loro attività normale. cosiddetto decreto taglia spese, che il decreto Bersani, sulle spese intermedie, agiscono su tutti i settori della pubblica amministrazione, ma faccio notare che questa cosa è particolarmente pesante in quei settori che sono sottofinanziati rispetto alla media europea e alla media internazionale.

tagli che devono essere rapidamente superati. Parlo di questi tagli come dei tagli al dritto allo studio. Io ritengo inaccettabile che, anche in un momento di emergenza finanziaria, si finanzi il dritto allo studio al di sotto del riconoscimento dei legittimi diritti delle persone che, per condizione di reddito, avrebbero diritto alla borsa di studio e credo che dovremo provare a recuperare prima della prossima finanziaria, usando a questo fine le risorse reperibili, se, come io credo, si aprirà con questa finanziaria una nuova fase di sviluppo del Paese. Noi, nel parere che abbiamo fornito, all'unanimità su questo punto, nella settima Commissione, avevamo anche indicato una strada da perseguire in questa direzione. Ormai è diventato un luogo comune degli ultimi dibattiti giornalistici paragonare l'università italiana a quella inglese

dobbiamo stabilire che questo non si può fare all'interno del Fondo di trasferimento ordinario così com'è. Dovremmo costruire una strategia, se possibile, capace di andare oltre questa stessa legislatura, che mantenga costante il Fondo ordinario e decidere al contempo che tutti gli incrementi del Fondo verranno assegnati all'università tramite valutazioni. Abbiamo un'occasione per discutere di questo. Nella finanziaria è annunciato il varo, da parte del Ministero dell'università, della nuova Agenzia nazionale per la valutazione. Ebbene, discuteremo, ci confronteremo - credo - in maniera unitaria su quali dovranno essere le caratteristiche di questa Agenzia ma, attenzione, se non doteremo il sistema di risorse necessarie per fare in modo che le valutazioni diventino poi premi e incentivi alle università migliori, rischiamo di creare un'Agenzia nazionale di valutazione in cui

previsto anche un bando - una novità positiva della finanziaria - per assumere 3.500 giovani ricercatori in tre anni. Credo che l'esistenza di uno stesso valutazione capace di premiare e di punire sia anche la condizione perché quelle modalità di reclutamento avvengano finalmente su base innovativa e rompano tutti gli schematismi clientelari.

che anche in questa finanziaria - mi auguravo di no - si registri una difficoltà presente per tutta l'ultima legislatura e anche in quella precedente: la difficoltà che ha la politica di investire sul futuro del Paese.

aggiungerei anche il merito per i giovani studenti e per i giovani ricercatori. Dopo tutto, questa capacità di usare i meriti e i bisogni è stata da sempre una caratteristica fondamentale dello schieramento cui appartengo.

onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, raramente una finanziaria è stata oggetto di così grande attenzione, alla stregua di un grande evento mediatico. Si tratta di un documento senz'altro importante che cerca di dare attuazione al programma di maggioranza, un treno che passa alla stazione una volta l'anno da cui ognuno vorrebbe cogliere qualche vantaggio o, perlomeno, assicurarsi che il carico di fiducia che gli ha affidato non venga intaccato. Questa finanziaria, a partire dal testo originale licenziato dal Governo, è stata oggetto di innumerevoli modifiche, ha alimentato enormi speranze, proposte avanzate dai vari Gruppi politici, dai singoli parlamentari, ognuno dei quali deve legittimamente far capire al suo elettorato che esiste, che ha fatto il possibile, che ha presentato le sue proposte. Il tutto ampiamente comunicato ai *media*. Il risultato è un testo rimaneggiato, quasi completamente ricostruito, migliorato, per alcuni, per altri peggiorato. Una finanziaria che ha avuto il merito di interessare in qualche modo tutti i cittadini, le varie organizzazioni, le associazioni, le istituzioni, una finanziaria *factotum*. Credo veramente che questo sia il punto. Con la finanziaria si affrontano, purtroppo in modo a volte superficiale, surrettizio e strumentale, temi di importanza, di spessore che meriterebbero ben altro approfondimento che un dibattito affannato che non può essere portato a termine e che culmina con la scrittura di un maxiemendamento del Governo, che recepisce senz'altro le istanze più pressanti, ma che rischia di mortificare il dibattito e lo sforzo compiuto anche dai parlamentari, siano essi di maggioranza o di opposizione. Uno strumento da riformare - credo che sia stato condiviso da tutti - nella sua struttura, nella sua leggibilità, nei suoi metodi, nel suo percorso e nei suoi contenuti. Ho apprezzato l'impegno del presidente Morando condiviso, mi pare, dalla Commissione, di avviare sin da gennaio proposte operative per migliorare questo importante strumento. Veniamo agli obiettivi. Questo documento affronta un problema importante, sostanziale e condiviso, al fine di garantire la rispettabilità del Paese: parlo della riduzione del disavanzo, del contenimento del debito pubblico, un obiettivo - credo - condiviso da tutti, che ci garantisce di stare in Europa, che ci permette di iniziare un percorso di riduzione del debito, condizione essenziale per permettere qualunque progetto per il futuro. Gli altri obiettivi annunciati, quali il rilancio dell'economia e il perseguimento di una maggiore equità sociale, senz'altro condivisibili, si prestano invece a letture diversificate, a volte contraddittorie. L'opinione pubblica è confusa, il sentimento più diffuso è comunque quello dell'insoddisfazione, insoddisfazione ampiamente alimentata dai *media*, dalle parti politiche, da tanti opinionisti; un mormorio in un clima di confusione generale con questo eco di fondo: aumento delle tasse. Altri obiettivi sono essenziali e condivisibili, quali la lotta all'evasione e all'elusione fiscale o il contenimento della spesa pubblica. Questa finanziaria ha sollevato tanti problemi, ha individuato alcuni mali endemici della nostra società, alcune roccaforti di privilegi e di *lobby*, ha tentato alcune soluzioni ed ha avuto il merito di interessare veramente l'opinione pubblica: ci sono state numerose manifestazioni, in particolare di piazza, quelle più politiche, quelle più corporative, fino all'insoddisfazione della nuova classe operaia. Queste sono la prova che essa non deve essere sottovalutata, perché il Paese ha veramente bisogno di chiarezza e di certezze. Occorrerà lavorare per dare risposte ponderate ed approfondite su temi fondamentali quali il lavoro, un equo prelievo fiscale, il grosso tema citato degli incapienti, la sicurezza, la ricerca, la scuola. Vorrei ora soffermarmi su alcuni aspetti che attengono all'organizzazione dello Stato e al rapporto con le sue articolazioni: le Regioni e le autonomie locali. Dal punto di visto istituzionale l'orientamento politico è quello di procedere nell'applicazione della riforma del Titolo V della Costituzione e quello di favorire i tavoli di confronto e di intesa più operativi, più dinamici. Sul lato della disciplina e riduzione della spesa pubblica, richiesta in modo determinato anche dall'opinione pubblica e dal mondo economico, l'orientamento è di razionalizzare le spese, tramite l'applicazione di sani princìpi federalistici, quali la sussidiarietà e la solidarietà. Ho quindi notato, con una certa preoccupazione, il tentativo di scaricare tutto sulle autonomie locali e sulle Regioni lo sfondamento dei limiti della spesa pubblica. Occorre senz'altro responsabilizzare il sistema territoriale italiano, premiando però chi gestisce meglio, ma porre però nel contempo attenzione a compensare le situazioni di debolezza e di fragilità. Una buona norma che prelude a un giusto federalismo fiscale è prima io credo quella del versamento diretto dell'addizionale IRPEF nelle casse dei Comuni. Lo Stato, *in primis*, con il suo Governo e con il Parlamento deve porsi il problema del contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica. Il sistema regionale e delle autonomie locali deve allora essere coinvolto in modo più responsabile, garantendone il ruolo, le funzioni e l'autonomia. Ho notato poi con qualche preoccupazione l'orientamento volto a sminuire il ruolo particolare delle autonomie differenziate. Cerchiamo forse di omologare il sistema regionale? Le autonomie speciali sono state riconosciute per delle ragioni ben precise, storiche, culturali, geografiche, economiche e linguistiche particolari. Le Regioni a Statuto speciale rappresentano la punta di diamante del federalismo e del regionalismo e devono perciò essere messe in condizione di tracciare il percorso verso nuove forme di assunzione di responsabilità a livello territoriale. È quindi ora di dare piena attuazione all'autonomia fiscale delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, definite da specifiche norme di attuazione, come pure è inderogabile disciplinare il coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali. La sperimentazione per l'applicazione del patto di stabilità previsto per le Regioni e le Province autonome è di buon auspicio, ma la sperimentazione deve avere un tempo celere e nuove regole dovranno al più presto essere definite da una norma di attuazione degli Statuti speciali. Non può essere accettato il concetto che le procedure per il controllo del patto siano omologate a quelle delle Regioni ordinarie; si tratta, nel caso delle speciali (è bene ricordarlo chiaramente), di un accordo, di un'intesa. Ci sono, infine, degli effetti delle norme tributarie statali che devono trovare sistemi di compensazione, poiché le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome hanno accolto la necessità di contribuire allo sforzo economico generale assumendosi alcune funzioni dello Stato da concordare, e già sopportano spese importanti, quali scuola e sanità. Essendo l'unico senatore della Regione autonoma Valle d'Aosta eletto in una circoscrizione uninominale, quindi rappresentante della Regione, voglio soffermarmi sull'impatto di questa finanziaria sullo sviluppo e sulle aspettative della Regione autonoma Valle d'Aosta. Ribadita la necessità di maggiore attenzione verso le autonomie speciali, voglio soffermarmi su alcune misure che troviamo comprese nel testo della finanziaria. Con soddisfazione ho verificato l'impegno a realizzare alcune infrastrutture importanti per la viabilità e il collegamento internazionale: parlo della sicurezza della galleria del Gran San Bernardo e del suo accesso e di un primo intervento, con l'accoglimento di un nostro emendamento, per l'ammodernamento della linea ferroviaria Torino-Chivasso-Aosta. La Valle d'Aosta è l'unica Regione d'Italia ad essere dotata di un collegamento ferroviario con le linee nazionali e internazionali assolutamente insufficiente e obsoleto, allorquando si tratta invece di una linea di interesse generale, che raggiunge la Valle, ma che attraversa una buona parte della Provincia di Torino. Un plauso al Governo per aver voluto dare questo segnale positivo e tangibile, che risponde anche ad un accordo politico dei parlamentari con il Governo Prodi e con questa maggioranza. Ricordo però che la Valle d'Aosta aspetta risposte precise circa la cessione della caserma «Testafochi», attraverso l'intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro della difesa, come previsto da apposita norma di attuazione statutaria in materia di edilizia universitaria. A seguito poi degli eventi alluvionali del 2000, dopo aver riparato i danni, credo in modo celere ed esemplare, c'è necessità di proseguire con un programma di difesa del suolo, per far fronte alle gravi fragilità idrogeologiche determinate e avviate dall'evento alluvionale dell'ottobre 2000. Esiste poi la necessità di garantire una gestione corretta del Parco nazionale del Gran Paradiso, che interessa la Regione Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, assicurando personale adeguato e iniziative soprattutto per valorizzare il territorio e l'offerta turistica. La nostra università, nata di recente, deve potersi sviluppare, rispondendo ai soli limiti al controllo previsti dall'applicazione del patto di stabilità interno alla regione. Non può essere equiparata a un'università statale. Sul piano più generale, dobbiamo rilevare un lieve miglioramento dei fondi per la montagna. Ci accingiamo a presentare un disegno di legge condiviso che potrà incidere sulla promozione e sulla valorizzazione del ruolo e delle opportunità che la montagna offre. Devo dare atto che il confronto parlamentare e la concertazione avviata dal Governo con le istituzioni e i soggetti interessati hanno determinato miglioramenti sostanziali alla finanziaria, volti a correggere misure a volte vessatorie o difficilmente comprensibili. Voglio pure sottolineare alcune misure che ne hanno migliorato l'impatto sull'intero Paese e, in particolare, su un sistema economico e sociale delicato come quello di una Regione di montagna. Cito alcuni esempi: l'alleggerimento tributario per le piccole e medie imprese; l'esenzione dal trasferimento del TFR all'INPS per le imprese con meno di cinquanta dipendenti; la riformulazione degli studi di settore; la fissazione di importanti franchigie per la tassa di successione a favore dei parenti in linea diretta e i coniugi; una misura in favore dei fratelli per il passaggio di proprietà delle imprese; un'importante agevolazione per i portatori di *handicap*; l'esenzione IVA per le piccole aziende agricole. Ancora: i finanziamenti a favore dei piccoli Comuni e delle comunità montane; la riduzione dell'IRAP; la riduzione dell'aliquota dei contributi previdenziali per gli apprendisti; e, infine, la revisione della curva IRPEF a sostegno delle famiglie con figli e il ritiro della proposta sulla tassa di soggiorno. In conclusione, credo che oggi chi ha dichiarato il proprio leale sostegno al Governo Prodi, condizionato però al rispetto di un accordo dai contenuti precisi, che prevede anzitutto un'attenzione e un atteggiamento positivo del Governo e della maggioranza verso le autonomie speciali, chiede di avviare un processo di modernizzazione d'intesa con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (come richiesto da tutti i Presidenti delle Regioni e delle autonomie speciali nella dichiarazione di Aosta del 2 dicembre 2006 in occasione di un'interessante audizione tenutasi ad Aosta con le Commissioni affari costituzionali della Camera dei Il mio giudizio politico sulla finanziaria è quindi un giudizio cauto, che accompagno ad un pressante invito per uno sforzo volto a valorizzare meglio l'apporto istituzionale del sistema delle Regioni e delle autonomie locali, ed in modo particolare delle autonomie speciali. Richiedo un impegno a considerare meglio le specificità del nostro sistema Valle d'Aosta nel suo complesso: un impegno, quindi, a dare risposte puntuali ad alcune necessità impellenti per lo sviluppo della nostra università della caserma «Testafochi») e per l'assetto della sicurezza del nostro territorio. Un impegno per la montagna, in generale, che non reclama privilegi ma la valorizzazione delle sue peculiarità e delle sue grandi potenzialità con misure adeguate e pertinenti. Il mio voto, senz'altro, sarà favorevole anche per permettere l'approvazione di questa finanziaria e dare subito le risposte ad un Paese disposto - credo - ad accettarne la sfida implicita, sperando però caldamente

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la finanziaria al nostro esame ponga una grande questione morale: il senatore Ranieri, con l'onestà intellettuale che lo caratterizza, qualche giorno fa ebbe a dichiarare su «l'Unità»

obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età». Sono le stesse identiche finalità della riforma Moratti,

a questo scopo sono destinati 220 milioni di euro, come ad altre dieci finalità. Quindi, 220 milioni di euro all'anno per ben dieci distinte finalità; 30 milioni, fra l'altro, soltanto per un investimento in infrastrutture e nuove tecnologie. Dunque, a fronte di una spesa di circa 500 milioni di euro in più, ci saranno, sì e no, 120 milioni di euro complessivi per l'assunzione di nuovi insegnanti. Con riferimento poi al discorso del precariato della scuola, si replica quanto abbiamo visto con quella autentica farsa relativa al precariato della pubblica amministrazione; i posti disponibili dal settembre 2006 al settembre 2009 sono - lo ha dichiarato chiaramente il Governo nella relazione tecnica - 116.000, da questi devono essere detratti altri 33.000 posti organico per i tagli che questa finanziaria contiene.

Il professor Parisi, fisico, consigliere del ministro Mussi, ascoltato accademico nel mondo della sinistra, aveva su «l'Unità» dichiarato, qualche giorno fa, che la diminuzione di risorse rispetto al 2006 sarebbe pari a 544 milioni di euro. Cito un tecnico molto vicino alle posizioni del Ministro. La CRUI addirittura ha stimato in quasi 1 miliardo di euro la diminuzione di risorse tra tagli e mancati adeguamenti in relazione alle nuove esigenze. che il decreto Bersani taglia 250 milioni di euro sulle spese intermedie; sono, tra l'altro, quelle risorse proprie dell'università; penalizza le università virtuose; sono le risorse che derivano dalle tasse universitarie, dai contributi delle imprese, dal frutto delle ricerche, dai brevetti; non sono quindi i trasferimenti dello Stato. Voglio ancora ricordare che questa finanziaria consolida 242 milioni di euro. Voglio ricordare che in questa finanziaria non ci sono i soldi sul fondo di finanziamento ordinario per pagare gli scatti stipendiali che, come si sa, ammontano a circa 350 milioni di euro. Lasci perdere, senatore Ranieri, lo stanziamento di 750 milioni di euro per la ricerca privata. Basti ricordare che nel decreto del luglio 2005, il precedente Governo arrivò a stanziare addirittura 1 miliardo di euro per la ricerca Al di là di questo, non c'è un disegno strategico, e ciò si deduce da molti altri aspetti. Al riguardo dobbiamo ripercorrere molto rapidamente ciò che si è fatto in questi mesi; sono stati ritirati i decreti sulla programmazione universitaria che per la prima volta operavano un minimo di razionalizzazione meritocratica, più soldi a quelle università che hanno un più adeguato rapporto FFO-spese per il personale e penalizzando appunto quelle università meno efficienti.

Siamo arrivati al paradosso di prevedere la possibilità per il Governo di sopprimere gli enti di ricerca, di modificare ampiamente la struttura degli enti di ricerca con semplice regolamento, violando la Costituzione; dopo dieci giorni il Governo ha accolto le nostre dure proteste, le proteste del mondo dell'accademia e della ricerca e ha modificato con un disegno di legge appena approvata. Non c'è in questa finanziaria nessun fondo per la valutazione; vorrei inoltre segnalare che in questa finanziaria si prevede per il 2008 addirittura un taglio sul fondo di finanziamento ordinario pari a 200 milioni di euro, pari a 200 milioni di euro, e lo sottolineo. Senatore Ranieri, come possiamo allora parlare di sviluppo, di dialogo sul futuro, quando non si finanzia la riforma della valutazione? Quando si prevede addirittura che in futuro, in prospettiva, ci saranno ulteriori tagli al sistema dell'università?

italiane e, quindi, l'università ha espulso questo Governo, ha chiesto a questo Governo di non farsi più vedere negli atenei italiani. Credo sia un fatto gravissimo, mai successo prima, su cui occorre meditare molto attentamente. Voi avete trovato persino i fondi per i gatti randagi. Scusate, lo dico con tutta la simpatia che si può provare per gli animali randagi: avete in questa finanziaria aumentato pure le risorse per questo capitolo e non siete stati capaci di trovare risorse per la ricerca e per la nostra università. Avete addirittura proposto in una prima fase di tagliare gli stipendi dei docenti universitari, causando la sollevazione del mondo della ricerca e dell'università: ricordo che furono raccolte in poche settimane oltre 4.000 firme, grazie ad alcuni professori universitari che si mobilitarono in questo senso. Allora è chiaro: avete ingannato gli italiani per fare una politica che danneggia l'Italia e che dovreste cambiare radicalmente. Mi dispiace che un galantuomo come il ministro Mussi, una persona seria, sia stato in qualche modo preso in mezzo, stritolato da contese politiche che riguardano la vostra maggioranza. Qualcuno ieri sera, quando ho denunciato questa clamorosa dell'università abbiano giocato problemi interni ai DS o forse problemi connessi al futuro Partito Democratico e ai relativi equilibri politici. Avete giocato sull'università italiana per le vostre beghe politiche: tutto questo non è accettabile.

Mi domando: che cosa ci regaleranno Prodi e il suo Governo oggi? La finanziaria che ci ha propinato ha cambiato centinaia di volte il suo volto, mandando in fibrillazione artigiani, imprenditori, pensionati, ricercatori scientifici, anche i ragazzi del «Motor Show» di Bologna, che hanno espresso con vivacità la loro protesta contro l'aumento delle tasse automobilistiche. Cosa ci regalerà domani,

Verrebbe da ridere nel sentire queste affermazioni, ma bisogna ricordarsi che nel frattempo i problemi restano e sono gravi. Non mi scandalizzo perché sia stata messa la fiducia sulla finanziaria, ma mi scandalizzo perché stanno difendendo una manovra che è errata nel suo insieme e che non sta in piedi. Prodi e il suo Esecutivo stanno confondendo il pedale del freno con quello dell'acceleratore, convinti come sono che la loro azione muoverà l'economia e ridistribuirà risorse nel Paese. Non lo dicono i sondaggi de «La Padania», di «Libero», de «Il Giornale», lo dicono i sondaggi dei fogli vicini a questo Governo che gli italiani ormai sono arrivati all'esasperazione e non riescono più a sopportare la saccenza di chi si presenta come il sommo depositario della scienza e della conoscenza economica. Non si riuscirà mai a capire il senso delle loro azioni, o meglio, ci si rende conto sempre di più che si è sviluppato all'interno della maggioranza e dell' Esecutivo un vero e proprio mercato delle vacche, una vergogna! E che dire dell'atto di ruberia, nei confronti di coloro che hanno depositato i loro soldi in banca, per sistemare i precari? Che cosa vuol dire il fatto che si sono dimenticati di questi soldi? Uno può fare la scelta di aprire un conto corrente e non movimentarlo mai. Chi ha detto che la gente si è dimenticata di questi soldi? Allo stato attuale la disciplina dei depositi cosiddetti è contenuta nel codice civile all'articolo 586, con una procedura che si applica in ogni caso a tutte le eredità giacenti. E poi, signor Presidente (e le parla uno che in banca ha vissuto per alcuni decenni): gli istituti di credito ben si guardano dall'investigare su chi è il legittimo titolare di quei conti o chi sono i possibili legittimi suoi eredi; alla banca interessa solamente, anzi preferisce, avere a disposizione quelle somme sulle quali impunemente lucrare. Questa azione illegale fa il paio con quanto è successo con l'altro atto di ruberia attuato dal Governo Amato nel luglio del 1992, quando si prelevò il 6 per mille dai risparmi degli italiani. E poi, la sistemazione dei cosiddetti precari è a vita? Dovete considerarne Dovete considerarne bensì il costo durante la loro attività lavorativa, ma anche successivamente, quando saranno in pensione: quante volte pensate di poter attingere dai cosiddetti conti dormienti? Quando ne avrete esaurito l'ammontare a cosa penserete? Ai posteri l'ardua risposta o meglio a chi dopo di voi dovrà sistemare una eredità così pesante. Questa norma si affianca con quella sul TFR che avete dirottato dalla libera disponibilità delle aziende e dai lavoratori verso altri lidi, per bilanciare le vostre iniziative su fantomatiche realizzazioni infrastrutturali che invece, alla luce dei fatti, state continuamente bloccando. Il 1° aprile di quest'anno, una settimana prima delle elezioni politiche, avevo diffuso un'agenzia sull'argomento che l'ANSA aveva raccolto; così dicevo: «I furbetti dell'Unione stanno distogliendo l'attenzione di questa campagna elettorale con il pesce d'aprile della tassazione dei BOT. Ma il vero obiettivo sarà sicuramente il TFR, che fa gola alla sinistra, da sempre, già prima dello statuto dei lavoratori. Il loro vero obiettivo è mantenere le mani ben salde sul TFR dei lavoratori, perché questo è il vero *business* su cui la sinistra ha scelto di investire. Migliaia di milioni di euro a disposizione su cui mettere le mani». Disgrazia nostra, questa profezia si è avverata! Ma veniamo a un altro punto di questa scellerata finanziaria: è stata introdotta l'estensione per i cittadini extracomunitari delle detrazioni per carichi di famiglia per tutti i loro parenti a carico e residenti nei Paesi di origine. Non so se vi rendiate conto di quale enorme esborso comporterà questa norma, ma la si capisce dall'intento populista dell'intera manovra. Non era il caso forse di dare un'occhiata a quello che succede anche nel resto d'Europa? O dobbiamo, anche da questo punto di vista, essere i primi della classe magari dimenticandosi di soccorrere maggiormente i nostri anziani in difficoltà? In Francia, per riconoscere *benefit* ai familiari di lavoratori extracomunitari la condizione è che questi siano residenti nel Paese da un periodo minimo di qualche anno, e mi sembra che la Francia sia considerata un Paese democratico. In Germania è previsto il riconoscimento per i familiari dei lavoratori extracomunitari se residenti nel territorio dell'Unione Europea o in Svizzera. In Germania, signor Presidente, hanno il problema di una forte comunità turca, come lei ben sa: bene, è stato fatto un accordo bilaterale per riconoscere queste agevolazioni anche nel Paese di origine ma con un importo concordato e rapportato al tenore di vita della Turchia. In ogni caso, in tutte le Nazioni europee c'è massima attenzione a non disperdere inutilmente risorse ed è posta massima attenzione nella loro elargizione. Ditemi come potrà essere efficacemente controllata da parte dei nostri uffici tributari la regolarità della documentazione prodotta. Non è che con decreto legislativo successivo venga prevista un'autocertifìcazione? Non è che con un decreto legislativo successivo si pongano sanatorie come quelle poste per tutti quegli stranieri che si sono appropriati del *bonus* bebé di mille euro a figlio? «Tanto tuonò che piovve» potrebbe intitolarsi così l'ultima parte del mio intervento. È bastata, infatti, un'intervista dal suo *buen retiro* di Buenos Aires, infarcita da un messaggio golpista, e l'Unione si è calata le braghe regalando prima 14 e ora 24 milioni di euro per gli italiani all'estero. Non sono certamente milioni che andranno a soccorrere quegli italiani all'estero in difficoltà, ma entreranno nelle tasche dei COMITES, dei CGIE, dei patronati e di certi imprenditori amici degli amici. amici. Ripeto, agli italiani all'estero «normali» non andrà una lira! Mettendo sul piatto della bilancia il suo voto determinante, è riuscito a venderlo nel migliore dei modi; abile, come lo è sempre stato, fin dagli anni '70, quando praticava i salotti buoni militari di Buenos Aires, come quando il 24 ottobre 1981 portò, come Presidente di Feditalia, «il rispettoso saluto di tutta la collettività italiana» al generale Roberto Viola, dittatore dell'Argentina. È lo stesso che nel maggio del 1982 venne a Roma, a capo di una delegazione del COMITES argentino, per convincere i nostri governanti ad appoggiare l'Argentina nella guerra delle Malvinas-Falkland. È lo stesso che, ricevuto dall'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, ricevette dallo stesso l'invito ad alzarsi e a lasciare il Quirinale. Signor Presidente, non riesco a capire come questa maggioranza possa subire ricatti portati avanti da simili personaggi che sono antitetici con l'idea di resistenza che sempre bisogna tener ben salda di fronte a qualsiasi tipo di prevaricazione dei diritti umani.

che è stata commissario europeo dei trasporti durante la nostra Presidenza nel secondo semestre del 2003. Nei cinque anni come Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ho avuto modo di conoscere, di frequentare e di apprezzare Loyola de Palacio; sento quindi il dovere di ricordare e di testimoniare quanto il suo operato sia stato determinate ed essenziale per la costruzione della politica infrastrutturale e trasportistica dell'Unione Europea e del nostro Paese. Quando, nel giugno del 2001, proposi in sede comunitaria la rivisitazione delle reti TEN e la redazione di un programma organico di infrastrutture della nuova Europa a 28 Stati, la de Palacio, nel suo ruolo di commissario ai trasporti della Unione Europea, appoggiò subito la proposta e si impegnò in prima persona a che ciò diventasse un atto compiuto. Fu lei a definire subito un gruppo di esperti ad alto livello formato, per la prima volta, non solo dai 15 Paesi, ma dai 28 Paesi. Fu lei a chiedere e ad ottenere che tale gruppo fosse coordinato da Karel Van Miert, cioè da una figura di rilevanza comunitaria incontestabile; fu lei a imporre tempi certi nella redazione del quadro programmatico (solo 12 mesi); fu lei a dare, come *input* dominanti nella redazione del programma, la difesa dell'ambiente, il rilancio della rete ferroviaria, il superamento della politica miope della realizzazione di nuovi valichi, la massima attenzione per la ottimizzazione dei processi logistici attraverso il progetto Galileo. Fu sempre lei a volere che l'intero programma venisse approvato prima della conclusione della legislatura del Parlamento europeo del 2004; fu lei che condivise pienamente la nostra proposta di supportare l'intero programma con un chiaro e misurabile volano finanziario, e fu lei che, nel semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea, venne a Napoli nel Consiglio dei ministri europei delle infrastrutture e dei trasporti e presentò ufficialmente nel luglio 2003 l'intero programma. Nel mese di aprile 2004 il Parlamento europeo approvò il programma delle infrastrutture e dei trasporti della nuova Europa, approvò cioè la rivisitazione globale delle reti TEN. Ricordo che dopo il voto mi telefonò e mi disse: «Siamo artefici di una rivoluzione copernicana utile per l'Europa, peccato che molti ancora non l'hanno capito». Ed è stata sempre la de Palacio a ricoprire il ruolo di coordinatrice di uno dei progetti chiave dell'intero programma: il Corridoio 5. Quando nel mese di aprile l'ho incontrata mi ha confidato che stava lavorando con la stessa tenacia, con la stessa caparbietà con cui aveva lavorato per l'attuazione di ciò che lei chiamava «il sistema arterioso delle infrastrutture comunitarie» e mi disse che l'Europa non poteva essere privata del Corridoio; in proposito, mi fece un esempio felice: «Senza il Corridoio 5 la Comunità sarebbe un organismo senza spina dorsale». Questa è solo una tessera del mosaico di azioni e di risultati della de Palacio. Non ho infatti ricordato il suo impegno per la sicurezza stradale, la sua condivisione ed il suo supporto ad effettuare ogni anno a Verona la Conferenza dei ministri dei trasporti, non solo europei ma dell'intero pianeta, per dibattere sul tema della sicurezza stradale e per trovare insieme le soluzioni per abbattere questo assurdo dramma, questa vergogna della umanità. Non ho ricordato l'impegno profuso per superare i momenti più critici dell'Alitalia, non ho ricordato il suo lavoro capillare per dare concretezza alle Autostrade del mare e non ho, infine, ricordato l'encomiabile lavoro portato a termine, solo otto mesi fa, nella definizione della *Wider Europe*. Loyola de Palacio era riuscita, in soli 11 mesi, coordinando 47 Paesi della Unione Europea e del bacino del Mediterraneo, a produrre uno strumento complementare, quello delle reti TEN, uno strumento uno strumento che trasforma strutturalmente il Mediterraneo e lo rende da bacino geografico a grande teatro geo-economico. Un lavoro, mi confidava spesso, utile per la pace. Potrei continuare ad elencare quanti risultati la de Palacio ha regalato all'Europa, quanto ha dato al nostro Paese; in realtà, i suoi meriti saranno compresi, apprezzati, misurati solo quando capiremo quanto, in soli pochi anni, la tenacia di una persona sia riuscita a produrre, sia riuscita a produrre, a cambiare e a costruire concretamente. Loyola de Palacio è andata via portando con sé una grande soddisfazione: ha insegnato a tutti noi che la politica del fare alberga anche in Europa; ha insegnato a tutti noi che le infrastrutture e i trasporti sono l'unica vera occasione per costruire l'integrazione comunitaria e ha gridato a tutti noi che la logica degli integralismi e delle contrapposizioni ideologiche

realizzato. Credo che sia molto giusto quello che lei ha detto, senatore Lunardi, facendo sì che il Senato italiano tributasse un omaggio di riconoscenza alla memoria della commissaria. La Presidenza si associa alle parole del senatore Lunardi e del vice ministro Pinza e, a nome di tutti, esprime il suo sentimento nei confronti della scomparsa di una figura così eminente della politica

anch'io ovviamente, a nome del Gruppo dell'UDC, mi associo ai sentimenti che sono stati testé espressi a favore di una persona che ha davvero ben rappresentato, per il suo ruolo e le sue capacità, non solo la sua Nazione ma l'intera Europa. Ritornando alle vicende un po' più meschine, potrei dire, rispetto a certi esempi molto più nobili che ci riguardano, ed entrando nel merito di una vicenda che è approfondimento di questa legge finanziaria, non posso non rilevare come sarebbero in realtà bastati molti meno soldi di quelli previsti, e ben 15 miliardi di euro, per riportare il *deficit* tendenziale del 2007 sotto il 3 per cento del PIL, rispettando così i parametri europei. Invece, la manovra economica che affannosamente il Governo Prodi cerca in questi giorni di condurre in porto, nonostante l'acclarata presa d'atto di 33 miliardi di maggiore gettito tributario, ha superato la soglia dei 40 miliardi di euro. È di una prevedibilità imbarazzante, scriveva alcune settimane fa «l'Espresso», riferendosi alla finanziaria 2007, ed aggiungeva che vi si registra una totale incapacità di porre un freno al dilagare della spesa pubblica e un'ossessionante tendenza all'aumento della pressione fiscale. Si tratta di un giudizio negativo, secco, lapidario, sicuramente non annoverabile ad una stampa ostile al Governo di centro-sinistra, che ha visto, in appena sette mesi di attività, bruciare a suon di fiaschi e di fischi e contestazioni il ridotto margine elettorale che gli aveva consentito di vincere, seppure di stretta misura, le recenti elezioni politiche. Nessuna delle condizioni di partenza (sviluppo economico, equità sociale, risanamento) può ritenersi soddisfatta, tant'è che lo stesso governatore Draghi ha comunicato, come più volte ricordato anche nella giornata odierna, che nel rapporto dell'ultimo trimestre il PIL di questo Paese ha subito un arretramento, passando dallo 0,8 per cento allo 0,3 per cento, a conferma pertanto che non è aumentando le tasse che si fa crescere lo sviluppo. Il voto di fiducia sul provvedimento, chiesto prima alla Camera ed ora al Senato, come è ormai noto è servito e serve non tanto a blindare la manovra, ma la maggioranza, condizionata affatto dal dire perché si governa quanto piuttosto dallo stare lì, perché altrimenti è consapevole di tornare a votare. Per tutta la giornata di ieri l'Aula del Senato ha inventato acrobazie lessicali, è stata costretta a parlare di nulla, per dover reggere all'inverosimile la finzione di essere nonostante tutto una Repubblica parlamentare. Già, perché all'attesa del parto del maxiemendamento (di certo non breve e tanto meno indolore) si è aggiunta la perla di un'informazione resa alle agenzie di stampa prima ancora che all'Aula del Parlamento. Il Governo, fino all'ultimo secondo impegnato ad inseguire modifiche ed aggiustamenti, ha fatto, disfatto e riscritto la manovra più volte fino a quest'ultima stesura composta di oltre 1300 commi (1365, in verità) e risultata interamente sostitutiva della manovra finanziaria originaria. Tutto ciò ha regalato al Paese incertezza ed insicurezza, alimentate non tanto dallo scandalo sul voto di fiducia (per serietà, ammettiamo di averne visti diversi in trent'anni di leggi finanziarie approvate), quanto piuttosto dal fatto che mai era accaduto nel passato che le Commissioni bilancio di Camera e Senato non fossero state in grado di completare l'esame del disegno di legge. Nella manovra non si interviene se non in modo marginale sulla riduzione della spesa pubblica: i tagli sono concentrati sul comparto della sanità e degli enti locali, i quali reagiranno con tutta evidenza al calo dei trasferimenti aumentando le imposte o, in alternativa, tagliando i servizi individuali che avvantaggiano le famiglie e le classi più deboli. Le dimensioni annunciate dei tagli superano di gran lunga quelli attuati con le finanziarie dei precedenti Governi, ivi compreso l'ultimo di centro-destra; eppure, nonostante le contestazioni dei cittadini, non sono stati visti, ad onor del vero, sindaci in mutande protestare per le vie romane. Gli aumenti previsti riguarderanno i servizi individuali, gli asili nido, le scuole materne, l'assistenza domiciliare per gli anziani, i trasporti, l'IRPEF, l'ICI, il cui aumento tra l'altro sarà determinato, in virtù del contestuale trasferimento del catasto ai Comuni previsto dalla finanziaria entro il novembre 2007, dalla moltiplicazione dell'aliquota per l'aumento delle rendite catastali. Sul comparto della sanità si è abbattuta la stessa scure di tagli e si è fondamentalmente evidenziata l'assenza di una strategia di fondo capace di affrontare e coniugare organicamente da un lato le esigenze e dall'altro il contenimento della spesa. Eppure, le premesse facevano immaginare altro, altre erano le aspettative e le attese: ma, come ben si sa, di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno. Nel recente patto per la salute si era scorta una manifesta tendenza alla disponibilità nei confronti delle Regioni, alle quali venivano in maniera fin troppo generica riconosciute risorse indipendentemente dall'accertamento di una reale volontà, da parte di quelle considerate meno virtuose, ad elaborare convincenti piani di rientro. La stessa disponibilità alla comprensione però non si è intravista nelle varie stesure della manovra, soprattutto quando si è disposta l'introduzione dei *tickets* per il pronto soccorso. Un *ticket*, ci sia consentito, più simile ad un semaforo che ad una cosa seria,

che sussiste invece ancora oggi per il codice bianco; forse sarebbe il caso di pensare ad una sorta di pregiudizio politico. Il provvedimento lascia molti dubbi sull'effettiva convenienza dell'imposizione che, così come è stato fatto notare dalle Regioni che già nel passato si erano avviate per questa strada, richiederebbe altresì più attente valutazioni da fare su riscossioni e costi previsti per la sua attivazione. Tutto ciò evidenzia non solo un esproprio delle competenze regionali: che fine ha fatto - ci domanderemmo - il Titolo V della Costituzione? E ancora, vi saranno i soliti ricorsi alla Corte costituzionale, solitamente promossi nei confronti del Governo dalle cosiddette Regioni rosse? Oppure, questa volta, le ragioni di principio si troveranno a lasciare il posto a quelle, ben più pragmatiche, delle convenienze comunque elargite? Per l'introduzione del *ticket* sul pronto soccorso si è usato, come finto pretesto, il fatto che servisse per regolare gli accessi impropri, negando, in tal misura, che, invece, colpisce tutti in maniera indiscriminata, senza, in realtà, apportare correttivi che - partendo dalla testa, anziché dalla coda - possano affrontarne le cause. Queste risiedono, ad esempio, nel tentativo di superare la lunghezza delle liste d'attesa; tra l'altro - dal venerdì al lunedì - dei medici di famiglia, il cui ruolo dovrebbe necessariamente essere rivisto, rivalutato e riconsiderato in maniera più organica, e nella cosiddetta medicina di base o di distretto. Per le prestazioni di laboratorio automatizzabili, la versione originaria prevedeva un abbattimento delle tariffe del 50 per cento: l'attuale ridimensionamento dispone uno sconto del 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche per cento per le prestazioni di laboratorio. Nonostante la correzione apportata dalla Camera dei deputati, ritengo si sia davvero ingiustamente dimenticato che i laboratori privati spesso si sostituiscono al settore pubblico nel presidiare i territori e nell'erogare servizi ritenuti economicamente non vantaggiosi; ora, in virtù di quanto disposto, vedono compromessa la loro attività per l'attuazione di questo provvedimento. Troppo bassa è ancora - nonostante la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, riconfermata dal presente provvedimento - la stima (di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni per il 2008 e il 2009) relativa al fondo per la non autosufficienza; così come non è affatto condivisibile la norma che interviene sulla materia dei dispositivi medici, per i quali si assicura, come unico criterio di scelta e valutazione, il ribasso dei prezzi, a prescindere dall'elemento qualitativo.

che ci hanno messo in guardia dal rischio di vedere compromessa non solo la stabilità delle imprese e dei livelli occupazionali, ma anche la possibilità che gli investimenti in termini di ricerca e sviluppo possano, per convenienze economiche, realizzarsi al di fuori del territorio italiano. Concludendo, la filosofia cartellonistica della sinistra rifondarola («anche i ricchi piangano») ha ispirato, forse per evocare un'indimenticata lotta di classe, la manovra finanziaria del Governo di centro-sinistra.

adottando come giudizio totalmente negativo di sintesi a questa manovra il titolo del film di Massimo Troisi «Non ci resta che piangere», sperando che, con una dose di realismo in più e qualche titolo da *telenovela* in meno, si possano affrontare meglio - per il futuro, a differenza di ora - i problemi del Paese.

Presidente, innanzi tutto anch'io mi associo, a nome del Gruppo di Forza Italia, alle parole con cui l'ex ministro Lunardi ha voluto molto opportunamente ricordare, nel giorno della sua scomparsa, il commissario Loyola de Palacio, che ho potuto conoscere bene nella mia precedente esperienza al Parlamento europeo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei minuti che mi sono concessi non entrerò nel tecnicismo delle cifre né sottolineerò tutte le singole voci di una finanziaria ormai contestata da tutti (economisti, Confindustria, società di *rating*, eccetera). I colleghi che mi hanno preceduto, infatti, hanno già sottolineato egregiamente tutto questo e penso che coloro che mi seguiranno lo faranno con altrettanta precisione. Da un'ottica più politica, invece, vorrei sottolineare che la tormentata e contraddittoria manovra finanziaria di questo Governo era abbondantemente prevedibile. Basta ricordare i risultati delle elezioni politiche, vinte, nella sostanza, dai partiti della sinistra massimalista su quella moderata e, quindi, causa dello spostamento a sinistra del baricentro della maggioranza. Se non si parte da qui, non si comprende una finanziaria con più tasse che tagli, in cui le misure per la ridistribuzione - la cosiddetta equità - prevalgono nettamente sulle misure per lo sviluppo. E non si capisce nemmeno da dove derivino alcune idee, se non dall'ideologia comunista ortodossa, che cozzano con le elementari leggi dell'economia. Ne cito due a mo' di le leggi dell'economia ci insegnano che non è possibile attuare alcuna politica di ridistribuzione in un contesto economico depresso o con indice di crescita vicino allo zero. Solo dopo fasi di forte crescita è possibile correggere la distribuzione automatica della ricchezza con misure di maggiore equità. Ma la prevalenza della sinistra ideologico-massimalista ha costretto il Governo ad adottare provvedimenti di falsa equità poiché hanno caricato il peso su tutte le categorie sociali, anche le meno abbienti. E qui si spiega la politica delle tasse. Secondo esempio: l'utopia del lavoro fisso per tutti e subito. Anche qui la sinistra massimalista ha costretto a misure assurde in una economia moderna ma ha obbedito alla sua ideologia, che esalta demagogicamente il lavoro come diritto affidato allo Stato, in una logica che esclude il merito, l'iniziativa, l'individuo come soggetto del futuro e si affida invece allo Stato, al partito, al sindacato. E tuttavia la sinistra massimalista non è contenta, poiché considera che la finanziaria non è abbastanza di sinistra, tanto da far affermare al segretario del Partito dei Comunisti Italiani, Oliviero Diliberto, che la legge finanziaria «contiene mucchi di nefandezze, molti bocconi avvelenati, difficilissimi da mandare giù» ma alla fine dovrà essere votata perché, cito testualmente: «bisogna trovare una via di mezzo fra la critica e l'appoggio in modo tale da non fare cadere il Governo». Questa situazione spiega l'andamento *stop* *and* *go* dell'*iter* della finanziaria in Parlamento che, del resto, la stampa ha, suo malgrado, dovuto registrare. Anche qui faccio degli esempi: «la Repubblica»

«La Stampa»: «L'allarme delle università: finiti i soldi». Due giorni dopo: «Più soldi all'università. Mussi: non basta». É di ieri l'altro l'annuncio del «Corriere della Sera» sulla regolarizzazione di 300.000 precari; è di ieri la smentita, non sono 300.000, sono 8.500. Il presidente Prodi, compresso da spinte e controspinte, per ora se l'è cavata stralciando e rinviando i problemi, tramite un'invenzione ingegnosa: l'avviamento di «tavoli di concertazione». Ne ricordo alcuni: tavolo sul Mezzogiorno, cabina di regia sui trasporti, tavolo per Milano, unità speciale per lo sviluppo economico di Napoli, tavolo sul terremoto Umbria-Marche, tavolo Regione Calabria, tavolo su Taranto, tavolo sul collegamento ferroviario Torino-Lione, tavolo sul Mose. tavolo sul Mose. Credo che dovremmo cercare di capire le conseguenze politiche che questa situazione comporta per il Governo, a prescindere dai sondaggi sul gradimento presso gli italiani. Non mi soffermo sull'ipocrisia del Presidente della Confindustria, il quale ora dichiara: «È con con gli ammortizzatori innovativi immaginati da Marco Biagi che va affrontato il precariato, non con l'abolizione della normativa che porta il nome del professore». Ancora: «Tutti oggi dobbiamo per prima cosa fare i conti con il mercato. Anche il centro sinistra non può ignorare i cambiamenti». *No* *comment*, salvo chiedere al Presidente se mentre faceva votare per l'Unione ne avesse mai letto il programma, chiedergli dov'era, durante i comizi elettorali di Bertinotti, Diliberto e compagni, chiedergli se ha mai conosciuto - almeno per sentito dire - la teoria economica dei partiti e dei movimenti comunisti. Ma non è Montezemolo la cosa più importante.

sconta l'allontanamento degli operai dipendenti da aziende private, quelli che avevano determinato la vittoria dell'Unione; secondariamente, è quantomeno originale il fatto che coloro che hanno fischiato Epifani, Bonanni e Angeletti che il Governo considera beneficiari della distribuzione del reddito. Forse non se ne sono ancora accorti. Infine, c'è da domandarsi se il Governo non abbia perso anche l'appoggio dei sindacati che finora, pur pur con molti distinguo, lo avevano appoggiato. Signor Presidente, probabilmente chi riceverà l'eredità di questo Governo e di questa finanziaria dovrà lavorare molto per rimediare a tutto ciò che è stato fatto e che è testimoniato dalla finanziaria.

una finanziaria di lacrime e sangue, una finanziaria con questo impatto profondo che coinvolgesse tutti gli strati sociali e che ha iniziato a dividere questo Paese? I dati che tecnicamente

al lavoro nero e all'elusione fiscale l'ha fatta il Governo Berlusconi, perché questi sono dati strutturali entrati nelle casse dello Stato), dai lavoratori autonomi, che non sono dei criminali come vengono dipinti, passando agli artigiani e ai piccoli imprenditori, fino al lavoro dipendente. Ciò significa che parte dei lavoratori precari - questa finanziaria reca

Era necessaria una finanziaria di lacrime e sangue? Noi diciamo di no. Era necessaria una finanziaria di lacrime e sangue per distribuire prebende e mantenere il consenso politico elettorale, per poter far favori agli amici degli amici e alle cooperative rosse, per creare i tavoli, per creare una sorta di nuovo assistenzialismo, una sorta di terzo Stato. E ancora: per poter magari assumere nelle agenzie

il primo di tutti gli operai, il Presidente di Confindustria, il Presidente operaio, a cui qualche regalo si è fatto. Si è tracciato un quadro delle rottamazioni. Io voglio

aumento delle rendite catastali, soprattutto nel settore agricolo, che dovrà pagare di più in un momento in cui l'agricoltura versa in condizioni difficili. Ebbene, come faranno i Comuni, visto che il personale non si trasferisce?

solari su edifici di nuova costruzione. Casualmente sono già pronte le cooperative per ridefinire i criteri pronti per le nuove costruzioni. al comma 306: casualmente si parla di un regime preferenziale per l'edilizia residenziale convenzionata, che pagherà pochissimo di imposta ipotecaria e catastale; mentre invece per tutti gli altri sarà l'ira di Dio! Casualmente, alle nuove società immobiliari quotate

ha fatto dire ad un segretario di partito: finalmente abbiamo una banca. Sto parlando dell'impero Unipol! Ecco, questa è la questione morale che voglio sottoporre agli amici di sinistra: in questa finanziaria è previsto che saranno distribuite almeno 1.000 nuove ricevitorie per il gioco, che almeno 500.000 italiani cominceranno a dedicarsi ai nuovi giochi di abilità elettronica nel 2007. Diventeranno un milione nel 2008,

ci sono! Ma vede, Presidente, la fame di poltrone di questo Governo è immensa: il Credito sportivo è stato annullato, è partecipato al 75

E la nuova sfida sarà sulle banche popolari, sottosegretario Pinza, cui riconosco l'onestà intellettuale, perché fate sempre un grande parlare dell'Europa. Ebbene, l'altro giorno una sentenza europea ha stabilito che le banche popolari vanno bene così come sono con le quote capitarie, perché sono il frutto del lavoro e del risparmio dei nostri cari. Ebbene, lei ha subito risposto negativamente, siete pronti a fare un'altra legge per cambiare! Ma come è questo andamento a doppia velocità, per cui quando l'Europa dice che una cosa va bene e magari parla di Pacs o quant'altro, siete pronti a cedere la sovranità popolare, mentre, quando si parla di fare gli interessi di qualche famiglia, magari trasversale,

volevate salvare il possibile ed il giorno dopo l'Alitalia viene privatizzata e magari qualcuno si arricchisce? Ci volete venire a dire chi si è arricchito in questo Paese, speculando sui titoli dell'Alitalia? Ho posto questo problema ieri al ministro Padoa-Schioppa; non si è saputo niente. Vogliamo sapere chi è l'*advisor* della vendita di Alitalia, perché non vorrei che fosse qualcuno per il quale magari hanno lavorato cinque personaggi del vostro Governo che magari si continuano a fare le privatizzazioni non per gli imprenditori ma per i prenditori, quelli che prendono del pubblico per mettere nelle proprie tasche (e il pubblico siamo tutti noi). Si tratta allora, Presidente, vessatoria nei confronti di quella parte del Paese che è orgogliosa di tirare la carretta, che è orgogliosa di poter lavorare, che contribuisce non solo al benessere di questo Paese ma al benessere mondiale. Chiedo scusa, signor Presidente, per questo

Stiamo parlando di una realtà produttiva su cui voi avreste messo le mani e su cui voi state causando dei danni, basta vedere l'andamento dell'ultimo trimestre. Si è ridotta la crescita. Visco dice che tutti quei soldi arrivano perché hanno visto questo Governo; certo, dico io, appena hanno visto la faccia di Visco hanno mollato subito il portafoglio: «Pronti! Siamo pronti per scappare, andiamocene». E molti stanno scappando*,* E molti stanno scappando*,* stanno andando in Svizzera, perché non si sentono più tutelati. Provate ad andare dai commercialisti e chiedetegli come funziona per poter andare in Svizzera; c'è la coda, perché avete fatto mancare un elemento importante: il livello di fiducia nello Stato. Il tessuto produttivo di questo Paese ha già cominciato a produrre meno. Rispetto all'ultimo trimestre, il vostro Governo ha visto ridursi

allo 0,29 per cento. I vostri primi due provvedimenti ci costeranno il prossimo anno 300.000 posti di lavoro: 300.000 compagni, 300.000 posti di lavoro in meno. E allora avete voglia, potete continuare a creare il tavolino, il tavolone, l'agenzia, dare un milione di euro e creare l'Ente italiano montagna, la Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS (che ha sede, ovviamente, a Roma),

Qui stiamo parlando di lavoro fittizio, là parlavamo di lavoro vero, parlavamo di lavoro di persone che creavano ricchezza, che rendevano forte il nostro Paese. In questa finanziaria, e concludo, Presidente, oltre alla questione morale legata al gioco, c'è poi anche un'altra questione. Questa finanziaria è stata il grimaldello per scardinare l'articolo 29 della Costituzione, lo ricordavano ieri gli amici dell'UDC. Attraverso questa finanziaria e la tassa di successione (su cui, compagni, indietro tutta, perché prima la tassa di successione era una cosa nefanda, adesso avete già cambiato parzialmente idea),

proviamo a pensare alla famiglia allargata, ammettiamo la poligamia». La poligamia l'avete già sancita dal momento in cui le detrazioni IRPEF sono possibili in base allo stato di famiglia di altri Stati, per cui il cittadino dell'Algeria presenterà lo stato di famiglia, ovviamente vero, del paesello dove ha tre mogli e voi gli concedete le detrazioni. Questo principio dunque lo avete già scardinato. Ma il concetto di famiglia non si può esimere da un confronto parlamentare serio. Venite in Parlamento a gennaio, se ci riuscite, e decidete cosa volete fare da grandi, decidete cos'è la famiglia: una, due tre mogli; un uomo, due uomini, tre uomini, un gatto, tutti assieme appassionatamente.

affronterò l'argomento che mi compete, cioè la finanziaria nei settori della ricerca, dell'università e dell'istruzione da tre punti di vista: la scelta strategica, le luci e le ombre e la connessione con la vita degli uomini e delle donne che in questi luoghi studiano e lavorano. Il primo punto è l'elemento sovraordinatore ed è quello sul quale è più pesante e allarmato il nostro giudizio: questa finanziaria, nei settori delicati della ricerca, dell'università e dell'istruzione, drammaticamente rappresenta la fatica, la lentezza, la difficoltà di cambiare e procedere con un altro ritmo e con diversi paradigmi. Non si colloca, insomma, all'altezza di una risposta alla globalizzazione e alle nuove caratteristiche della società della conoscenza. La globalizzazione spinge alla dealfabetizzazione di massa e all'eccellenza elitaria, alla privatizzazione dei saperi e alla frammentazione dei sistemi educativi. Non è facile andare contro corrente, ma molte Nazioni, non solo europee, in vario modo e con diversi livelli di consapevolezza e determinazione, contrastano questi processi, investono in ricerca pubblica, potenziando il sistema universitario e ridiscutendo l'efficacia e la validità della scuola primaria e superiore. Quindi, questa finanziaria non assolve ancora in pieno all'impegno programmatico dirimente, cioè a quello, dopo una stagione neoliberista sfrenata dopo il binomio Moratti-Tremonti, di ricostruire l'idea di uno Stato che concepisce il sapere come bene comune e come diritto universale. al nostro esame ha comunque una storia, un progressivo mutare e migliorarsi, soprattutto nel campo della pubblica istruzione. Qui qualcosa si è mosso e i punti positivi sono molti, anche se parziali, isolati e non legati l'uno all'altro da un respiro unitario e coerente. Si potrebbe dire: sono piccoli passi in avanti. Indichiamo con forza il carattere negativo di alcuni provvedimenti che vengono presentati come necessari, in particolare l'innalzamento dello 0,4 per cento del numero medio degli alunni per classe e la cosiddetta clausola di salvaguardia, che derivano dal permanere nella nostra alleanza di visioni economicistiche, tese al dimagrimento dell'apparato pubblico, come se in esso tutto fosse inefficiente e improduttivo. Questa finanziaria innalza l'obbligo scolastico fino ai sedici anni nell'istruzione e, di conseguenza, porta a sedici anni l'età minima per entrare nel mondo del lavoro. È una svolta, una decisione storica, che in cinquant'anni il Parlamento italiano non è riuscito a varare, un'opportunità d'innalzamento della cultura del Paese che dovremmo maggiormente valorizzare, su cui investire energie politiche e intellettuali, coinvolgendo, nella costruzione del futuro biennio unitario, le soggettività che abitano la scuola. Significa, cioè, intervenire nell'attuale situazione per cui il 98 per cento dei ragazzi che finiscono la scuola media si iscrivono alla scuola secondaria superiore, ma solamente il 70 per cento arriva al diploma. Bisogna, insomma, costruire una scuola che istruisce ed educa e non sia sentita dagli adolescenti come una gabbia e una costrizione. Avremmo preferito un testo più chiaro, non condizionato dagli interessi immediati della formazione professionale, più nettamente contrario a qualsiasi sospetto di doppio canale, più capace di mettere fine agli accordi tra Stato e Regioni che, di fatto, hanno anticipato il carattere di classe

a risoluzione il problema dei precari docenti, purtroppo non degli ATA. È questo il segno che la politica può essere vicino alle speranze degli uomini e delle donne, praticare l'«ora e il subito». I precari della scuola hanno fatto sciopero, manifestato davanti al Parlamento e in molte piazze d'Italia. Hanno inondato la posta elettronica, non solamente della maggioranza, di comunicati e ci hanno anche narrato le loro vite. Sono uomini e donne plurilaureati, abilitati, che da anni lavorano nella scuola senza diritti pieni. A loro abbiamo restituito il mal tolto, abbiamo dato ciò che per decenni era scandalosamente negato; abbiamo fatto un atto di giustizia sociale che fa bene alla scuola e al Paese, perché diminuisce la precarietà e, dando continuità ad un insegnante che nelle sue classi lavora, lavoriamo contro la disgregazione sociale. Questo provvedimento apre simbolicamente le porte di quest'Aula alla società, è uno scatto di democrazia, rende quest'Aula meno separata e autoreferenziale. Spero che non sarà l'ultimo.

I sindaci delle grandi città, lo scorso anno, scesero platealmente in piazza contro la finanziaria Berlusconi che tagliava 1,6 miliardi di euro, 3.200 miliardi di lire, tanto per ridare valore a queste cifre che alle volte ci paiono poco significative. Questa finanziaria aggiunge un ulteriore taglio agli enti locali di 2,2 miliardi euro, 4.400 miliardi di vecchie lire. Veltroni, l'anno scorso, voleva spegnere i lampioni di Roma, quest'anno - per essere coerente - dovrebbe smontarli e rivenderseli. I Comuni dovranno ridurre i servizi o aumentare le entrate attraverso un aumento dell'ICI, addizionale IRPEF e tutte le tariffe a servizi individuali che gestiscono; di fatto un aumento mascherato, indiretto della pressione fiscale sui cittadini. I Comuni, gli enti locali in genere, in questi anni hanno in molti casi ammodernato, razionalizzato e ottimizzato i costi delle loro strutture e l'efficienza dei loro servizi. In molti casi certamente, non in tutti, ma in molti casi lo hanno fatto, non fosse altro perché hanno un rapporto diretto con i cittadini elettori, sono in prima linea rispetto alle esigenze dei cittadini. Hanno aumentato peraltro le competenze e la qualità dei servizi gestiti direttamente in ossequio al principio di sussidiarietà. Molti di voi conoscono i centri per l'impiego, *ex* uffici di collocamento, che erano impresentabili quando erano gestiti a livello centrale e che oggi in molte Città e Province, grazie alla gestione molto più vicina al territorio, sono diventati strutture di livello perlomeno europeo. Come altrettanto può essere evidenziato il trasferimento a livello locale e regionale della viabilità o della gestione del territorio dal punto di vista idrogeologico. Sempre più cose, in effetti, sono trasferite a livello locale, spesso gestite molto meglio di prima, e purtroppo sempre meno risorse. Anche in questa finanziaria si possono trovare molti esempi; un caso significativo di questo trasferimento di competenze e parallelamente riduzione di risorse è rappresentato dai commi 143-*bis* e 146; da una parte si autorizza il prefetto a stipulare convenzioni con gli Enti locali per intervenire con risorse locali sulle funzioni di polizia e, dall'altra parte, si dice che per il 2007-2008 occorrerà ridurre del 5 per cento la spesa corrente per la gestione dei presidi di polizia sul territorio ottimizzando e razionalizzando, di fatto chiudendo e riducendo il numero dei presidi sul territorio, a meno che non intervengano gli Enti locali. Vorrei solo segnalare ai colleghi parlamentari, ai colleghi senatori, qualora qualcuno lo ignorasse, che ormai poco più del 10 per cento delle risorse di parte corrente di un Comune proviene dallo Stato centrale; il resto viene prelevato direttamente sul territorio. In una situazione di questo genere, questa finanziaria si comporta come se gli enti locali fossero delle sue emanazioni dirette, fossero delle succursali rispetto alle quali s'interviene di autorità con dirigismo, con centralismo, imponendo norme, senza considerare che invece ormai c'è una forte autonomia e una dimostrazione di forte capacità - perlomeno in molte zone del Paese - di gestione efficiente ed efficace dei servizi. Questa capacità gestionale e questa autonomia finanziaria richiederebbero una legislazione rispettosa e soprattutto un'attenzione agli enti virtuosi, cosa che non si ritrova in questa finanziaria. Le richieste dell'ANCI, ragionevoli e spesso condivisibili, sono state in gran parte ignorate da questa finanziaria. L'ANCI, e dunque i Comuni, avevano richiesto di eliminare dal patto di stabilità i trasferimenti straordinari, le spese elettorali i cofinanziamenti dei contributi europei.

quando ho scoperto che il combinato disposto dei commi 1111 e 1119 stravolge completamente il quadro di riferimento nel quale, con grande difficoltà, gli enti locali in questi anni hanno cercato di costruire una politica e un sistema integrato di gestione e raccolta dei rifiuti, che ci portino ad un livello

Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli antichi iniziati sostenevano che dal caos nasce l'ordine. Non conoscevano però la finanziaria del Governo Prodi: un caos che partorisce solo disordine. Disordine istituzionale, economico e sociale, che il Paese avverte come una minaccia alla propria stabilità, coesione e voglia di futuro. Da troppi mesi, infatti - attorno al disegno di legge sul quale il Governo pone oggi la fiducia - assistiamo ad un continuo sabba infernale, con parole e numeri che si scatenano senza pudore alcuno per la verità. Producendo un'interessata confusione di sensi e di significati, funzionale allo stravolgimento della realtà, al nascondimento dell'oggetto in discussione, al disegno mistifìcatorio del Governo. Ogni tentativo di dibattito attorno alla finanziaria è sempre stato del resto travolto: dalla danza delle ore e delle cifre; da milioni di euro che cambiavano destinazione nello spazio dello stesso giorno; da promesse di finanziamenti che si rivelavano immediatamente inesistenti; da provvedimenti annunciati con gran clamore e poi subito ritirati; e da dichiarazioni che venivano smentite da altre dichiarazioni, anch'esse successivamente smentite. Per la serie: menzogne in libera uscita. Fino ad arrivare al massimo del ridicolo: alla contestazione in piazza di esponenti governativi, che pur dichiaravano di condividere e sostenere la manovra. Per non parlare, poi, delle continue trasformazioni subite dal disegno di legge finanziaria. La cui incessante metamorfosi ci ha portato, in realtà, a dover fare i conti con ben tre, successive e distinte, finanziarie. La prima, varata dal Consiglio dei ministri il 3 ottobre, per una manovra da 34 miliardi e 700 milioni di euro. La seconda, uscita dalla Camera dei deputati il 19 novembre col maxiemendamento di 812 commi, per un importo complessivo nel frattempo lievitato a 35 miliardi e 400 milioni di euro. La terza finanziaria è, infine, quella che uscirà da quest'Aula, senza però che il Senato abbia potuto, effettivamente, conoscerla, valutarla e discuterla. Perché questa è, in realtà, una finanziaria imposta dal Governo, attraverso il ricorso al voto di fiducia su di un maxiemendamentone di 1365 commi, che ribadisce sostanzialmente la prevista manovra da 35 miliardi e 700 milioni di euro. Una finanziaria «prendere o lasciare», da approvare per astratta scelta ideologica o per cieca fede politica; e che ha, di fatto, esautorato il potere del Senato a tutto favore del Governo. L'unico elemento di continuità delle tre finanziarie - oltre alla capacità di scontentare tutti (ma proprio tutti!) - è però rappresentato dal continuo ricorso alla pressione fiscale. Una pressione che deve essere, tra l'altro, calcolata sommando ai 35 miliardi e 700 milioni di euro di questa «finanziaria - tutta tasse» anche i 6 miliardi di euro già previsti dal decreto Visco-Bersani. L'operazione finanziaria (attuata dal Governo Prodi, per consentire allo Stato di mettere le mani nelle tasche dei cittadini) arriva perciò a sfiorare i 42 miliardi di euro, ossia 84.000 miliardi di vecchie lire. Mentre, lo stesso ministro Padoa-Schioppa ha ammesso, in più di un'occasione e con sconcertante cinismo, che per soddisfare Bruxelles e risanare i conti pubblici, bastava fare effettivamente una manovra di soli 15 miliardi di euro. Ed allora perché quei 20 miliardi e 700 milioni di euro in più (cui vanno sommati i 6 miliardi del Visco-Bersani)? A che servono? Alla crescita produttiva non certamente; come hanno sottolineato tutti gli organismi economici italiani ed internazionali, OCSE compreso, lamentando l'assenza di riforme e di tagli alla spesa pubblica improduttiva. Né servono ad una maggiore equità, viste le proteste di tutte le categorie sociali, compresi gli operai di Mirafiori. Ed allora, a che servono? A realizzare un'operazione di trasferimento di potere. Perché togliere soldi ai singoli e alle famiglie, alle imprese e agli enti locali, per concentrare tutte queste risorse nei Ministeri del Governo centrale, lasciandole alla discrezionalità di questi ultimi, significa modificare radicalmente l'equilibrio su cui si regge il rapporto Stato-cittadino. E' perciò in tale desiderio di puro e totale dominio della politica sulla società che va cercato il senso di questa finanziaria. Una finanziaria di potere, al servizio delle clientele del potere. Un altro elemento di continuità presente nelle tre finanziarie è dato dalla penalizzazione di quello che doveva essere il fiore all'occhiello del nuovo Governo di centro-sinistra: l'innovazione, la cultura, la ricerca, l'università e la scuola. Prendiamo i beni culturali. Qui, in finanziaria, è evidente la scelta a favore dello spettacolo, attraverso il rifinanziamento (sia pur modesto) del FUS e del cinema, ma a scapito della conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio artistico. Faccio un esempio concreto. Ho visto accolti diversi emendamenti della maggioranza che distribuiscono un po' di soldi a pioggia o istituiscono strutture o musei più o meno fantasiosi, ma ho visto bocciato un emendamento, dotato di copertura, che chiedeva di finanziare il definitivo restauro e recupero dei beni ancora danneggiati dall'alluvione di Firenze del 1966. Beni collocati presso l'Archivio, la Biblioteca nazionale e la Sovrintendenza di Firenze, ma di proprietà dello Stato. La sensazione è che il caos della finanziaria, foriero di disordini, serva comunque alla maggioranza e al Governo per meglio coprire regalie e favori. Piccoli interessi di bottega che niente hanno a vedere con una logica di programmazione. Certo, nel dibattito di questi giorni, è emersa la necessità di riformare la legge finanziaria, di ripensare questo strumento di allocazione programmata delle risorse, che è obbiettivamente imploso. Resta però il fatto che qualsiasi modello istituzionale presuppone comunque un Governo omogeneo e coerente al proprio interno. Proprio ciò che non è e non può essere il Governo Prodi. Così contraddittorio e caotico da trovare solo nella gestione e nel mantenimento del potere la propria ragion d'essere. La verità, allora, è che questa finanziaria, dove confusione programmatica e sordida manutenzione del potere si intrecciano, è semplicemente fatta ad immagine e somiglianza di questo Governo, il quale potrà forse incassare la fiducia richiesta, ma è ormai sfiduciato dalla maggioranza degli italiani che, con l'approvazione della finanziaria, avranno sicuramente una ragione in più per fischiare Prodi. *(Applausi dal Gruppo FI).* PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Fernando. Ne ha facoltà. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, perché questa finanziaria non attua il programma dell'Unione? Il programma era davvero condiviso e rappresentava un serio compromesso, un accordo di Governo tra varie posizioni e progetti socio-politici o era solo un passaggio tattico, una fase politica in cui faceva premio il prioritario e pur condivisibile obiettivo di vincere le elezioni e togliere il Governo al centro-destra? Io non so nel versante più centrista, ma per Rifondazione, i Comunisti Italiani, i Verdi e Consumatori quell'accordo era un accordo vero, un compromesso a cui si è creduto e tuttora, pur con meno entusiasmo si crede, per realizzare il massimo di giustizia sociale e di nuovo sviluppo; pur all'interno di un'alleanza strategica con forze, indubbiamente moderate, ma che con noi si sono fatte carico di realizzare quel programma nell'interesse generale del Paese. Invece, già in alcune accentuazioni durante la campagna elettorale, poi nella stessa formazione e composizione del Governo, ma ancora di più in seguito fino a questi giorni non sono certo mancate autorevolissime analisi politiche del tipo: nell'Unione c'è un blocco maggioritario riformista moderato che ha cultura ed esperienza di Governo, nonché i giusti rapporti nazionali e internazionali, per garantire una politica compatibile con gli equilibri esistenti, le altre forze hanno un ruolo ancillare e sono isolabili e sostituibili (come, non casualmente, la stampa italiana controllata dai più grossi gruppi finanziari e industriali ha sostenuto, dapprima invocando la grande coalizione, alla tedesca, e ora facendosi mallevatrice di un allargamento al centro). In verità, tale idea forza era già contenuta nelle riforme elettorali miranti a costringere le forze politiche minori a dipendere dalla magnanimità di quelle maggiori, ma di ciò discuteremo nel proseguo della legislatura. Chi sta dentro quel progetto, ma non vuole metterla giù dura e cruda, sostiene che è colpa del Governo precedente (con i rimborsi IVA e sparizione dei fondi Alta Velocità) se in finanziaria non sono previste risorse per attuare le scelte di giustizia sociale e di nuova qualità dello sviluppo contenute nel nostro programma. Da tale assunto, pur in parte vero, ma smontabile, si fa discendere un ulteriore, e ancor meno condivisibile, ritorno al vecchio "prima si risana, poi si sviluppa", che il programma dell'Unione definiva un errore delle passate esperienze di Governo. La questione della pace (con l'evidente contraddizione tra gli impegni di guerra in Afghanistan e la mancata sospensione dell'accordo militare con il Governo israeliano, a fronte dell'embargo nei confronti delle Autorità di Governo palestinesi, per tralasciare le incredibili dichiarazioni di autorevolissimi uomini di Stato e di Governo rilasciate nel corso delle cerimonie in occasione del tardivo ritiro delle nostre truppe dalla guerra irachena) ed ora questa finanziaria. In più, si profila all'orizzonte un secondo tempo che, invece di rappresentare un tardivo ritorno al programma, ci viene presentato come foriero di ulteriori liberalizzazioni e di messa in discussione del diritto costituzionale, ancorché di programma, ad una pensione dignitosa dopo una vita di lavoro. Sono elementi che pongono un serio problema a tutta l'Unione, ma in particolare alla sinistra e alla sua componente comunista. Chi finge di non vedere o non credere nei sondaggi può andare tra la gente o prestare attenzione alle prese di distanza, penso alle dichiarazioni iniziali di Epifani "questa è la mia finanziaria" e ora a quelle attuali e ai vari, e variamente espressi, distinguo che, rispetto a finanziaria e politiche di Governo, ora giungono da autorevoli *leader* e da importanti settori del centro‑sinistra. La vittoria elettorale con la sconfitta del Polo di centro-destra e di Berlusconi, che ne era e resta il vero *dominus*, aveva creato illusioni, aspettative e benevole predisposizioni anche in chi non ci aveva votato. Ce ne siamo accorti e tutti lo abbiamo ripetuto nei recenti mesi estivi, ma ora il clima è molto cambiato e recuperare la fiducia e il consenso di chi è stato deluso è ancor più difficile che acquisire nuovi consensi. consensi. Anche recentemente, molti opinionisti hanno indicato proprio nelle promesse mancate uno dei maggiori *handicap* elettorali del centro-destra. Se le cose stanno come tanti indicatori ci evidenziano, bisogna con urgenza correre ai ripari e l'unica strada possibile è aggiustare questa finanziaria nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. È possibile farlo attraverso leggi, decreti e circolari attuative, che evidenzino un ritorno allo spirito, e forse anche, se necessario, alla lettera del programma elettorale, in modo che il Paese possa cogliere e capire la direzione di marcia, l'inverarsi dell'ambizioso progetto originario. Mettiamo allora da parte il ricorso a pronunciamenti e richiami a comando del superliberista commissario europeo o dei suoi funzionari; le mire egemoniche; gli interessi di bottega e il parlare d'altro, altrimenti ci giocheremo il contatto e il contratto sociale con le nuove generazioni, con chi vive del proprio lavoro e con chi fa un'enorme fatica a guardare al presente ed ancora peggio al futuro con serenità. Possiamo e dobbiamo riprovarci, ma se non è questa la strada che insieme si decide di ripercorrere, se si pensa di potere uscire dai binari o di sganciare vagoni o di non rispettare regole basilari di pari dignità tra alleati, allora la sinistra, e ancora più chi si ritiene comunista e sente il compito di tenere aperte le vie per la positiva evoluzione della partecipazione democratica, dell'organizzazione sociale e produttiva e del rapporto uomo‑natura, non potrà continuare ad assumersi responsabilità non sue e a temporeggiare fino a quando non saremo già andati a sbattere. È una riflessione per ora latente, ma che, se le cose non cambiano, si renderà necessaria e cogente, non per un malinteso orgoglio ideologico, o ancora peggio orgoglio di partito, ma neanche solo per assolvere al sacrosanto dovere di salvare la sinistra e la sua credibilità dalla altrimenti prevedibilissima disfatta elettorale dell'Unione. C'è anche un'altra questione a cui erroneamente non prestiamo la necessaria attenzione: fonti attendibili parlano di 1.800.000 cittadini coinvolti nell'attività della malavita organizzata; tantissimi giovani non trovano lavoro o lo trovano precario; i lavoratori in età matura, espulsi dal processo produttivo; le donne non occupate; i piccoli imprenditori in difficoltà, ma anche lavoratori che, smarrita una coscienza di classe nella moderna parcellizzazione del lavoro, si vedono travolti - e da soli - di fronte a enormi difficoltà della famiglia. Pensiamo con più attenzione a quanto avviene in interi quartieri di Napoli, ma anche in altre periferie urbane e mettiamo tutto ciò in rapporto a quello che può produrre vivere queste situazioni con una difficoltà culturale a mantenere una criticità verso i disvalori del dio denaro, fuori, e a volte apertamente contro, i tanti momenti di coinvolgimento sociale, civile, politico, culturale e finanche religioso, che finora hanno aggregato, garantito socializzazione civile e tenuta viva la nostra democrazia. In questo quadro, in questa situazione, è cresciuto un moderno sottoproletariato che vive una profonda crisi e non possiamo pensare che sia attrezzato per aspettare i nostri rinvii e guardare avanti. Come è già avvenuto in Italia in passato, ed in tempi più recenti in Paesi e popoli dell'Est o del mondo arabo (molto c'è di questo dietro l'integralismo religioso) se anche a sinistra non ci saranno progetti, se la sinistra non sarà credibile, queste masse andranno a destra. Io voterò quindi questa finanziaria sbagliata, e che resta tale nonostante le parziali aperture (significative in sé, ma ininfluenti nel modificarne l'impianto) e nonostante l'accoglimento di alcuni emendamenti che ho condiviso con il Gruppo, in particolare con i Verdi, frutto del lavoro e dell'impegno di Natale Ripamonti in Commissione bilancio. Ma non darò il mio voto di fiducia, come cortesi ma pressanti sollecitazioni di vecchi e nuovi compagni, amici e colleghi hanno caldeggiato, per non far cadere Prodi o perché, come senatore ferrarese e come rappresentante del Partito dei consumatori abbiamo come si usa dire con un brutto termine - portato a casa qualcosa. Tra l'altro, non ho ancora ben capito se, quando e su quali soccorsi finanziari potranno sperare i 1.200 cooperatori che, con il fallimento della Costruttori di Argenta, hanno perso tutti i risparmi delle loro famiglie e in questi mesi sono faticosamente aiutati dal sacrificio solidale dei soci lavoratori di altre cooperative. Io darò questa fiducia, perché voglio ancora credere che si possa tentare una ripartenza dell'Unione e del suo progetto per l'Italia. Continuerò a rappresentare il Partito dei consumatori, a collaborare strettamente con l'Associazione Verdi Ambiente e Società e con l'ADUSBEF, che ho il dovere di ringraziare per avermi aiutato con la loro competenza a definire delle proposte delle proposte e delle ipotesi finanziarie e tecniche che avrebbero meritato una maggiore attenzione del Governo. Ma come diciamo a Ferrara, e forse anche altrove, "le uova sono buone anche dopo Pasqua" e quindi insisteremo, sperando in un maggior ascolto nei prossimi mesi. Quelle messe a punto sono valutazioni e proposte che abbiamo già diffuso tra precari e pensionati, che mettono al centro anche il tema dei saperi, della ricerca e dell'innovazione, ma che qui non ho il tempo di illustrare, avendo scelto di svolgere un intervento focalizzato sul tema dei difficili rapporti tra la sinistra e il riformismo debole dell'Unione. Sarei quindi grato al Presidente se potesse disporre la pubblicazione della restante Il mio voto di rinnovata fiducia nelle funzioni e nei compiti dell'Unione e del suo Governo, finché la ragione dei fatti non dimostrerà l'inutilità di tali sforzi, non mi impedisce di esprimere una profonda critica politica a questa finanziaria, né a quegli atti e decisioni che, certo non solo a mio personale avviso, sono o saranno ritenuti errori e decisioni incoerenti rispetto al programma

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione della finanziaria 2007 sotto forma di maxiemendamento vanifica il lavoro svolto dai colleghi senatori e dalle Commissioni parlamentari.

che è stato emendato decine di volte, che è scomparso e ricomparso come un fiume carsico, creando un fortissimo disagio non solo alla stragrande maggioranza dei cittadini ma anche alle Aule parlamentari che dovevano istituzionalmente esaminare ed eventualmente modificare il testo governativo. Sulla testa del Parlamento, quindi, si vuole approvare una finanziaria che è figlia dell'arroganza politica di questo Governo e del suo *premier* Romano Prodi. L'alleanza stretta che il presidente Prodi ha coltivato con la sinistra estrema del nostro Parlamento ha assunto un peso decisivo sulle principali scelte di politica interna, economica ed estera del nostro Paese. Il successo ottenuto da Rifondazione Comunista in materia di immigrazione, l'abolizione del respingimento alle frontiere, la sanatoria di fatto di oltre 300.000 clandestini attraverso l'abnorme rigonfiamento del decreto flussi, la demolizione della Bossi-Fini, stanno a testimoniare l'impronta determinante della sinistra estrema nella finanziaria 2007; e non è finita qui. Voglio solo ricordare il ridimensionamento della politica della sicurezza del nostro Paese: solo la Polizia di Stato perderà nel prossimo triennio circa 12.000 addetti, con pesanti decurtazioni sia sui rinnovi contrattuali che sulle retribuzioni. È di fronte a tale scempio politico ed istituzionale che tutti i gruppi dirigenti dell'economia, della finanza, dell'informazione, del nostro Paese, che pure avevano simpatizzato per il centro-sinistra, sono ora fortemente delusi dall'azione di Governo e cercano in ogni modo sbocchi nuovi per uscire da questo pantano le cui responsabilità ricadono esclusivamente su Prodi e sulla sua compagine governativa. E che dire del Mezzogiorno? Le fasce più deboli e meno protette della nostra società risentono fortemente dell'asfissiante pressione fiscale prevista in questa finanziaria. Manca del tutto una politica del Mezzogiorno; anzi, nelle Regioni del Sud (Calabria, Campania e Puglia), ormai, si vive in un clima di forti contrasti sociali, con una criminalità organizzata che, non adeguatamente contrastata dal Governo,

i servizi del Sud sono tutti, ormai, al collasso: i treni vengono soppressi sulle tratte ioniche; le opere pubbliche sono bloccate; la legge obiettivo approvata dal Governo Berlusconi - che aveva conferito un forte impulso all'economia del Sud - è stata completamente annullata, provocando, di fatto, un blocco delle grandi opere meridionali (compreso lo Stretto di Messina, che rappresentava l'icona della modernità del nostro Paese). I Comuni, sia di centro-destra sia di sinistra, sono all'opposizione del Governo Prodi e, pur rappresentando il primo baluardo della democrazia nel nostro Paese, vivono momenti di forte disagio istituzionale, a causa di un Governo miope, che ha perso ogni utile contatto con la realtà circostante. È per queste ragioni, egregio presidente Calderoli, che non solo non voteremo la fiducia, ma, anzi, lavoreremo assieme alla stragrande maggioranza degli Italiani per far cadere questo Governo, che può essere definito, senza tema di essere smentiti, il peggiore, il più arrogante ed il più deludente della nostra storia repubblicana.

e la sicurezza. Essa ha rappresentato un fiasco colossale: credo che nessuno di noi avrebbe immaginato, per la maggioranza, un disastro del genere.

perché sono scontenti assolutamente tutti (ed è difficile comprendere come si possano scontentare tutti). Lo stesso discorso di chi mi ha preceduto - il senatore Rossi

Ora, questa finanziaria ha scontentato tutti e, naturalmente, anche la componente degli operatori della difesa e della sicurezza, i quali, molto rispettosi delle norme e delle leggi, non hanno dimostrato in piazza:

invano: nonostante le infinite retromarce ed aggiunte di emendamenti che hanno caratterizzato questi ultimi tre mesi, infatti, per quanto riguarda la difesa e la sicurezza, poco o nulla è stato fatto.

ed il tradimento perpetrato nei confronti di questi uomini, che costituiscono uno dei pilastri istituzionali del nostro, come di tutti gli Stati del mondo.

e le nostre possibilità di incidere positivamente verso un maggiore sviluppo del nostro Paese, secondo quanto avevamo promesso. Purtuttavia, per quanto riguarda il discorso della difesa e della sicurezza, come prima preoccupazione, quella di tutelare il personale. Cioè, nonostante ci fossimo trovati in una situazione obiettivamente difficile, che abbiamo ribaltato soltanto nell'ultimo anno - perché quello che sta accadendo oggi, con l'aumento incredibile ed imprevedibile delle entrate e con uno sviluppo che si avvicina al 2 per

A differenza delle 18.000 lire, del famoso rinnovo del contratto fatto dal Governo di centro-sinistra precedente, noi abbiamo consentito un rinnovo del contratto più che dignitoso; abbiamo finanziato un riallineamento di certe carriere; abbiamo consentito la parametrazione delle varie categorie, altra esigenza fortissimamente sentita dal personale, che aveva ottenuto dai Governi precedenti solo la promessa di realizzazione, mentre noi l'abbiamo realizzata e finanziata; abbiamo stanziato 300 milioni di euro, cioè circa 600 miliardi di vecchie lire, per la realizzazione del riordino delle carriere. Questi sono i punti fondamentali

poi, nella finanziaria si riducono del 15 per cento le risorse per il reclutamento e quindi, da una parte, si prevede un aumento di impiego nelle operazioni di 2.500 uomini, dall'altra, se ne tolgono 14.000.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la posta per il riordino: noi, come ho detto, per tre anni, abbiamo fornito risorse; poi è venuto in Commissione il vice ministro Minniti dicendo che, in prospettiva, vi saranno più risorse e invece non hanno stanziato neanche una lira,

però contemporaneamente hanno ridotto l'acquisto di beni e servizi, che vuol dire 400 milioni in meno. Allora, perché continuare? I cittadini di tutti i ceti, di tutte le categorie hanno già sentenziato il fiasco. nei confronti del personale? Perché chi prevale, nell'ambito della compagine governativa, è una frangia, non molto numerosa ma determinante, che ha continuato, per tutta la sua esistenza, ad essere contraria, in opere e in prediche, nei confronti del personale delle forze armate e del personale delle forze dell'ordine: ecco perché non andranno molto lontano. *(Applausi dal Gruppo* Senatore Ramponi, lei ha cominciato a parlare alle ore 18,52 e 39; quindi, è bene che faccia rivedere l'orologio da un abile orologiaio, perché ha parlato per nove minuti. È iscritto a parlare il senatore Viceconte. Ne ha facoltà. Presidente, onorevoli colleghi, con questa finanziaria il Governo Prodi blocca in modo irreversibile il processo di infrastrutturazione organica del Paese già avviato e attivato dal Governo Berlusconi. Il Presidente del Consiglio per tenere insieme la sua variegata coalizione rosso-verde con qualche raro puntino bianco è costretto ad accettare i ricatti e i *diktat* dei vari ministri, come Pecoraro Scanio e Bianchi, Bianchi, che per loro filosofia politica devono dire sempre e comunque no ad opere pubbliche oggettivamente improcrastinabili anche contro l'interesse del nostro Paese. Ecco allora che si dice no al Ponte sullo Stretto di Messina, all'asse viario Umbria-Marche, all'asse ferroviario Torino-Lione del Corridoio 5, al valico ferroviario lungo l'asse Genova-Milano e altre ancora, solo per l'esigenza interna all'attuale Governo mirata alla tenuta della maggioranza. Il centro-sinistra ha voluto, con argomenti pretestuosi e polemiche strumentali, ridimensionare il significato positivo dei risultati ottenuti dal Governo Berlusconi. Questa legge finanziaria è una legge ingiusta che non risana i conti e non produce alcuno sviluppo del Paese. Tutti gli italiani sono colpiti negativamente da una manovra finanziaria scritta in un laboratorio intriso di tecnicismo, di propositi vendicativi, di una ingiustificata e assurda ansia livellatrice e pauperista. Ma il Paese, l'Italia ha già reagito; i due milioni di persone a Roma ne sono l'esempio lampante. Grazie al sistema di tassazione pensato e attuato dal Governo Berlusconi, il gettito derivante dai tributi è cresciuto dell'11 per cento, facendo segnare maggiori incassi per oltre 37 miliardi di euro. Il Governo Prodi non ha il coraggio di prendere atto del proprio fallimento. Oggi basterebbe una manovra intorno allo 0,8 per cento del PIL per poter rispettare i parametri di Maastricht. Il risultato di questa politica finanziaria, con l'aumento di due punti della pressione fiscale, sarà mettere in seria crisi la ripresa economica e la crescita del nostro Paese nel 2007. Il nostro Mezzogiorno, di cui tanto parla questo Governo, si trova ingiustamente privato di ben 4 miliardi di euro scippati al FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) che quando eravamo al governo del Paese con Silvio Berlusconi presidente il centro-destra aveva destinato a nuove infrastrutture e a nuove opere pubbliche. La stagione della legge obiettivo, in cui tante opere pubbliche sono state progettate, condivise con le Regioni, cantierate e alcune ultimate, è stata bloccata. È veramente assurdo che il Governo Prodi pensi di destinare solo 3,3 miliardi di euro nel triennio 2007-2009 per il rifinanziamento del programma della legge obiettivo. È inconcepibile pensare di collegare al fondo TFR i finanziamenti a favore delle Ferrovie per l'Alta velocità, per investimenti in materiale rotabile e per la rete ordinaria. Il Fondo TFR appare sempre più come una specie di artifizio contabile e, pertanto, risulta assolutamente incerto se non addirittura inammissibile, oltre che ancora soggetto al giudizio di EUROSTAT. Anche l'OCSE il 28 novembre scorso ha severamente bocciato la manovra Prodi. Un'ulteriore incapacità di questo Governo di dare risposte univoche per il rilancio del Sud è stata dimostrata sul tema dell'utilizzazione delle accise sulla benzina. Questo Esecutivo, strabico nell'azione politica, ha ritenuto opportuno riconoscere tale diritto soltanto alla Regione Sicilia che raffina il petrolio e non alla Regione Basilicata, che è il più grande produttore di petrolio del nostro Paese, riuscendo da sola a ricoprire circa il 15 per cento del fabbisogno energetico nazionale. Pur sottolineando di non aver nulla contro la Sicilia, noi contestiamo un provvedimento che discrimina i lucani trattandoli come cittadini di serie B. Vorrei rivolgere un invito alla senatrice Finocchiaro, la cui sensibilità è nota, ad indurre il Governo a rivedere questa posizione considerando che non solo la Sicilia, che comunque rimane penalizzata, ma anche la regione Basilicata, seppur piccola, fa parte del Mezzogiorno e quindi dell'Italia. Questa finanziaria non convince e non piace al Paese. Il Paese, signor Presidente del Consiglio, purtroppo per lei e per il suo Governo, vuole già voltare pagina. Le nostre famiglie non potranno sopportare la stangata che il Governo Prodi ha preparato con aumenti indiscriminati dei costi per le prestazioni sanitarie, per le tasse automobilistiche, con carichi di balzelli sul risparmio, sulle successioni, sulle donazioni e sulla casa. Economisti di livello internazionale da tempo rilevano pubblicamente che sarebbe stata sufficiente una manovra composta per circa 15 miliardi di euro. Dove saranno destinati i 25 miliardi di euro in più? Su nuove spese correnti dirette solo a sostenere macchine burocratiche inutili e costose, oltre che dannose, per soddisfare le pressanti richieste dei sindacati protetti dalla sinistra estrema e radicale che condiziona e detta legge all'interno di una maggioranza parlamentare piena di pesanti e ormai insanabili contraddizioni. Per queste ragioni esprimiamo un forte dissenso al Governo Prodi, autore di una manovra priva del necessario impulso alla crescita e alla competitività del sistema Paese. Il Paese ha bisogno di ben altro! Ha bisogno di coraggio, di fiducia e di credere in una Italia libera e forte, in cui siano stimolati i fattori dello sviluppo e ridotti i costi dello Stato nei comparti della spesa corrente. Noi parlamentari di Forza Italia rimaniamo a fianco dei cittadini di questo Paese per dare voce a chi è esasperato e deluso, per continuare a difendere quelli che vogliono il vero sviluppo nel rispetto della dignità di ogni cittadino. *(Applausi *(UDC)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, quanto sia fatta male questa finanziaria perché eccessiva, perché punitiva dei ceti medi produttivi, senza essere di aiuto e di vantaggio per i deboli, soprattutto senza una strategia, un progetto - lo hanno detto, prima ancora dei tanti colleghi dell'opposizione intervenuti, gli esponenti della sinistra. Ricordiamo le frasi di Chiamparino, di Cofferati, della presidente Bresso ed in ultimo di Amato, di Fassino, o l'intervento - che abbiamo ascoltato poco fa di un esponente della maggioranza. Lo hanno detto le contestazioni di Mirafiori, le grandi manifestazioni di Roma e di Palermo fatte dall'opposizione, ma anche quelle fatte dalla sinistra Ed è stato in quelle manifestazioni che abbiamo ascoltato gli *slogan* più duri, più difficili verso il Governo. Ne cito solo uno, che si può dire: «Un

tant'è vero che il parere votato in Commissione dalla maggioranza ha contenuto ben 12 pesanti osservazioni. La maggioranza non ha avuto il coraggio di essere conseguente e di porre almeno quelle come condizioni, ma questo ha dimostrato che, al di là del gioco delle parti, anche la maggioranza era insoddisfatta e solo alcune di queste osservazioni sono poi state accolte nel testo definitivo del maxiemendamento. Ma, al di là dei provvedimenti,

quando il presidente Prodi ha presentato i documenti finanziari aveva dichiarato con orgoglio di essere riuscito a non aumentare le tasse, a redistribuire la ricchezza, a far partire lo sviluppo; cioè il miracolo in poche parole! Ed ha mantenuto questa convinzione, nonostante le critiche mai così diffuse nel Paese, mai così tante, provenienti dai settori della sua maggioranza, nonostante i sondaggi unanimi nel rilevare il calo del consenso, i giudizi delle società di *rating*. Anzi, di fronte a queste proteste, ha affermato: «Protestano tutti; dunque vuol dire che va bene!». Una frase che ricorda quella, molto pericolosa: «Tanti nemici, tanto onore!». A chi contesta, risponde: «Voi siete strumentalizzati». Orbene, questo - a mio parere - è un atteggiamento che dimostra una forte presunzione intellettuale ed umana, prima ed ancora che politica, che se continua può trasformarsi in arroganza e che significa un pericoloso distacco dalla volontà popolare. In secondo luogo, una delle critiche più frequenti che la maggioranza passata di centro-destra si era sentita rivolgere era: «Voi non concertate!». Ricordiamo tutti le grandi disquisizioni tra concertazione e consultazione. Ebbene, queste accuse vi erano nonostante quella maggioranza avesse sottoscritto il Patto per l'Italia; nonostante quella maggioranza, per fare riforme importanti come la legge Biagi e quella sulle pensioni, avesse discusso per due o tre anni. Questa maggioranza, invece, fa il decreto Bersani-Visco all'improvviso; un decreto che tocca pesantemente le professioni o altri interventi e con lo stesso sistema fa la finanziaria. Guardate che le categorie hanno protestato con voi, prima ancora che per il merito, per il metodo con cui portate avanti i provvedimenti. Mi sembra che stia emergendo un nuovo tipo di figura di concertazione:

Terza osservazione. È vero, colleghi, che la finanziaria è sempre un provvedimento complesso e difficile ed è vero altresì che è sempre ben ascoltare, cambiare, accogliere proposte migliorative, ma in questa occasione la finanziaria è cambiata ogni giorno. Ci sono stati provvedimenti annunciati e poi ritirati, anzi provvedimenti contrari a quelli proposti,

Quanti esempi potremo fare? Quante volte abbiamo letto di *ultimatum*, di minacce, di ricatti per l'appunto da parte della maggioranza? Questo significa una cosa precisa e, ripeto, Significa che c'è una profonda e lacerante divisione all'interno della maggioranza, che finora è stata aggiustata, sono stati trovati dei compromessi in nome della sopravvivenza. Ma guardate che compromessi fatti per questi motivi, compromessi al ribasso, hanno portato in questo caso all'ampliamento della manovra, a fare pochi tagli e a mettere tante tasse, a non avere, ed è pericolosissimo, alcun progetto, nessuna linea strategica. Ebbene, non di questo comportamento, non di questa mentalità ha bisogno il Paese. Al Paese occorrerebbe continuare quel processo di ammodernamento che era stato iniziato, pur con ritardi e difetti, nella legislatura passata, ma di questo non si parla più. Anzi, si fanno passi indietro. Se penso a cosa sta succedendo nella mia regione Piemonte per quanto riguarda la TAV e l'autostrada Asti-Cuneo, devo essere non solo preoccupato, ma assolutamente arrabbiato.

Non solo si fanno passi indietro, ma si preannunciano da parte vostra volontà controriformiste - penso, ad esempio, alla legge sul lavoro - che, ripeto, assolutamente non vanno bene. Concludo dicendo: la presunzione, dunque la mancanza di concertazione, di coinvolgimento, dunque i dissidi della maggioranza sono fattori che, al di là di questo provvedimento, sono fonte di grave preoccupazione per il futuro del Paese.

il ricorso alla fiducia da parte del Governo fa interrompere in continuazione, in questo primo scorcio di legislatura, quel quel dialogo virtuoso tra maggioranza e opposizione attraverso cui si applica una norma costituzionale, quella della partecipazione dei cittadini, mediante le rappresentanze politiche presenti in Parlamento, alla gestione e alla definizione degli scopi e degli aspetti della gestione politica del nostro Paese. Lo abbiamo detto anche in altre circostanze, ci siamo anche permessi di evocare la responsabilità di chi ha, nel nostro ordinamento, nella nostra Costituzione, potestà, capacità e possibilità di intervenire su questo argomento, che è pericolosissimo. Infatti, come diceva Lelio Basso tanti anni fa, noi viviamo in un sistema democratico e il contenuto di democraticità si garantisce

fiducia su un provvedimento si interrompe il circuito virtuoso di colloquio tra maggioranza e opposizione. Questo è grave sotto il profilo politico, ma anche sotto il profilo costituzionale.

Paese? Volevo fare questa denuncia a nome del mio partito e del mio Gruppo perché noi non riteniamo che la politica sia uno scontro continuo. Siamo una forza politica che vuole il colloquio e lo dimostriamo nelle Commissioni giorno per giorno, quando cerchiamo di avviare un dialogo che - ahimè - non c'è, non per colpa nostra, ma perché i rappresentanti della maggioranza - in quest'Aula come nelle Commissioni

Viviamo in un Paese nel quale vi sono istituzioni nobili, ad esempio gli istituti e le scuole di formazione pubblica: l'Istituto diplomatico italiano, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola Vanoni per la formazione di alti dirigenti. Ebbene, non si può con un tratto di penna cancellare queste realtà,

affrontare il problema della formazione pubblica, ma sicuramente - disse queste testuali parole - queste benemerite scuole di formazione pubblica non possono essere cancellate così, se non attraverso un provvedimento condiviso in Parlamento. L'abbiamo vista la condivisione! C'è una norma che cancella la Scuola superiore, cancella l'Istituto diplomatico, cancella la Scuola Vanoni, cancella altre scuole per creare un'agenzia pubblica di formazione. Pensavo che il

vi rientra anche la formazione della dirigenza tecnica, finanziaria ed economica, attraverso la Scuola «Vanoni», che non è di oggi, ma è una scuola che esiste da tanti anni, non c'entra, non l'ha fatta il Governo Berlusconi! Si tratta di scuole consolidate, guidate per tanti anni da Ministri di

far accenno a qualcosa che è sgradevole - un mezzo per accontentare qualcuno che non è più parlamentare, non è più Ministro, ma vuol fare quello che faceva la funzione pubblica una volta: occuparsi della formazione della classe dirigente nel nostro Paese. Riguardo al anche colleghi della Margherita sono intervenuti in Commissione, pregando di non far cessare un'esperienza essenziale nell'emancipazione

per cambiare la dirigenza, si elimina; si trovano dei sotterfugi - che poi sono ridicoli, perché lo capiscono tutti - per azzerare questa classe dirigente. Teniamo conto che non è nemmeno un ente pubblico; è un'associazione, un consorzio in cui prevalenti sono i Comuni Allora i Comuni, le Province, le Regioni avrebbero dovuto segnare il cammino di una riforma del FORMEZ. Anche sul FORMEZ avevamo avuto delle garanzie che non sono state mantenute. Presidente,

Se la pubblica amministrazione è così centrale nelle politiche attive dei nostri giorni, negli obiettivi che voi e noi abbiamo per delineare l'orizzonte,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in conseguenza delle iniziative del Governo in materia economica e finanziaria è indubbio che i cittadini, soprattutto quelli più deboli, hanno ormai la percezione di un Governo nemico, che comprime la libertà di iniziativa, che crea nuove e più diffuse povertà, diffuse povertà, che considera i suoi cittadini come sudditi, ma soprattutto come presunti criminali fiscali da spiare e da controllare in ogni loro manifestazione. Chi produce profitto, chi si impegna rischiando propri capitali, chi si sacrifica per dare una speranza in più ai propri figli, chi svolge un lavoro professionalmente autonomo, chi sviluppa impresa è considerato un soggetto socialmente pericoloso, negativo, antisociale, quasi amorale che in quanto tale il Governo ritiene opportuno combattere e perseguire. Questo Governo ha fallito in ogni direzione, ma soprattutto nella parte che avrebbe dovuto maggiormente caratterizzare la sua azione politica: le fasce più deboli sono diventate ancora più deboli, i pensionati e gli operai hanno meno disponibilità economiche, la solidarietà sociale si è ridotta ad un semplice *slogan* e i cittadini con minori possibilità hanno minori opportunità di riscatto. Quello che mi preme sottolineare è che questo Governo non ha titolo a governare perché non ha una legittimazione elettorale e perché in Senato non ha una maggioranza di parlamentari eletti. Questo Governo si regge in modo esclusivo sulla base di un risultato elettorale ancora incerto e che dovrà essere definito attraverso il nuovo controllo delle schede e sulla base anche del voto determinante dei senatori a vita. Un risultato elettorale incerto non poteva legittimare la costituzione di un Governo con una maggioranza così ristretta e di fronte ad una situazione di così grande incertezza il rispetto verso gli elettori il senso dello Stato avrebbero dovuto indurre il centro-sinistra a percorrere la strada di un ritorno immediato a nuove elezioni. Sul secondo punto, che riguarda il voto dei senatori a vita, determinante per la permanenza di questo Governo, credo non si debba abbassare la guardia. L'articolo 1 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo: questo articolo è un pilastro fondamentale ed irrinunciabile a cui ogni altra ragione deve uniformarsi e piegarsi. Il valore assoluto di ogni democrazia si fonda sul voto dei cittadini e le maggioranze che sostengono un Governo devono essere costituite da rappresentanti democraticamente eletti. Quando questo principio viene disatteso si può determinare, come si è determinata oggi in Senato, una grave violazione delle regole democratiche. Questa non può definirsi democrazia, ma un colpo mortale per la democrazia stessa. Non possiamo tacere al Paese che il voto dei senatori a vita viene usato come un grimaldello per manomettere le regole democratiche. Soprattutto agli ex Presidenti della Repubblica, che hanno rappresentato l'unità nazionale, si chiede come si possa costituire un partito da usare sempre e comunque contro l'opposizione democraticamente eletta. Dobbiamo oggi guardare, visti questi comportamenti, ad alcuni messaggi inviati alle Camere non come frutto di un'esigenza di riflessione sui problemi delicati della vita del Paese, ma come strumenti di lotta politica. Emblematico è il messaggio sul pluralismo dell'informazione: un messaggio apparentemente fondato sull'esigenza di tutelare libertà e democrazia, che però oggi, alla luce di questi comportamenti, solleva il dubbio che sia stato strumento per sferrare un attacco al Governo Berlusconi e alla Casa delle Libertà. Un attacco che, richiamando quel messaggio, si è riproposto puntualmente con un disegno di legge vendicativo e punitivo come quello recentemente presentato dal ministro Gentiloni. A coloro che sono stato considerati i Padri nobili del nostro Paese, che hanno rappresentato le più alte cariche dello Stato e che hanno illustrato il nostro Paese per grandi meriti, rivolgiamo un invito perché non consentano di essere ascritti tra coloro che hanno affondato le regole della democrazia e che hanno soppresso la sovranità popolare. Questi elementi sono di per sé sufficienti per chiudere definitivamente una fase politica negativa, su cui incombe l'assenza delle regole democratiche, e aprire una fase politica nuova. Occorre infatti, e concludo, ricreare le condizioni perché vi sia certezza democratica e un Governo che sia in grado di garantire e tutelare i diritti di tutti i cittadini.

Non so se lei ha la stessa impressione, signor Presidente, ma la mia è che i colleghi del centro-destra abbiano sempre lo stesso schemino un po' consunto dall'inizio del dibattito.

della Commissione bilancio del Senato. È cambiata moltissimo perché dà, mette, assume, con diverse misure, un impegno maggiore nella direzione dell'equità e della giustizia sociale, rafforza e dà corpo ulteriore al lavoro per contenere i costi dello Stato. Pensate agli articoli e alle scelte che si fanno per diminuire i costi della politica, molto forti, molto importanti: per la prima volta, si va incontro ad un'esigenza che i cittadini sentono, ma anche ad un'esigenza, credo, della democrazia (con l'abolizione di tanti consigli d'amministrazione inutili, e ci sono nuovi contenuti per dare più spinta e più slancio all'idea dello sviluppo. Vi è un atteggiamento di attenzione verso i ceti più deboli, verso il mondo del lavoro, con misure come l'articolo 1 della finanziaria,

saranno redistribuite avendo come parametro fondamentale l'attenzione al mondo del lavoro e ai ceti più deboli. Così, per quanto riguarda uno slancio maggiore all'idea di sviluppo, viene data un'attenzione particolare alla piccola impresa, al mondo dell'artigianato. Leggetela, perché è davvero così. ho parlato della Commissione, ma forse dovrei parlare della maggioranza della Commissione, perché, purtroppo, l'opposizione di centro-destra si è dispersa in un meccanismo di ostruzionismo rifiutando l'idea di un confronto vero, di discutere questioni vere, di fondo, stando alla propaganda; l'abbiamo sentito anche qui. Lo direi ai colleghi del centro-destra, se ci fossero.

scuola - non ha materie prime, ma le compra, le trasforma e le vende: non vendiamo più niente, per dirla in un modo un po' rozzo. È una strada che porta all'impoverimento del Paese.

l'appello a leggere la finanziaria, come è stata trasformata dal lavoro della maggioranza parlamentare qui al Senato. Prendo la parte relativa ai trasporti e alle infrastrutture.

Non c'è l'abbandono dell'idea di realizzare le infrastrutture importanti per il nostro Paese (e anche la portualità è infrastruttura importante). Esiste

parte. Nascono nuove opportunità e nuove risorse, dando il via ad un processo che è sempre stata una delle richieste della portualità italiana: l'autonomia finanziaria. Anche questo sta scritto, chiedete agli operatori.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, come primo elemento non posso esimermi dal mettere in evidenza, innanzi tutto, l'entità di questa finanziaria: circa 35 miliardi di euro disegnano una manovra oggettivamente «pesante», mentre sarebbe bastata una manovra di circa 20 miliardi per rispettare le richieste europee. È stata invece respinta la proposta di stabilizzare il debito avanzata da una rete amplissima di economisti; è stata rifiutata l'ipotesi di spalmare la riduzione del debito su due anni. Dentro questa cornice, va collocata l'analisi del provvedimento, necessariamente articolata, che mette in luce i passi in avanti compiuti, i positivi elementi di discontinuità rispetto alle manovre del centro-destra, ma anche gli aspetti che inducono a gravi e fondate preoccupazioni. La manovra mette in atto, attraverso la riforma delle aliquote IRPEF e del nuovo regime di detrazione e assegni famigliari, una positiva redistribuzione verso la fasce di reddito basse, mentre quelle medio-alte subiscono un aggravio. Di fronte all'elevato livello di evasione fiscale, ritengo molto positivo l'impegno di questo Governo nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. La nostra opinione è che i 33 miliardi di gettito recuperati dovranno andare prioritariamente a migliorare la condizione dei ceti sociali più deboli, attraverso l'aumento della spesa sociale e dei redditi più bassi, come i lavoratori precari, i pensionati al minimo, gli incapienti. Giudico negativamente, invece, i pesanti tagli ai trasferimenti agli enti locali, che si tradurranno in addizionali IRPEF, nuove tasse di scopo, aumento dell'ICI, nonché in riduzione dei servizi sociali e aumenti delle tariffe. La prospettiva è che il saldo, tra vantaggi fiscali e aggravi sulla tassazione locale, sia, per larghi settori popolari, tutto negativo. Con una mano si dà, con l'altra si prende. A questo si aggiungono i tagli alla sanità. La rieintroduzione dei *tickets* è una misura che contestiamo profondamente perché iniqua e perché mette in difficoltà le persone più deboli come gli anziani e i migranti. Ritengo positiva l'esclusione dei *tickets* per i codici verdi del pronto soccorso, e su questo provvedimento c'è stato un impegno particolare del Gruppo di Rifondazione Comunista. Restano purtroppo confermati i *tickets* sui codici bianchi e soprattutto quelli di 10 euro sulle ricette, una misura, questa, che ha sollevato le giuste proteste dei pensionati, venuti a manifestare anche sotto questo Palazzo! Ma quali sono i settori che guadagnano maggiormente da questa manovra? Come ammesso dalla stessa Confindustria, sono innanzi tutto le grandi imprese e in particolare quelle produttrici di armamenti: a cominciare dalla riduzione di cinque punti del cuneo fiscale, dunque del costo lavoro, oltre 6 miliardi vengono destinati appunto alle imprese. Inoltre, il 40 per cento del taglio di questo cuneo, cioè del costo del lavoro, non ha riguardato i lavoratori dipendenti, come promesso in campagna elettorale, ma è stato usato per il recupero fiscale a favore di tutti i contribuenti indistintamente. Si tratta di risorse che, nonostante alcuni parziali incentivi, non vengono finalizzate alla creazione di nuova occupazione a tempo indeterminato, né a favorire l'ingresso delle donne nel lavoro, né a ridurre significativamente la piaga del lavoro giovanile precario. Ancora una volta si punta a un recupero di competitività internazionale basato sulla riduzione del costo del lavoro, come se non bastasse all'Italia avere uno dei più bassi livelli salariali in Europa e uno dei più alti tassi di flessibilità del lavoro e invece di affrontare in tempi stretti il superamento della legge n. 30 del 2003, oggi si parla di aprire un «tavolo per la produttività» per intervenire ancora di più sulla flessibilità degli orari incidendo anche sulle condizioni di lavoro. La scarsa competitività delle nostre imprese sta nella loro arretratezza tecnologica: infatti, destiniamo una delle più basse percentuali di spesa in ricerca e continuiamo a mantenere la gran parte dei nostri ricercatori in una situazione insostenibile di precarietà. Per quanto riguarda il settore della scuola, rilevo anche qui luci e ombre: importante la stabilizzazione di 150.000 lavoratori, sacrosanto mantenere le graduatorie per i precari, ma per il miglioramento delle strutture scolastiche sì prevede poco o nulla, mentre si destinano 150 milioni alle scuole private. Un'altra rilevante fetta di risorse viene destinata al finanziamento della cosiddetta mobilità lunga per 6.000 lavoratori delle grandi imprese, le quali potranno ristrutturarsi utilizzando risorse pubbliche per i prepensionamenti, mentre le crisi delle piccole imprese vengono scaricate duramente sui lavoratori in termini di licenziamento. Perché queste differenze di trattamento? Anche per questi lavoratori bisognerà prevedere al più presto adeguati ammortizzatori sociali. Un altro provvedimento che ha incontrato il dissenso dei lavoratori (penso ad esempio all'assemblea della FIAT dei giorni scorsi) è l'avvio dei fondi pensione senza un accordo preventivo nella coalizione. Da un lato, si è di fatto espropriata la volontà dei lavoratori in merito a una quota di salario differito con il meccanismo del silenzio-assenso; dall'altro lato, la nostra contrarietà riguarda la mancata attivazione di fondi pensione pubblici presso l'INPS, così come previsti nel programma dell'Unione. Il vero nodo è l'insufficiente copertura della pensione dopo la riforma Dini. È innanzitutto questa che va ripensata per garantire pensioni dignitose ai lavoratori giovani e ai precari. Ritengo comunque che qualsiasi intervento sulle pensioni debba partire da un aumento di quelle minime e debba essere concordato preventivamente attraverso una consultazione democratica dei lavoratori. Registro positivamente una misura sulla quale siamo riusciti a migliorare il testo qui al Senato: mi riferisco agli interventi di maggiore controllo sulle imprese volti ad affrontare la piaga delle morti sul lavoro, che solo nel 2005 sono state oltre 1.200! Ritengo importante a questo proposito l'impegno del mio Gruppo che ha determinato un accordo per l'assunzione di ulteriori 200 ispettori del lavoro. Giudico invece negativamente il fatto che non si è attuata una misura incisiva di contenimento dei costi della politica e soprattutto che non siano stati ridotti i compensi milionari dei *manager* pubblici. Infine, signor Presidente, desidero dedicare quest'ultima parte del mio intervento a uno degli aspetti più gravi di questa finanziaria: si prevede un aumento inaccettabile, visti i sacrifici che vengono chiesti ai lavoratori e ai pensionati, delle spese militari, cinque punti percentuali in più rispetto all'ultima legge di bilancio. Solo per nuovi investimenti nella difesa si stanziano 1.700 milioni di euro per il 2007: è quasi il doppio del bilancio di competenza dell'università e della ricerca! In tre anni saranno destinati complessivamente 4,5 miliardi di euro. Colleghi del centro-sinistra, in queste ultime settimane registriamo un clima di sfiducia (che commetteremmo un grave errore a sottovalutare), soprattutto da parte di quei settori sociali che hanno pagato duramente l'entrata nell'euro e che oggi senza alcun meccanismo di recupero del potere di acquisto dei salari (ruolo svolto in passato dalla scala mobile) si trovano a non arrivare alla fine del mese. Sono le fasce della popolazione che più hanno nutrito fiducia verso il nostro Governo, sperando, con l'avvio di una nuova fase, di uscire da una situazione al limite della sopportazione. Cito solo, ad esempio, come manchi ancora una politica seria di edilizia popolare; e le risorse chieste da Rifondazione sono rimaste purtroppo a livello simbolico. Numerose famiglie spendono per l'affitto o per il mutuo più della metà dei loro redditi; sono centinaia di migliaia gli sfratti previsti, un fenomeno sociale gravissimo, che non ha eguali tra i Paesi europei avanzati. come ho detto, la finanziaria contiene alcuni elementi positivi, ma purtroppo, anche molte cose negative. La voterò per senso di responsabilità e per impedire che si determini un quadro politico ancora peggiore di quello attuale. Detto ciò, superata questa finanziaria, ritengo che, invece di annunciare una «fase due» imperniata su riforme strutturali a base di elevamento dell'età pensionabile e di una generale liberalizzazione dei servizi pubblici da affidare ai privati, si debba tutti insieme rimediare a questo clima di sfiducia. Se il Governo Prodi vuole mettersi in connessione con il suo popolo,

Signor Presidente, colleghi senatori, credo sia davvero ingeneroso asserire che l'opposizione si sia in qualche modo sottratta al confronto: ne sono testimoni i colleghi della Commissione bilancio, ne è testimone il Paese. La verità è che ci siamo trovati di fronte ad una situazione abbastanza anomala: ci siamo trovati di fronte una legge finanziaria che poteva cambiare ogni ora, che poteva cambiare in ogni luogo e che, in effetti, cambiava, sfogliando anche le pagine dei quotidiani, da un giorno all'altro, ma non poteva essere cambiata dall'opposizione. Era una regola non scritta: sono stati respinti emendamenti di estremo buon senso,

ore e ore di trattative con la Confindustria per decidere come gestire tale misura del TFR, ad un dato momento, questo Governo di centro-sinistra - che aveva ed ha al suo interno una sinistra orgogliosa, che era partita con il manifesto «Anche i ricchi piangano» e non so più cos'altro - - permetterà all'opposizione di rimarcare, ed a quella sinistra in particolare, che è davvero curioso sottrarre la retribuzione differita di un lavoratore senza che sia nemmeno accolto l'emendamento che prevedeva di chiedergli la firma, perché questo è accaduto! Allora, francamente,

di dare a tutti i suoi membri la massima disponibilità nel ripulire il testo e nel migliorarlo nei suo aspetti tecnici), sotto l'aspetto politico, non vi sia stato un solo momento in cui questa maggioranza abbia inteso davvero dialogare, non solo con l'opposizione, ma con il Paese. Ed è per questo che oggi si registra un isolamento che, francamente, si manifesta come circolare, perché coinvolge, in maniera assolutamente non discriminata, tutti i settori del Paese, da ultimo anche i rettori, che - a quanto mi è parso di capire - si in una sorta di interdizione all'accesso alle università per il Governo; ma non solo i rettori: dovevano piangere i ricchi, ma è finita che fischiavano gli operai.

ci è stato spiegato che rimaneva invariata la previsione strutturale dei 5 miliardi di aumento di entrate per il prossimo anno. Questa

l'opposizione non può essere in qualche modo imputata di questa rigidità che, per contro, all'interno della maggioranza era invece assolutamente molle e flessibile. È vero che è cambiata la finanziaria nel maxiemendamento, è vero che è cambiata rispetto a com'era uscita dalla Camera, ma è cambiata accentuando i suoi aspetti stravaganti, con queste curiosissime norme sulla rottamazione (su cui altri si sono soffermati), è cambiata creando sistemi di agevolazione per le società quotate in Borsa che gestiscono gli immobili, che sono più agevolate del singolo proprietario di una singola casa che affitta. È cambiata perché è diventata più surreale, non più solida, non più credibile, non più vicina alle critiche che venivano da tanti settori e da tante fasce del Paese. se questo è il momento di scarsa lucidità che ha vissuto il dibattito interno alla maggioranza e quindi poi, inevitabilmente, la relazione che si è stabilita con l'opposizione, io credo che più del nostro dovere, che è stato quello di contrastare con argomenti questa manovra, con proposte che erano fattualmente perseguibili, con richieste logiche anche di rispetto della dignità delle parti sociali e dei lavoratori, più di questo non credo che ci si potesse chiedere. Lo abbiamo fatto e abbiamo anche avuto la capacità di appassionare il Paese intorno al tema della finanziaria. Io non sono una persona che indulge facilmente alla propaganda, lo dico con franchezza: l'enorme manifestazione di piazza San Giovanni, non è stata la causa delle difficoltà in cui si dibatte, in questo momento, il governo Prodi, non è stata una prova muscolare del centro-destra, ma è stata lo specchio dei danni che ha provocato questa maggioranza in poche settimane, allontanandosi di una distanza siderale da qualsiasi rapporto con quello che un tempo veniva chiamato il Paese reale, ma che io oggi chiamerei più che altro i segmenti sociali che, in fondo, avevano anche favorito la vittoria di questa maggioranza. Questo è ciò che è successo. Se poi qualche collega, anche nella foga del dibattito,

diventerà moneta sonante nelle buste paga dei cittadini, nelle delibere che alzeranno le tasse nei Comuni, nelle delibere che reintrodurranno i *tickets* e che alzeranno le tasse nelle Regioni. Mano a mano che tutto questo accadrà, la mobilitazione di questo Paese per ridurre lo spazio di sopravvivenza della vostra coalizione credo che diventerà sempre più incessante e sempre più tambureggiante.

farà al nostro Paese. I tanti interventi hanno toccato in modo molto interessante parecchi aspetti. Io vorrei toccarne un numero molto ristretto. Intanto, dal punto di vista economico, che dovrebbe essere ed è il punto principale di questa manovra, si si potrebbe sintetizzare in questo modo: noi, il Governo Berlusconi, riducendo le aliquote delle imposte siamo riusciti a far salire il gettito; manovra abbiamo sicuramente un ampio aumento delle aliquote e delle imposte, quanto al gettito vedremo i risultati: sicuramente ci saranno coloro che pagheranno che pagheranno di più, ma il gettito bisognerà vedere come andrà, perché purtroppo le attività di molti subiranno un netto peggioramento con conseguente riduzione dell'imponibile, e quindi, anche aumentando le aliquote, c'è il rischio di una riduzione del gettito, per cui si crea allo Stato, un danno ai cittadini, una riduzione della libertà dei cittadini. Questa finanziaria, però, non si accontenta di toccare l'ambito economico, ma spazia su ogni ramo dello scibile e della legislazione. Dalla coalizione che si batté con tanto impegno nella campagna referendaria opponendosi a qualunque modificazione della Costituzione in nome della salvaguardia del ruolo del Parlamento,

iniziata sette mesi fa, la maggior parte dei provvedimenti viene approvata con un voto di fiducia; con pochi voti, per di più vincolati dalla fiducia, si fa la maggior parte della legislazione.

le Camere, in realtà, sono ridotte a mera ratifica di decisioni prese altrove, a volte all'ultimo momento, spesso raffazzonate anche dal punto di vista formale e molto spesso rovinose per il Paese.

ma la finanziaria dovrebbe limitarsi al compito che la legge le affida, e cioè effettuare gli aggiustamenti dei conti e assumere provvedimenti di carattere finanziario necessari al buon andamento dello Stato per l'anno seguente.

«Con l'occasione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi

su un modo di legiferare - invalso da tempo -» (non si limitava solo all'ordinamento giudiziario) «che non appare coerente con la *ratio* delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata "articolo per articolo e con votazione finale"». L'insieme di quanto ho detto spingerà con assoluta certezza me a votare contro questa legge finanziaria. Spero che il presidente Ciampi, alla luce di quanto scrisse al Parlamento, vorrà quanto meno astenersi dal votare, seguendo in questo una prassi di posizione *super partes* assunta generalmente dai senatori a vita, dagli ex Presidenti della Repubblica, soprattutto su questo su questo provvedimento che moltiplica per cento le anomalie che egli segnalò due anni fa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono tra coloro che auspicava un maggiore coraggio da parte del Governo nella direzione di una redistribuzione vera delle ricchezze di questo Paese, in un aiuto concreto per i meno abbienti, in sforzi reali per dare dignità al lavoro, sicurezza e per garantire comunque a questo Paese, che è stato devastato dal precedente Governo, un minimo di equità e di possibilità di futuro. Alcuni sforzi sono stati fatti, ma credo che, nella sua completezza, questa finanziaria non corrisponde al programma che avevamo elaborato elaborato per il Governo, anche se a giustificazione di certo vi sono i gravi precedenti in relazione alla questione del bilancio e alla questione della ricchezza da crescere. Talvolta, però, mi pare che sia dato più ascolto agli umori della Confindustria che alle reali esigenze della classe operaia, del precariato e di tutte quelle persone che in questi anni si sono impoveriti di fronte, appunto, ad un ad un Paese che portava le divergenze di reddito ad alti livelli, anche con é*scamotage* da condoni a quant'altro. Credo che anche sull'ambiente lo sforzo poteva essere maggiore, ma di questo parleranno altri colleghi durante il dibattito. Mi vorrei soffermare essenzialmente su un *vulnus*

In effetti, è molto difficile dire alle persone di dover fare sacrifici perché non vi sono risorse, che è necessario stringere un po' la cinghia per far crescere questo Paese, Paese, non trovare i soldi per gli emofiliaci e trovarli per le spese di armamento e di distruzione. È difficile dire a un precario di portare ancora pazienza perché per ora non riusciamo ancora a strutturare un lavoro dignitoso con le garanzie necessarie e poi, invece, appunto dare soldi ai generali, alle armi e su questo settore investire. Poiché, però, parte del Governo e anche della maggioranza hanno detto che non è vero che vi è stato un aumento delle spese militari, preferisco leggere, perché rimangano agli atti, gli esatti numeri per cui posso dire e dico che purtroppo vi è stato un forte aumento nel settore armiero. La spesa militare mondiale ha raggiunto livelli molto allarmanti, avvicinandosi pericolosamente ai record della Guerra Fredda e non stupiscono i ripetuti appelli alla sua drastica riduzione lanciati da James Wolfensohn, negli ultimi anni della sua presidenza della Banca Mondiale. Nel 2005 la spesa globale ha raggiunto il record di 1.118 miliardi di dollari, che corrisponde al 2,5 per cento del prodotto lordo globale e a una spesa media *pro capite* di 173 dollari per ogni abitante del pianeta.

L'Italia é al settimo posto e con una spesa *pro capite* di 468 dollari; e, in base alla spesa *pro capite*, l'Italia si colloca al quinto posto: dopo gli USA

Finmeccanica - con un ruolo dello Stato che resta centrale nella sua proprietà - è il decimo gruppo industriale al mondo per produzione di armi e, come ha ricordato 1'«Herald Tribune» dello scorso 6 settembre, il nostro Paese è il secondo al mondo per le esportazioni mondiali di armi leggere. La nota aggiuntiva 2007 del Ministero della difesa continua a sostenere che la spesa militare italiana corrisponde allo 0,84 per Una percentuale che contraddice quella della NATO, che la calcola all'1,8 per cento, e quella del SIPRI (Istituto di ricerche sulla pace di Stoccolma), l'organismo indipendente, che nel suo annuario 2006, basato sulla media dei dati resi noti dai maggiori organismi internazionali responsabili di difesa e sicurezza, la fissa al 2 per cento. Rispetto al 2006, con un totale di 18.787,2 miliardi di euro, la finanziaria 2007 porta il totale a 21.364,5 miliardi: un aumento del 13,7 per cento, che comprende l'incredibile fondo di 1,7 miliardi previsto al comma 492 dell'articolo 18. Credo non ci dovrebbe preoccupare tanto la spesa per il personale, anche se incide con la percentuale abnorme - un'altra anomalia italiana - di oltre il 72 per quanto piuttosto quella per armamenti, che anche il Governo attuale sembra, in modo miope, voler incentivare: la portaerei Conte di Cavour (quasi un miliardo di euro, sistemi d'arma esclusi),

Il programma di governo dell'Unione 2006-2011 contiene tre riferimenti alla necessità di politiche di disarmo. a pagina 90: «Un'azione concertata nella lotta al terrorismo come minaccia globale e per il rafforzamento dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica deve essere affiancata da un rinnovato impegno per la lotta alla povertà, per il disarmo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa». Sempre nel programma di governo dell'Unione si legge, a pagina 91: «Sulla base dello spirito originario della legge 185/90, (commercio delle armi), l'Unione si impegna a che vi siano trasparenza e un più cogente rispetto delle disposizioni che impediscono il commercio delle armi in Paesi che violano i diritti umani o che siano collocati in aree di conflitto, nonché a sostenere l'adozione in ambito ONU di un trattato internazionale sul commercio delle armi. Come terzo punto, sempre in quel programma, a pagina 109, leggiamo: «L'Unione si impegna, nell'ambito della cooperazione europea, a sostenere una politica che consenta la riduzione delle spese per armamenti». Purtroppo, signor Presidente, non trovo nulla di tutto ciò nella finanziaria 2007. La spesa per armamenti è spesa di morte e viene riconfermata. Chiedo pertanto al Governo che: in primo luogo, avvii urgentemente l'attuazione dei tre punti citati del programma, sulla base del quale è stato votato; che l'Italia chieda all'Unione Europea di avviare iniziative per il disarmo globale, graduale, ma certo; in terzo luogo, che il nostro ambasciatore alle Nazioni Unite, dove l'Italia è, dal prossimo gennaio, membro del Consiglio di Sicurezza, riceva istruzioni precise per iniziative in sede ONU a favore di una nuova stagione di disarmo multilaterale; e, infine, che, con la prossima legge finanziaria, le spese per armamenti vengano ridotte. Presidente, le notizie secondo le quali vi era stata una riduzione della spesa militare all'interno della finanziaria, o comunque un non aumento, sono purtroppo notizie che non corrispondono al vero. Credo che il Governo si debba impegnare seriamente sui tre punti che erano parte del programma dell'Unione e che debba impegnare seriamente l'Italia come membro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

varie associazioni, e, onestamente, che debba ascoltare il buon senso, se vogliamo davvero far capire che dobbiamo sforzarci, che vogliamo costituire un Paese nuovo, che ogni soldo è utile per aiutare gli ammalati, per aiutare i bisognosi, per aiutare le aziende a crescere, cioè tutto ciò che vogliamo, credo, sia maggioranza che opposizione. È ormai inaccettabile che un tale mare di soldi venga dato per la morte e, tra l'altro, speso anche malissimo, venga dato a un sistema che non solo non porta ricchezza ma rischia di gonfiare, come evidenziano gli economisti più avvertiti a livello internazionale,

Presidente, l'Italia è sopravvissuta alla corruzione giolittiana, alla dittatura fascista, al Sessantotto, al

tant'è vero che smentisce tutti i catastrofismi e i «declinisti». Ha smentito l'Ufficio studi della Banca d'Italia e ha smentito il professor Innocenzo Cipolletta dell'Ufficio studi di Confindustria, il quale è stato ben remunerato dal Governo di centro-sinistra per le sue menzogne. Ha smentito anche grandi economisti o ritenuti tali. Il CENSIS parla di un *boom* silenzioso che era già iniziato quando gli altri declinavano il «declinismo». Era già iniziato l'anno scorso, nel 2005. Consiglierei anche ai colleghi della sinistra

era forte prima che questo Governo si insediasse. L'IRES è cresciuta di 3,5 miliardi di euro grazie alle norme introdotte nel 2005

Il livello delle esportazioni del quarto trimestre del 2005 era identico a quello del secondo trimestre del 2006. L'Italia nel 2005 esportava già

salvato il Paese. Dall'altra parte, c'è la FIAT in ripresa perché il Governo Berlusconi disse alla famiglia Agnelli di impegnare i loro soldi nell'impresa e non più di finanziarla, come avveniva in passato. Signor Presidente, a proposito delle polemiche Nord‑Sud, saprà certamente che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno è costato meno di quanto lo Stato italiano ha speso negli ultimi 50 anni per sostenere la FIAT. Ancora, in questa finanziaria ci sono le tracce di questo tipo di politica; c'è la mobilità lunga per 6.000 operai della FIAT e c'è la disperazione e la disoccupazione per i dipendenti delle piccole imprese. Ci sono le agevolazioni alle società immobiliari quotate in Borsa, come la Pirelli, e ci sono invece le penalizzazioni per il pensionato proprietario di un piccolo appartamento. Questa è l'Italia del centro-sinistra, questa è l'Italia che vede un Governo contestato all'interno della sua stessa coalizione. coalizione. Abbiamo ascoltato i colleghi del centro-sinistra polemizzare con questa finanziaria e dire che è una finanziaria da buttare. Gli italiani questo lo hanno capito e per questo si mobilitano nelle piazze, per questo contestano Prodi nelle piazze e per questo noi, del centro-destra, abbiamo un grande compito, quello di salvare il Paese

dico subito che domani voterò la fiducia al Governo, semplicemente perché sono convinto che a questo sono vincolato dal voto degli elettori che mi hanno portato qui. Certamente mi hanno votato perché il centro-sinistra sostituisse il Governo Berlusconi che ci ha preceduto, e quindi non vogliono che io adesso faccia cadere questo Governo. Ma se dovessi esprimere in questo voto la mia valutazione di questa finanziaria, devo dire che il mio voto non potrebbe che essere negativo. Voglio ricordare solo due punti, due norme - per così dire - che non avrebbero dovuto esserci in questa finanziaria, e che invece ci sono. La prima questione è scoppiata oggi, e la leggeremo sui giornali di domani: il comma 1346: una normetta di poche righe, per iniziati. È una di quelle norme che, se non si ha un'approfondita cultura giuridica alle spalle, non si capisce cosa dicano.

Una cosettina da niente. Senonché l'effetto di questa norma è una sanatoria generalizzata per gli amministratori pubblici che sono in questo momento davanti alla Corte dei conti assoggettati al giudizio per avere arrecato danno all'erario. La gran parte di questi giudizi - il procuratore generale davanti alla Corte dei conti ha scritto stamattina ufficialmente al presidente Salvi una lettera - andrà in fumo, andrà prescritto;

questa proposta di modifica era andata nella cosiddetta cabina di regia, dove la maggioranza considerava e valutava le modifiche da fare. Nella cabina di regia è stato detto un secco no; la maggioranza in Senato aveva detto con chiarezza che quella modifica non si doveva fare. La proposta di emendamento era stata respinta. Ma quella porta che era stata chiusa, nottetempo è stata riaperta qualcuno. E si è voluto fare una sanatoria, perché bastava aggiungere poche parole: il presente comma non si applica ai giudizi in corso. Bastava scrivere questo per evitare il problema, che invece Un principio, tra l'altro, di civiltà giuridica. Questa innovazione non viene chiesta oggi per la prima volta. È almeno una dozzina di anni che si prova a modificare quella norma sulla responsabilità davanti alla Corte dei conti. stata sempre respinta. Io stesso l'ho fermata più volte. Dietro - diciamolo - c'è il mondo degli amministratori, in particolare il mondo delle autonomie. Guardate, in modo del tutto trasversale, quindi non mi applaudite da quei banchi lì di fronte, perché ci sono anche i vostri dietro queste cose. queste cose. Il mondo delle autonomie è un pilastro della nostra democrazia, ma sappiamo anche - e lo sappiamo perché oggi ce lo dicono i giornali e le inchieste - che è un mondo nel quale bisogna riportare ordine.

Si deve intervenire: secondo me il presidente Marini dovrebbe - e lo può ancora fare - dichiarare inammissibile questo emendamento perché è ordinamentale, non ha posto in una finanziaria ed è senza copertura, perché siccome non farà pagare il risarcimento allo Stato, ovviamente costa

La seconda questione riguarda il tetto ai superstipendi. Con il senatore Salvi ed altri autorevoli colleghi avevamo proposto una norma che poneva un tetto generale alle retribuzioni pubbliche parametrandole a quella del primo presidente della Corte di cassazione.

caso la maggioranza in Senato era d'accordo, perché questo emendamento da noi proposto ha ricevuto l'assenso della cabina di regia e quindi della maggioranza.

ma si è ridotta grandemente nell'applicazione, perché ora - per certe tecnicalità che non è importante citare - si applica solo ad una frazione minimale dei dirigenti pubblici.

Io credo che queste cose vadano dette in chiaro. Come ho già detto voterò la finanziaria,

ma quando si fanno le cose giuste, non quando si fanno le cose sbagliate. Io voterò la finanziaria perché gli elettori mi hanno votato per mi hanno votato per sostenere questo Governo. Ma non hanno votato questo Governo perché facesse queste politiche. Qui c'è una contraddizione che bisogna sciogliere. I fischi che ha ricevuto il Presidente del Consiglio, le nostre orecchie di parlamentari che fanno il loro mestiere sul territorio li avevano già sentiti, e da tempo. E se qualcuno ce lo avesse chiesto, avremmo potuto avvertire che erano in arrivo. allora, che dobbiamo recuperare il senso di una vicinanza all'opinione pubblica di questo Paese, dobbiamo ritrovare le correnti profonde, perché appunto non si governa con i sondaggi, ma quando si avvertono e si prendono le correnti profonde e non quando si favoriscono e si praticano clientele e favoritismi, non quando si va contro quello che si è promesso agli elettori. Dov'è, voglio chiedere al presidente Romano Prodi, l'impegno per la trasparenza, contro i costi impropri della politica, che è nel programma elettorale del centro-sinistra, e che lo stesso Presidente ha più volte richiamato?

che sia sfuggita anche all'esame della Commissione bilancio, perché comunque questa norma determina una riduzione delle entrate, non ci sono santi. Non vedo il Sottosegretario presente, ma credo che anche il presidente Morando abbia abbia avuto chiarezza di ciò dopo che c'è stato l'esame in Commissione. Non so, perché entriamo in un campo opinabile di prassi parlamentare, ma, come Presidente di turno, vorrei segnalare al Governo, nella sua assoluta

ad una operazione di questo tipo, dico subito che non ho alcuna difficoltà a chiedere al Presidente del Senato di conferirmi nuovamente la possibilità di convocare la Commissione bilancio.

la Presidenza del Senato mi autorizza a riconvocare la Commissione per esaminare quella norma - solo quella norma - e proporre qualche soluzione, io non ho alcuna esitazione a farlo. Per le vie Per le vie brevi, lei lo sa, avevo provveduto a qualche consultazione per vedere se questo era possibile, ma non avevo avuto un riscontro positivo. Se questo riscontro

manomissione del testo oggetto della fiducia. Se, invece, l'opposizione dovesse in qualche modo convenire sull'opportunità comunque di espungere questa parte del testo dal nostro esame, io non avrei alcuna difficoltà a convocare la Commissione per verificare se la Commissione abbia quest'orientamento, per poi tornare in Aula ed eventualmente formulare un consiglio al Presidente del Senato. Se lei mi dice questo, io senz'altro provvedo.

l'importante dichiarazione del Presidente della Commissione bilancio, insisto con il Presidente del Senato perché convochi al più presto la Commissione bilancio. mi pare che la soluzione prospettata dal presidente Morando sia condivisibile. Naturalmente, non c'era stato il tempo materiale per verificare tutta

a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, alla richiesta di modifica della norma introdotta. Al di là delle coperture, è intollerabile che esistano cittadini che non siano uguali di fronte alla legge. Ritengo sussistano le condizioni per potere riparare ad una norma così inaccettabile.

venga riportata in Commissione, ovviamente sottolineando il fatto che purtroppo il «nottetempo» ha provocato molti problemi,

noi ci rendiamo conto dei contenuti importanti e salienti di questo comma, pertanto siamo ben d'accordo e disponibili a trovare soluzioni. Certo è che non si può toccare questo testo;

sono dispostissimo alla riconvocazione della Commissione bilancio per esaminare la questione. Sulla base di una scelta del Presidente del Senato di conferirmi l'esame di questo punto della legge finanziaria per verificare se si possa dare dare luogo ad una decisione diversa da quella assunta stamattina, io questo incarico me lo prendo, ma solo se siamo tutti d'accordo nel ritenere che sarebbe meglio espungere il Governo è disponibile, io sono disponibile a mia volta a convocare la Commissione bilancio e a verificare se c'è questo consenso. Se i Gruppi dell'opposizione, in particolare, sollevano una questione procedurale sull'intangibilità del testo, io mi guardo bene dall'insistere su questa proposta, sia ben chiaro.

trattare la questione perché obiettivamente non ci sono le condizioni minime perché questo possa avvenire.

l'orientamento è quello di continuare con l'ordinario programma dei lavori che era stato stabilito. Questa è la posizione di Forza Italia;

Presidente, senatrici, senatori, rappresentanti del Governo, è stato detto ieri, nella discussione sul bilancio dai banchi dell'opposizione, che questo è un Paese dove le famiglie hanno una larga propensione al risparmio. Lo era, si potrebbe dire, prima del Governo e delle politiche neoliberiste del centro-destra. Tutti i giornali ieri davano la notizia che il 20 per cento delle famiglie è a rischio di insolvenza e che c'è un allargamento della fascia di povertà. Si può vedere, nella condizione sociale del nostro Paese, che in questi cinque anni si è fatto un grande balzo all'indietro, che le condizioni materiali di vita e di lavoro sono largamente peggiorate in proporzione diretta con il mancato intervento pubblico in economia, con le privatizzazioni, con la demolizione del sistema del *welfare* (costruito dal compromesso tra capitale e lavoro nel 1900), con i processi di deregolamentazione del mercato del lavoro. lavoro. Nei Paesi dove queste politiche sono state portate avanti con maggiore durezza le conseguenze sono maggiormente devastanti: è il caso del nostro Paese. [**Presidenza del che la legge n. 30 del 2003 fa uscire dal lavoro nero: non è così. Con la legge n. 30 non c'è più bisogno di lavoro nero perché quella legge ha invertito una tendenza secolare del diritto al lavoro, ha dato veste giuridica alle frammentazioni del lavoro preesistenti nei rapporti piuttosto che ambire a ricomporli e ad unificarli.

così dire liberi fischi in libero «Motor Show», ma quelli di una giovane classe operaia inserita in un processo produttivo che chiede alla politica di rendersi consapevole del carattere della globalizzazione e della costruzione che ha presieduto al suo affermarsi, ivi compreso l'uso della guerra preventiva, facendo crescere una critica di massa che, risalendo agli effetti devastanti di quella politica, migliori la sua condizione. chiedono alla politica di recuperare la sua capacità di porre la questione del lavoro nel suo valore (sia nel senso della critica al lavoro produttivo che in quella di un'indagine sulle possibilità del lavoro vivo), al centro della sua iniziativa, di assumere cioè l'orizzonte del lavoro come espressione della vita umana in quanto tale e, per questa via, la ricerca di nuove e più adeguate forme per la comprensione e la trasformazione dei fenomeni sociali. Ed è rintracciabile, io credo, da questo punto di vista (e per questo voto la finanziaria, la fiducia, e con me il mio Gruppo, pur tra le differenze che anche qui sono state legittimamente espresse), un tratto comune nei contenuti della finanziaria: c'è un cambiamento di tendenza, di inizio di lotta alla precarietà e all'insicurezza delle condizioni di vita e di lavoro. Credo che i risultati siano significativi: primo tra tutti, le modalità con cui si sono affrontate le questioni della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche dopo le drammatiche vicende di Campello sul Clitunno. Penso all'assunzione dei 300 ispettori, alla costituzione di un fondo per le famiglie

i livelli di diritto dei lavoratori in condizioni di precarietà, dalla maternità a rischio alle condizioni della malattia ed ai suoi contenuti.

significativa, seppur insufficiente, è la possibilità per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti di assumere LSU e LPU. Su questo però vorrei dire,

il Governo avrebbe potuto ascoltare di più chi proponeva nei contenuti della finanziaria un allargamento e un consolidamento a tempo indeterminato per tutti quei lavoratori. Ieri vi è stato, significativamente, un accordo, nell'azienda che, appunto, trasforma quei rapporti di lavoro: è il frutto anche, ovviamente, di un avanzamento del Governo; ma è il frutto, soprattutto, della testardaggine di quei precari e della loro lotta. Inizia così, anche attraverso questa via, una lotta reale alla condizione di precarietà e insicurezza della nostra società. finestra"). Colleghi, prima di lasciare la parola alla senatrice Negri, debbo chiudere due questioni rimaste aperte questa mattina. Avevo chiesto un momento di approfondimento rispetto all'ammissibilità di due punti del maxiemendamento. In una lettera, il ministro per i rapporti con il Parlamento Chiti poneva due questioni: una è stata risolta questa mattina; la seconda riguarda il comma 1119 (la questione dei CIP 6 sull'energia).

un errore materiale. Il secondo caso lo abbiamo risolto in senso positivo; ma, per quanto riguarda il CIP 6, nella stesura del comma si si parla di: «impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione», parole che andrebbero sostituite con le seguenti: «già realizzati ed operativi». Ora, con tutta la buona volontà - ho avuto modo di approfondire molto bene tale aspetto, che tocca interessi importanti - questo non può essere considerato un errore materiale; è un cambiamento delle cose, quindi, lasciamo il testo così com'è. La seconda questione che era rimasta aperta riguardava qualche dubbio di costituzionalità, già emerso in Commissione (era stata

Sono state sollevate questa mattina in Aula - ma precedentemente anche in 5ª Commissione, come riferito dal presidente Morando - alcune perplessità in ordine alla presenza nell'emendamento 1.1000 del comma 836, che apporta modifiche all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, in materia di entrate della Regione. Dal punto di vista della legittimità costituzionale, l'articolo 54 dello Statuto, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, autorizza la modifica delle norme del Titolo III dello Statuto medesimo, con legge ordinaria «su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione». E come risulta dagli atti del Consiglio regionale, quest'ultimo si è espresso favorevolmente in materia con risoluzione approvata il 24 ottobre di quest'anno. Per quanto concerne poi la genesi della norma in questione, va innanzi tutto premesso che essa costituiva inizialmente l'articolo 102 del disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 1° ottobre scorso (Atto Camera n. 1746). Tale norma, passata senza osservazioni attraverso il vaglio della Commissione affari costituzionali della Camera, diventava poi - a testo invariato - il comma 437 dell'articolo 18 del testo sul quale il Governo poneva la questione di fiducia alla Camera. Trasmessa la legge finanziaria al Senato, la 5ª Commissione non esprimeva osservazioni sulla norma in questione in sede di esame preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. La Commissione affari costituzionali trasmetteva a sua volta alla Commissione bilancio un rapporto favorevole, senza alcuna osservazione sul punto in questione. Il comma 836 dell'Atto Senato n. 1183 non presenta, quindi, aspetti di incostituzionalità. Queste erano le due risposte che dovevo dare. C'è ancora una comunicazione che riguarda

La mia è stata una riflessione che non può dar luogo ad alcuna ambiguità:

Naturalmente, con una visione costruttiva dei nostri rapporti interni, ho detto al presidente Morando che, se attorno a questa norma che ha suscitato parecchie perplessità e parecchie contrarietà, si trovasse un punto d'incontro tra tutti i Gruppi,

che precedenti importanti e strumenti del nostro sistema giuridico-amministrativo dimostrano che vi è la possibilità e vi sono gli strumenti, per il Governo, di intervenire immediatamente per risolvere un problema come questo che tocca la sensibilità di moltissimi nostri senatori. Questo strumento c'è, domani il Governo chiuderà la discussione e io mi auguro che si possa indicare una soluzione soddisfacente. [DE Signor Presidente, purtroppo, devo permettermi di non apprezzare la sua decisione per quanto riguarda

norma, perché, avendo fatto questo errore materiale e quindi sostituito la parola «realizzati» con «autorizzati» il resto del testo, Presidente, mi permetto

pensare che ci possa essere un decreto, questo è scritto nella norma, per poter valutare le eventuali deroghe. È palesemente un errore materiale.

ovviamente dopo un'attenta discussione e una valutazione anche di tutte quante le norme. Per di più è evidente

su due errori materiali e mi pare che il criterio finora usato tendeva ad affermare che veniva riconosciuto errore materiale quello su cui eravamo tutti d'accordo e errore non materiale, al di là della norma stessa, quello su cui qualcuno - chissà perché

a questa norma. Qui non si tratta di un refuso; il Governo ha deciso di fare diversamente. Oggi la maggioranza ha ribadito il no.

ci dica come è stata inserita questa norma, violando l'impegno verso la maggioranza di mettere nel maxiemendamento quello che la maggioranza aveva concordato e come vuole rimediare a questo errore.

«Il Ministro può emanare il decreto per eventuali deroghe agli impianti autorizzati». Quindi, è una norma inapplicabile. Ci sembrava di buon senso accogliere la sollecitazione del Governo. Tuttavia, visto che ci sono anche molte agenzie di stampa che fanno affermazioni contraddittorie, soprattutto del ministro Bersani, chiedo formalmente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento domani venga in Aula, in apertura dei lavori, per dare l'interpretazione autentica che il Governo dà su questa norma.

del presidente Matteoli, vi è un problema. Ritengo che sia indispensabile, dopo aver letto la posizione del ministro Bersani, che il Governo dica con chiarezza qual è la posizione sul CIP 6; se il Governo intende «realizzati» o «autorizzati». Diventa un punto dirimente rispetto al un giudizio che diamo sulla norma.

è stata dibattuta in Commissione, come viene discusso in questo momento *a latere*. Essendo emendamento del relatore e non l'emendamento di un senatore che è stato preso e inserito,

Diversamente, prendiamo atto che il Governo insiste nel mantenimento di questo comma e alle forze di maggioranza spetterà decidere se questo abbia un peso tale per votare o no la fiducia al provvedimento.

riconosce che la definizione di errore materiale richiede necessariamente la condivisione di tutta l'Assemblea perché è un elemento essenziale. Tuttavia, il Governo vuole ribadire che di errore materiale si tratta perché

del comma 1119 e la previsione del comma 1120, laddove nel primo si definisce che sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi agli impianti già autorizzati e nel secondo si prevede un decreto che potrebbe riconoscere in deroga Faccio presente tra l'altro che, in questo modo, cassando dal comma 1119 le parole «impianti già operativi» non si dà certezza a questi impianti. ritengo che l'opposizione avrebbe potuto, nell'interesse della chiarezza della norma, accettare questa classificazione di errore materiale. Tuttavia, poiché questo non è avvenuto,

il comma 4 dell'articolo 1 del maxiemendamento, recuperando un po' l'anima di questa manovra, che si dice l'abbia persa per strada, contiene un'osservazione importante, vale a dire che le maggiori entrate tributarie realizzate nel 2007 rispetto alle previsioni saranno naturalmente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; se eccedenti però saranno finalizzate a ridurre la pressione fiscale per conseguire quegli obiettivi di sviluppo e di equità sociale e saranno destinate ai soggetti incapienti. Questo comma, come dicevo, secondo me qualifica politicamente - è una sorta di manifesto politico di sintesi - il lavoro fatto dal Senato anche rispetto all'importante lavoro della Camera e capita esattamente nel cuore del dibattito che si sta facendo, e che fa particolarmente l'opposizione, sull'eccesso di introiti e di risorse che verrebbero dalla tassazione e sulla loro vana finalizzazione.

(ci invitava il senatore Mazzarello a prenderne visione). Sono stati anzitutto previsti provvedimenti efficaci sul tema della sicurezza, riconoscendo la specificità contrattuale dei lavoratori della pubblica sicurezza, significativi interventi nell'ambito degli enti locali, ad esempio la compartecipazione dinamica dell'IRPEF per il 2007. Sono state trovate importanti risorse per il contratto dei dipendenti pubblici, per il trasporto locale. In particolar modo, si è forse riusciti a sanare quella cesura, quella ferita, che, vale la pena di riconoscerlo, si era prodotta con il grande mondo della piccola impresa e dell'artigianato, con le misure di successione e le misure fiscali. Vale a dire, si è posto un rimedio politico a un problema squisitamente politico, che anche impropriamente, con un certo azzardo, era stato aperto.

più. Comincerà infatti a operare su uno dei cardini del processo produttivo, cioè sul lavoratore, l'effetto benefico del cuneo fiscale; certo, meno di quanto si sarebbe sperato, certo spalmato sulle nuove curve dell'IRPEF. forse lecito calcolare che tra l'effetto del cuneo fiscale, gli effetti delle detrazioni, specialmente per le famiglie numerose, l'innovazione dell'assegno familiare, portato fino a 21 anni nel caso di figli con lavoro non regolare o studenti,

Certo, ci sarà una quotidianità verificabile e degli effetti sulla quotidianità di tanti milioni di persone di un meccanismo di minor

perché doveva affrontare un'economia malata. L'opposizione continua a dire che l'economia non era malata, che il*deficit* non c'era, che il debito non era in una situazione critica

L'opposizione rifletterà - anche se ora non vuole riconoscerlo ‑ se la sua conduzione degli emendamenti presentati in Commissione bilancio si qualifichi o no come tecnica ostruzionistica, ma certamente non mi

delle risorse dalle tasche dei cittadini a ipotetici ministeri spreconi e clientelari, con poco rispetto per la formalità dell'Aula e del lavoro dei singoli senatori, sia di maggioranza che di opposizione. Si è parlato oggi di un clamoroso sistema di marchette. Io che non posso vantare nessun successo sul capitolo delle marchette, perché i miei emendamenti sulla Asti-Cuneo e sulle procedure di accesso ai fondi già stanziati per le alluvioni in Piemonte non hanno ricevuto alcuna attenzione, mi sento di dire, a conclusione di questi mesi di lavoro, che i due pilastri fondamentali della finanziaria siano stati rispettati. Il Governo riuscirà a stabilizzare la spesa pubblica,

abbiamo avuto la sensazione di avere un po' raschiato il fondo del barile, le difficili vicende che hanno coinvolto le questioni del fondo universitario, accanto alla positività invece dei 300 milioni annui dati al FIRST, però ci sollecitano e c'inducono a valutare che, quando si parla di fase due, si parla di un urgente e concreto problema.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in quest'Aula per la prima volta e, a parte l'emozione, sento tutto il peso della responsabilità e del ruolo al quale siamo chiamati. Dopo il ricorso alla fiducia votata dalla Camera dei deputati e richiesta anche qui in Senato, questo Governo completa l'opera di scippo effettuata in danno del Parlamento, ma soprattutto in danno dei cittadini italiani, che da questo organo costituzionale sono rappresentati. Gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto hanno già messo in rilievo i palesi limiti e le grandi incongruenze di questa manovra finanziaria; gli stessi limiti e le stesse incongruenze che sono diretta espressione di questo centro-sinistra. Anzi, proprio per quello che abbiamo visto in questi mesi sarebbe più corretto dire di questa sinistra. Una coalizione unita nel nome dell'anti-berlusconismo e impegnata, nel corso della passata legislatura, soltanto a tentare di manipolare l'opinione pubblica per ribaltare ovviamente il grande consenso popolare espresso a favore del presidente Berlusconi e della coalizione di centro-destra. Un'operazione che ovviamente non ha dato i frutti sperati, visto l'esito elettorale che fotografa il Paese in una situazione di sostanziale parità; parità offuscata, tra l'altro, da alcune ombre che occorre chiarire in fretta per evitare che queste elezioni siano annoverate tra le pagine nere della democrazia del nostro Paese. Il provvedimento che oggi ci troviamo di fronte rappresenta una vera e propria stangata per gli italiani; è fin troppo palese che questa finanziaria trasformista e pasticciata sia rappresentata da una nuova eccessiva oppressione fiscale sul sistema Italia, un'oppressione che si tocca con mano nel Paese, che aleggia nelle piazze, nei posti di lavoro, nei bar, tra la gente; una soffocante imposizione fiscale che non tiene conto del fatto che a maggiori tasse corrisponde un blocco dei consumi e, conseguentemente, una minore economia per il Paese. Le motivazioni di questa stangata sono da ricercare esclusivamente in una cospicua serie di spese, spesucce e regalie varie, nascoste nei meandri di questa manovra e dirette unicamente ad accontentare, amici, potentati e gruppi vicini a questo Governo. Basterebbe questo per rendersi conto quale visione strategica del Paese Italia abbia questo Governo. Un Paese che nei cinque anni di Governo precedente ha iniziato una lenta, ma graduale crescita; un'Italia che ha guadagnato ruolo e rispetto nei confronti degli altri Paesi e che oggi subisce un colpo mortale da questa maggioranza. Dal testo della legge finanziaria traspare, infatti, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di questo Governo di tassare tutto e tutti. Abbiamo di fatto una finanziaria che tassa i generi di prima necessità, la casa, l'auto, il ricorso al pronto soccorso; tutti provvedimenti che pesano maggiormente sulle tasche dei cittadini meno abbienti. Una finanziaria che tassa le rendite finanziarie, la successione *mortis* *causa*, ma - cosa ancora più grave - imbroglia gli italiani, facendo finta di dare con una mano, ma togliendo con l'altra. Alla carenza di interventi capaci di produrre benefici e generare effetti duraturi sull'economia del Paese, si aggiunge un'altra grande pecca di questo Governo: la totale assenza di interventi rivolti alla modernizzazione del Paese. Un'Italia che non può e non deve cedere il passo all'Europa e agli altri Stati, e che deve invece saper stare a pieno titolo all'interno di un sistema economico sempre più globalizzato. Una strategia per le infrastrutture del Paese sacrificata sull'altare di quelle frange di maggioranza che trincerandosi dietro un falso ambientalismo si frappongono ad ogni miglioramento della rete infrastrutturale italiana. Resterà vano, dunque, quel desiderio di crescita economica del Mezzogiorno d'Italia così come non avranno nessun esito le speranze di tanti giovani alla ricerca di un lavoro. Colleghi senatori, questa è una manovra finanziaria che non solo «affossa» il sistema Italia nel suo complesso, ma di fatto calpesta anche singoli diritti delle nostre comunità regionali iniziando tra l'altro da quelle che hanno una loro specificità costituzionale. Colleghi, ognuno di noi in quest' Aula è espressione di una regione, di un territorio, di una specificità ed oltre a rappresentare gli interessi dell'intero Paese è portato anche necessariamente a tutelare la propria identità regionale. Ebbene questa manovra finanziaria cancella con un colpo di spugna lo storico patto «solidaristico» tra Stato e regione Sardegna che fu incarnato nello statuto quasi 60 anni fa e del quale oggi non si vuole più lasciare traccia. La Sardegna, con la complicità esclusiva del Presidente della regione, riceve da questa legge finanziaria il più grave affronto alla propria autonomia. Il Governo Prodi, infischiandosene delle condizioni economiche, sociali e storiche della regione Sardegna scarica sulla sua popolazione l'intero costo della sanità pubblica e dei trasporti, compresa la continuità territoriale. Tutto in cambio di un fìttizio aumento del gettito IVA e, cosa ancor più grave, scrivendo la parola «fine» su una legittima vertenza sul pregresso che spetterebbe alla Sardegna per l'errato calcolo dell'IVA e dell'IRPEF dal 1993 al 2006. Colleghi senatori, oggi con questa norma si colpisce in modo letale una regione come la Sardegna. Oggi con questa finanziaria si penalizza l'economia dell'intero Paese, che sotto il peso di nuove tasse non riceve *input* dall'azione del Governo Prodi e da una maggioranza forse più preoccupata ad occupare le «morbide» poltrone dei centri di potere, piuttosto che della crescita del nostro Paese. Una finanziaria, onorevoli colleghi, «messa al bando dai cittadini». Da quella folla di 2 milioni di persone, pensionati, massaie, operai, impiegati, imprenditori, professionisti, giovani, che si è ritrovata in Piazza San Giovanni qualche giorno fa. Due milioni di persone, molte della quali giunte spontaneamente da ogni parte d'Italia per esternare il proprio dissenso su questa finanziaria e sull'operato del Governo Prodi, e alle quali si sommano i cortei di coloro che, in rappresentanza della loro categoria professionale, hanno manifestato pubblicamente il loro disaccordo in questi mesi. Pensiamo agli uomini impegnati nel sistema sicurezza o agli insegnanti. scesi in piazza per denunciare i vizi, le incongruenze e le pesanti penalizzazioni di questa finanziaria. Abbiamo assistito a cortei spontanei, ma soprattutto senza la presenza di quel braccio «armato» di una parte del sistema sindacale che è più impegnato a sostenere il progetto politico della sinistra e la carriera di alcuni di voi che a difendere il lavoro degli italiani. Con molta probabilità non sarà l'Aula a mandare a casa questo Governo, signor Presidente, ma tra poco l'onda d'urto provocata dalla protesta sarà tale e di tale portata che questo Esecutivo non avrà altra scelta se non quella di rassegnare le proprie dimissioni. Vi chiedo, onorevoli colleghi, quale fiducia si possa attribuire ad un Governo e ad un centro-sinistra che non rappresenta più la maggioranza degli italiani, ad un Governo capace di porre in essere tante e tali iniquità; ad un Governo che con la scellerata complicità del Presidente della Regione Sardegna vuole nuovamente vessare il popolo sardo. La risposta è sicuramente nessuna. Nessuna fiducia può essere infatti attribuita ad un Governo capace di riempirsi la bocca di grandi proclami e nel contempo di mettere in atto misure mirate unicamente all'accrescimento delle divisioni sociali e alla negazione dello sviluppo del Paese. Ad un Governo che anzi è costretto a dipendere dal voto decisivo dei senatori a vita e a ricorrere al voto di fiducia per imporre all'Italia le proprie decisioni. È per queste motivazioni, signor Presidente, che voterò contro la fiducia posta dal Governo. Per tutto questo credo che abbia, fin dal primo giorno, rotto l'emozione, perché la fiducia oggi mi ha impegnato molto a portare dentro quest'Aula gli umori e i malumori delle nostre genti.

con questa finanziaria, il problema del rapporto Stato-Regioni, più volte conclamato, subisce una pesante penalizzazione, così come il Titolo V, così come la legge n. 3 del 2001; basterebbe soltanto leggere con attenzione lo sbandierato finanziamento del Fondo sanitario nazionale: 96 milioni di euro nel 2007, 99 nel 2008 e 102 nel 2009. Il tendenziale, più volte sollecitato e reclamato dalle Regioni, era per il 2006, lo dico qui al rappresentante del Governo, di 101 milioni di euro, il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, evidenziato rispetto al 2006, nell'ultimo DPEF, quello che abbiamo approvato qualche mese fa, è superiore rispetto a quanto proposto. C'è da chiedersi, poi, che fine abbiano fatto i crediti pregressi delle Regioni, avendo fatto per cinque anni il Sottosegretario al Ministero della salute, so che era un ritornello fisso quello dei crediti pregressi delle Regioni, che - vedo - qui non trovano più alcun riferimento. È grave, preoccupante e diseducativa l'autorizzazione allo sfondamento senza limiti per le Regioni che non hanno completato il piano di rientro. Lo sfondamento cioè dell'IRPEF e dell'IRAP regionali, già per altro in qualche Regione attuato o in fase d'attuazione, che sicuramente non premia le Regioni più virtuose rispetto a quelle spendaccione. Oltre, quindi, al prelievo nazionale, i cittadini italiani hanno subito e subiranno anche l'aumento di IRPEF e di IRAP regionali, stimato mediamente tra 2.500 e 4.000 euro, come già avvenuto in qualche Regione (cito la Regione Lazio che meglio conosco). Per i piani di rientro regionali sono passati altri otto mesi e nulla è stata fatto rispetto agli impegni che erano stati assunti da parte delle Regioni e si parla ancora, in questa finanziaria, di affiancamento, allora c'è da chiedersi l'affiancamento di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre cosa abbia prodotto, quindi è un rinvio ad anno nuovo. Poi c'è la beffa dell'articolo 20 - l'augurio è che restino in piedi le linee guida sancite con la finanziaria del 2006, quella del precedente Governo - circa il rientro nelle casse dello Stato di soldi che risalgono al 1988, cioè pensate, pensate, è passato quasi un ventennio e non sappiamo ancora quei soldi come siano stati utilizzati, basterebbe andare a vedere come alcune Regioni abbiano utilizzato tali fondi: ci sono Regioni che hanno riutilizzato il 25 per cento dei soldi del 1988. I *tickets*. È stato abolito il codice verde, ma resta il codice bianco, con 25 euro. È ben nota la tendenza di ogni italiano, quando esce di casa, a decidere se deve andare ad un cinema,

sulle aziende farmaceutiche forse anche il 40 per cento prima a carico delle Regioni che non hanno saputo mantenere e controllare la spesa farmaceutica al di sotto del 13 per cento. Basterebbe vedere il precedente emendamento del Governo che non contiene questa formulazione per verificare quanto detto. Che dire poi della chicca contenuta nella finanziaria, dove si legge che i consiglieri referendari medici in servizio presso l'ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono svolgere attività professionali esterne, soltanto del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e sanitario degli Istituti di ricovero e cura? C'è da chiedersi quali prestazioni particolari offrano questi medici della Presidenza del Consiglio e, soprattutto, perché questa esclusione non venga

Qualcuno spera che oltre ai conti correnti anche i cittadini siano dormienti, ma non si faccia illusioni. Per tale motivo, non possiamo votare questa finanziaria. Come dice, giustamente, il segretario dei DS Fassino,

tralascio ogni commento relativo alla tormentata genesi del provvedimento oggi al nostro sommario esame. Essa, tra l'altro, non è stata ancora del tutto definita. Dato

che la battaglia parlamentare della Casa delle Libertà al fine di eliminare l'odiosa tassa di successione per le imprese agricole e, in genere, per le imprese familiari ha avuto un successo almeno parziale. Infatti, non avrebbe avuto alcun senso tassare alla stregua di altri beni patrimoniali fattori produttivi fondamentali per l'esercizio dell'impresa. Il quadro di riferimento comunitario, la maggiore competizione internazionale e altri fattori impongono una sufficiente capacità di investimento da parte degli agricoltori e l'imposizione della tassa di successione avrebbe colpito, se non strangolato, costringendoli ad indebitarsi, proprio i soggetti più attivi e giovani. A tale riguardo, il comma 1071 del maxiemendamento istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Dovremmo quindi rallegrarcene, ma quando poi andiamo a vedere che tale Fondo avrà una disponibilità finanziaria di soli 10 milioni all'anno, ne deduciamo che il Governo Prodi ancora una volta si produce in annunci privi di ogni concreto fondamento: una colossale presa in giro per i giovani agricoltori. Noto, inoltre, che il Governo dedica una certa attenzione al settore dei biocarburanti e delle biomasse. Al di là della fondata impressione di trovarci dinanzi ad una normazione estremamente farraginosa, che rischia quindi di vanificare ogni concreta realizzazione, dobbiamo notare che gli obbiettivi indicativi nazionali contenuti nel comma 367 non si discostano sostanzialmente da quelli indicati dal Governo precedente; in altre parole, non vedo quella particolare volontà innovativa tante volte strombazzata da numerosi esponenti del Governo e della maggioranza. Non vedo soprattutto una reale alternativa di nuove redditualità per gli agricoltori, né una seppur minima creazione di valore aggiunto. Quindi, signori, anzi signore del Governo, vediamo di non spacciare un'iniziativa sicuramente condivisibile di protezione ambientale per quello che non è; protezione ambientale va bene, nuove prospettive per l'agricoltura italiana manco l'ombra, prospettive di lucro notevoli per pochi importatori di semi ed oli vegetali, tra l'altro da Paesi che non si fanno certo gli scrupoli degli ambientalisti italiani in materia OGM. Il risultato è che è lecito prevedere un *trend* in aumento delle importazioni di tali *commodities* vegetali con i conseguenti effetti depressivi per le quotazioni presso le nostre borse merci del prodotto nazionale. Risultato finale, quindi: un'ennesima illusione per i nostri agricoltori, che si traduce, per contro, in notevoli profitti Governo della sinistra - per pochissimi soggetti che nulla hanno a che vedere con l'agricoltura italiana, ma che evidentemente godono di protezione governativa. Ben diverso, invece, è il comma 382, che effettivamente favorisce l'impiego a fini energetici di biomasse realizzate in Italia e, a tale riguardo, mi fa piacere rilevare che il suddetto comma copia integralmente un mio disegno di legge, presentato nei mesi scorsi. In questo caso sono veramente lieto di non accusare di plagio il Governo che, evidentemente, ha ritenuto di far suo ciò che l'opposizione ha individuato come concreta prospettiva economica per il settore; copiate un po' di più e forse avrete qualche fischio di meno. Noto poi che con il comma 1079 il Governo intende fare pulizia etnica dei commissari dei consorzi agrari per procedere ad una lottizzazione tendente a piazzare magari qualche «trombato» alle elezioni ed a completare il noto processo di normalizzazione «sovietica» dei consorzi agrari nell'orbita della Lega delle cooperative. A tale riguardo, spiace dover assistere alla definitiva confisca di strutture private, di proprietà privata degli agricoltori che hanno avuto un'importante funzione al servizio dei produttori agricoli per collocarle nel dominio della cooperazione rossa. Anche di questo ci ricorderemo quando ritorneremo al Governo molto presto. Con i commi 1087 e 1088 la finanziaria passa a considerare i piani nazionali di settore di tutti i diversi comparti della nostra agricoltura, compreso quello forestale. La dotazione finanziaria per il 2007 per tutto ciò, che dovrebbe rappresentare gran parte dell'azione del Ministero, di soli 10 milioni di euro. Vorrei capire se assistiamo ad uno spreco di denaro pubblico, e ciò sarebbe nel caso che questi 10 milioni fossero destinati alla preparazione dei piani nazionali - dato che questo è il lavoro dei dipendenti del Ministero ovvero se il Governo sia realmente convinto di concretizzare tutti, ma proprio tutti, i piani di settore di tutta l'agricoltura italiana con soli 10 milioni di euro; in tal caso, siamo dinanzi ad una spericolata presa in giro degli agricoltori italiani. milioni in più rispetto ai fondi già esistenti vengono poi destinati all'agricoltura biologica - anche questo è un paradosso - che rappresenta sì e no una frazione infinitesimale del tutto. alla conclusione, signor Presidente. Voglio ricordare che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali vedrà aumentare, e di molto, le risorse per il 2007 e ciò in piena coerenza con l'affermazione del partito della spesa di cui il Governo Prodi è vessillifero. Se l'aumento della spesa fosse indirizzato ad un reale sostegno delle imprese agricole e della pesca, non avremmo nulla da eccepire, ma la realtà è ben diversa, dal momento che tali nuove risorse saranno indirizzate verso una crescente burocratizzazione del settore, verso impieghi intraministeriali che non sortiranno alcun effetto positivo per gli agricoltori e i pescatori, che devono affrontare un mercato sempre più difficile. Infine, Presidente, nemmeno un rigo viene dedicato alla pesca professionale. Ricordo che tale settore, che si sviluppa lungo 8.000 chilometri di coste italiane, configura la più importante flotta del Mediterraneo ed è stato recentemente colpito da una disastrosa riforma comunitaria punitiva, che tra l'altro ha avuto il voto favorevole dell'Italia, contumace il Ministro rappresentato da impiegati al Consiglio Europeo. Il Governo di un ex Presidente della Commissione europea era rappresentato, al Consiglio europeo che ha deciso una riforma che uccide la pesca italiana, da due impiegati. Solo per fare un esempio, lo scorso anno per aiutare i pescatori ci inventammo l'IVA agevolata per la pesca: questo Governo l'ha fatta fuori, ha fatto marcia indietro. Voglio vedere se poi la Lega delle cooperative, attraverso la Lega pesca, vorrà protestare: finora non ho sentito alcun tipo di protesta da parte dei rappresentanti rossi dei pescatori, che però ho l'impressione li rappresentino sempre meno. Per tutto questo, e per molto altro ancora, signor Presidente, per il metodo indegno e inadeguato (è il mio giudizio, che, ne sono certo, corrisponde a quello di tutti gli agricoltori e di tutti i pescatori italiani), su questa prima e speriamo ultima finanziaria di Prodi il nostro

questa finanziaria ha ribadito il ruolo marginale dell'agricoltura nell'agenda politica italiana e la sua assenza nelle strategie economiche più importanti del nostro Paese. Di fronte allo spettacolo dalla crisi endemica dell'agricoltura italiana, verrebbe da dire sconsolati, parafrasando Prezzolini: l'agricoltura finisce, ecco quel che resta. Nella campagna elettorale di qualche mese fa non si accennò, né negli innumerevoli interventi propagandistici televisivi né in quelli sulla stampa, ai problemi dell'agricoltura, né il neo presidente del Consiglio Prodi ritenne di dedicare all'agricoltura qualche cenno nel suo primo intervento davanti alle Camere. In linea puramente tecnica, potremmo condividere in buona parte la fiducia del presidente del Consiglio Prodi verso il suo Ministro alla partita agricola, ma la sua palese ed insistita disattenzione verso l'agricoltura, il suo silenzio nelle occasioni istituzionali più significative, non possono non far sorgere sospetti su recondite simpatie verso le tesi antiagricole (né si sa definirle diversamente) espresse ed esternate l'estate scorsa dal professor Giavazzi sul «Corriere della Sera» e da tutti quegli economisti e politici che si battono, con scarsità invero di argomentazioni plausibili, per un ridimensionamento dell'agricoltura, o meglio del suo sostegno finanziario comunitario, che il silenzio di tanti responsabili del settore agricolo indubbiamente sta agevolando. Questa finanziaria, lo si riconosce senza sforzo, non riduce lo stanziamento complessivo per il settore agricolo rispetto al passato ed introduce qualche elemento positivo quale il nuovo impulso dato ai biocarburanti con l'aumento a 250.000 tonnellate del contingente annuo di *biodiesel* defiscalizzzato e senza aggravi in finanziaria. Pur tuttavia, i tanti interventi previsti sono del tutto insufficienti, con una vistosa assenza di coerenti visioni strategiche per affrontare e risolvere definìtivamente alcune carenze fondamentali del settore primario. Quindi, è doverosa una breve ma significativa elencazione. Innanzitutto, viene viene introdotto un obbligo alla commercializzazione dei biocarburanti ma nulla è previsto per rendere più stringente il legame con le politiche agricole delle materie prime. prime. Gli agricoltori attendono che l'opportunità offerta loro dalle bioenergie possa trovare sbocchi concreti ed immediati, anche per decidere se continuare a seminare o chiudere l'attività delle loro aziende e avviare i propri figli verso il triste destino, magari, del precariato.

luogo, l'applicazione del cuneo fiscale in agricoltura è quasi insignificante perché agisce sull'IRAP, poco applicata nel settore primario perché non considera il lavoro a tempo determinato, *magna* *pars* ormai del lavoro subordinato agricolo. per l'incentivazione degli appalti pubblici dei servizi alle imprese agricole e per l'incentivazione della vendita diretta ai consumatori sono previsti importi annui troppo ridotti e, comunque, assolutamente inidonei. Infine, il Fondo per l'imprenditoria giovanile (di appena 10 milioni annui, stanziati per il periodo 2007-2010, per complessivi 50 milioni nell'arco di questi cinque anni) è assolutamente insufficiente e, comunque, riutilizza le stesse risorse già stanziate nel 2004 con il decreto legislativo n. 99. In conclusione, manca negli stanziamenti delle risorse a favore dell'agricoltura una visione strategica complessiva per lo sviluppo dell'impresa agricola. Com'è stato efficacemente affermato, questa finanziaria agricola è un fluorescente caleidoscopio di vecchie e nuove misure, che, però, è difficile che risolvano completamente e definitivamente alcuni degli storici problemi dell'agricoltura italiana.

A quando anche i fischi sonori degli agricoltori a Prodi? Prevedo molto presto. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il dibattito della legge finanziaria si è sviluppato a tutti i livelli con particolare vivacità, sia per l'entità della manovra, sia per le modalità con le quali si è cercato di conseguire i tre obiettivi annunciati (il risanamento, lo sviluppo e l'equità). Devo sottolineare che questo dibattito ha messo a nudo tutti i contrasti e le differenze tra le forze politiche che sostengono la maggioranza la maggioranza ed ha portato alle proteste ed al disagio di molte categorie sociali e produttive. La decisione di presentare il maxiemendamento e di chiedere il voto di fiducia dimostra dimostra in maniera chiara e netta che la maggioranza non riesce ad elaborare un testo condiviso non dico con l'opposizione - si badi bene - ma, almeno, dalle forze politiche che sostengono l'attuale Governo. Quando una maggioranza presenta circa 2.000 emendamenti ad un disegno di legge presentato dal Governo fa pensare che sin dall'inizio vi sia stata la chiara volontà di arrivare a porre la questione di fiducia, creando ad arte l'alibi dell'ostruzionismo parlamentare. I fatti dimostrano che questo è stato attuato dalla stessa maggioranza, non certo dall'opposizione, la quale ha svolto il proprio ruolo in maniera responsabile e costruttiva (basti pensare ai diversi emendamenti migliorativi approvati in Commissione bilancio con il consenso delle forze politiche dei diversi schieramenti). schieramenti). Colgo l'occasione per sottolineare che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio del Senato è stato un'esperienza di grande responsabilità morale, sviluppata con impegno e costanza da parte di tutti i senatori della Commissione stessa, che hanno lavorato senza sosta per ben nove giorni, cercando di

Come è sua tradizione, il Gruppo UDC ha portato avanti una politica di confronto costruttivo e responsabile, per contribuire al miglioramento di questa legge finanziaria. Molti dei nostri emendamenti riguardavano questioni di ordine generale, che avrebbero dovuto trovare il consenso di quasi tutte le forze politiche, anche perché si muovevano nella direzione degli obiettivi su cui la stessa maggioranza aveva impostato la legge finanziaria. Le finalità dell'equità e dello sviluppo sono, ad esempio, alla base degli emendamenti presentati dall'UDC sulla questione del trasporto pubblico locale nella Regione Sardegna. La nostra proposta mirava ad evitare un vero e proprio scippo nei confronti dell'economia della Sardegna e a dare a dare concreta attuazione ad uno dei pilastri su cui si basa la solidarietà nazionale verso l'Isola, in maniera conforme allo spirito ed alla sostanza di tutte le intese stipulate tra lo Stato le Regioni, fondate sul principio che lo Stato concorre con la Regione nel governo

In questo caso si era trovata una convergenza con i componenti di maggioranza della Commissione finanze. E ancora come non riconoscere l'alto valore sociale e morale della proposta che mirava a garantire 1'erogazione di servizi essenziali per i non vedenti, servizi che di fatto vengono tagliati a causa delle disposizioni dettate dal Governo? Oppure parlando di equità, uno dei tre obiettivi cardine che si era posta la maggioranza, come non ricordare la richiesta dell'UDC di ripristinare le indennità di trasferta per i vigili del fuoco al pari di altre categorie di dipendenti pubblici? Per quanto riguarda lo sviluppo, ritengo invece che il Governo ha mostrato uno scarso coraggio nelle previsioni di investimenti in materia di infrastrutture, che sono la condizione primaria per la crescita economica di un Paese. In particolare l'UDC si è fatto promotore di diversi emendamenti al riguardo tra cui in particolare voglio ricordare un ordine del giorno approvato all'unanimità e fatto proprio dal Governo in sede di discussione del cosiddetto decreto Bersani.

e incentrato, in questa fase, sulla sollecita realizzazione della cosiddetta Pedemontana di Formia, attesa da decenni e fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza delle popolazioni di questa vasta area. Opera che, giova ricordarlo, ha concluso ai vari livelli, dal CIPE alla Regione, tutto l'*iter* procedurale ed è già inserita, oltre che nella legge obiettivo sui lavori pubblici, anche tra le dieci opere di prioritario interesse nazionale nella finanziaria dell'anno scorso. Il tratto in Campania risulta già integralmente finanziato e quindi a maggior e quindi a maggior ragione diventa incomprensibile il ritardo relativo alla naturale prosecuzione nel Lazio meridionale. Successivamente, in Commissione, sull'argomento è stato ripresentato l'emendamento all'articolo 18, comma 543-*bis*, a valere sui fondi della legge obiettivo, poi rielaborato e rinominato 545-7*bis*. Purtroppo, tale emendamento non è stato esaminato in quanto i lavori sono terminati poco prima di arrivare a discutere del comma in oggetto. In questo caso, a titolo personale e del Gruppo UDC, esprimo soddisfazione per l'accoglimento di questa proposta all'interno del maxiemendamento. Anche se l'entità dello stanziamento è minore di quanto da noi richiesto in fase emendativa, debbo riconoscere che questa decisione rappresenta un primo passo verso la risoluzione del gravoso problema dei collegamenti stradali tra Regione Lazio e Regione Campania. In conclusione, nonostante l'espresso rammarico per l'andamento dei lavori, desidero affermare che l'esperienza da me fatta quest'anno per la prima volta nella Commissione bilancio con questa finanziaria è un alto momento di responsabilità, che tutti i Senatori dovrebbero affrontare per avere un senso compiuto del proprio mandato, anche se rimane il rammarico in tutti noi di vedere vanificato questo lavoro con la richiesta di fiducia che il Governo ha presentato. Signor